L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto.

verifica del lavoro svolto fino a oggi dal Governo nel confronto con la Commissione europea per quanto riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. di un'occasione anche per fare una verifica sulle differenze in corso tra quanto definito con la terza relazione, che era la prima del nostro Governo, e la quarta relazione, così da poter avere dei punti di riferimento e dei parametri e cercare di cogliere di cogliere gli elementi raggiunti all'interno del percorso portato avanti fino a oggi, ma anche e soprattutto per fare una verifica sugli obiettivi che devono essere ulteriormente raggiunti e che rappresentano l'impegno dei prossimi mesi e anni. La terza relazione della scorsa estate rappresentava, in sintesi, una fotografia di un quadro molto complesso. Eravamo nel pieno dello stato di revisione e verifica degli obiettivi raggiunti sulla terza rata, avevamo una serie di difficoltà nell'ambito della verifica di questi obiettivi e - anche e soprattutto - eravamo alla vigilia di un tema che ha rappresentato uno degli elementi più importanti del dibattito in corso. Mi riferisco alla verifica della revisione del Piano che, come è noto, era uno dei punti centrali dell'azione programmatica del nostro Governo e che ha rappresentato fino a oggi, per quanto ci riguarda, uno dei risultati più importanti anche rispetto al confronto avviato a livello europeo. In questo contesto mi piace sottolineare e ripercorrere quello che all'interno della relazione viene individuato e raccontato rispetto al lavoro che si è svolto nel confronto con la Commissione europea per il raggiungimento degli obiettivi delle diverse rate e gli elementi più qualificanti dell'azione collegata alla revisione. Per quanto riguarda la terza rata, mi piace ricordare come nella fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi fu trovato con la Commissione europea un accordo molto positivo che consentì di spostare uno dei 55 obiettivi della terza rata alla quarta rata e che ci ha consentito, entro il termine previsto, il raggiungimento degli obiettivi e il pagamento della terza rata. Come molti di voi ricorderanno, in quell'occasione ci fu l'intesa che immaginò la soluzione prevista con lo spostamento di uno di questi obiettivi dalla terza alla quarta rata e la riduzione di un importo di 500 milioni di euro

fu l'avvio di una fase nuova dal punto di vista del confronto con la Commissione europea, se è vero come è vero che si decise, in quel contesto, di immaginare un percorso di revisione della quarta rata, ancor prima della revisione complessiva del Piano. Lo voglio sottolineare perché questo ha rappresentato uno degli elementi di assoluta novità nel rapporto con la Commissione europea e soprattutto, a differenza di quanto è accaduto anche per altri Paesi, l'individuazione di questo percorso rispetto alla quarta rata ci ha consentito di modificare una serie di obiettivi all'interno di questa rata e di raggiungere un secondo importante risultato,

Questo ha consentito la risistemazione dell'importo della rata, che ha visto un aumento dai 16 ai 16,5 miliardi poi incassati, e ha consentito al nostro Paese di incassare le risorse relative sia, come ho detto, alla terza, sia alla quarta rata. Pertanto, entro il 31 dicembre dello scorso anno, non solo il Governo ha ottenuto questi due importanti risultati, ma questo ha comportato anche la possibilità di incassare 35 miliardi complessivi che, insieme alle risorse precedentemente ricevute, hanno portato il nostro Paese ad avere un importo di risorse incassate pari a 102 miliardi di euro. Nell'ambito della relazione che è stata consegnata alle Camere, troverete la definizione dettagliata degli aspetti, degli obiettivi, delle modifiche che hanno accompagnato questo percorso e anche e soprattutto delle ragioni propedeutiche rispetto alla quarta rata, che ci hanno consentito di avviare la fase della revisione. Anche qui, dico

una vicenda che è ancora in corso e che in quella fase cambiò complessivamente gli obiettivi e le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè l'invasione dell'Ucraina, con il conseguente aumento del costo delle materie prime. Il secondo è la gravissima crisi energetica che portò in quella circostanza la Commissione europea a individuare soluzioni come, per esempio, quelle relative ad un nuovo importante regolamento, il REPowerEU, che avviava la fase di intervento da parte della Commissione europea rispetto alla necessità di adeguare i Piani nazionali di ripresa e resilienza dei Paesi

non solamente per un dato oggettivo, ma anche per intervenire su alcune altre questioni che sono altrettanto oggettive dal punto di vista del raggiungimento del risultato e sulle difficoltà che emergevano in modo molto chiaro all'interno del Piano. Il riferimento è a una serie di progetti erano stati inseriti all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che mai avrebbero potuto essere rendicontati o spesi nei termini previsti dal Piano. Voglio cogliere l'occasione di questa relazione perché sono passati molti mesi, anche con tantissime polemiche su questo, per definanziato dei progetti, come è stato detto più volte, per scelta. Il Governo ha fatto un'analisi dettagliata nel confronto con la Commissione europea, dalla quale sono emersi alcuni elementi. Il primo ai cosiddetti progetti in essere, quasi 68 miliardi di euro di progetti che erano precedenti al Piano e che, quindi, non avevano nessuno dei requisiti che avrebbero consentito di rendicontarli all'interno del PNRR

dalla quale non si può prescindere perché è la data entro la quale il Piano deve completare i suoi interventi. In questo contesto, è importante sottolineare il lavoro che è stato messo in campo, perché su una parte importante di questi progetti il Governo ha compiuto una scelta molto forte e molto coraggiosa, che è quella di individuare una serie di progetti e spostarli fuori dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, prendendo l'impegno di finanziarli comunque con altre risorse. Questa scelta che abbiamo fatto di mettere fuori dal Piano tali progetti era obbligata rispetto ad una serie di situazioni alle quali ho fatto riferimento. In questo caso, anche se l'ho già fatto in altre circostanze, desidero sottolineare (dato che è ancora oggetto di discussione), il tema degli interventi relativi alle opere piccole e medie rappresenta in modo molto chiaro il senso del lavoro che abbiamo fatto: mi riferisco a una misura di sei miliardi di euro che prevedeva circa un miliardo di euro per interventi sulla viabilità.

Nel decreto-legge n. 19 del 2024, che è incardinato in discussione alla Camera e che sarà oggetto di conversione nei prossimi giorni, all'articolo 1 abbiamo previsto la copertura finanziaria di tutti gli interventi che sono stati definanziati. Anche in consentirmi un chiarimento: noi non dobbiamo giustificare o inseguire la motivazione per la copertura finanziaria. Il Governo ha fatto un lavoro molto positivo ed importante che anche l'Associazione nazionale dei Comuni italiani con dichiarazioni chiare che sono state fatte nei giorni scorsi, mantenendo un impegno molto gravoso che avevamo assunto per coprire gli interventi fuoriusciti dal PNRR. Noi non dobbiamo quindi inseguire una nostra responsabilità. Non vorrei invertire il ragionamento, ma noi abbiamo assunto un onere rispetto a questioni che riguardavano errori oggettivi previsti all'interno del PNRR; abbiamo quindi attuato delle modifiche trovando una soluzione per questi progetti e creando le condizioni, con la revisione del Piano, per recuperare le risorse necessarie a far sì che - ed è un'altra parte importante della relazione che è stata consegnata al Parlamento - potesse nascere il capitolo aggiuntivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè quello dedicato a REPowerEU. Tale capitolo è molto rilevante, sia per le ragioni e gli obiettivi che la Commissione europea aveva indicato, ma anche e soprattutto perché è un dato di fatto oggettivo che il nostro Paese, nell'ambito dell'aumento spropositato del costo dell'energia, si è trovato in una situazione complessa, per la quale anche e soprattutto l'Italia avrebbe dovuto dare una risposta di merito. Non è un caso che all'interno del capitolo REPowerEU siano state fatte delle scelte molto concrete e lungimiranti rispetto al mutato scenario, se è vero come è vero che il Governo ha inserito nell'ambito di questa modifica una cifra pari a oltre sei miliardi di euro per la transizione energetica del sistema delle imprese e lo ha fatto con una serie di norme di indirizzo inserite all'interno del decreto-legge n. 19 del 2024, in via di conversione, che dà attuazione a tutte le modifiche inserite nell'ambito della revisione, oltre ad aver inserito risorse importanti sulle infrastrutture energetiche strategiche del Paese e una serie di scelte nell'ambito della revisione del Piano su settori strategici.

con interventi concreti pari circa 3 miliardi di euro, non sulla spinta dei trattori in piazza che polemizzavano col Governo, ma per una scelta precedente che è stata compiuta a dicembre dello scorso anno nell'ambito di questa revisione, dà l'idea della visione e della lungimiranza nell'ambito della revisione del Piano e anche degli obiettivi che il Governo ha messo in campo rispetto all'attuazione di questo tipo di intervento. Penso che uno dei risultati più importanti nell'ambito della revisione, anche per la valutazione che è stata fatta a livello europeo e per la dimensione del Piano, perché a me piace sottolineare, come elemento molto importante da non dimenticare, che nel confronto con gli altri Paesi, il nostro Paese emerge con *performance* molto positive. Non ce lo diciamo da soli, ma emerge in modo molto chiaro dal rapporto che la Commissione europea ha presentato nei giorni scorsi sugli obiettivi di medio termine, in cui indica l'Italia come il Paese con la migliore

di prendere per intero la quota a debito di 122 miliardi di euro. Mi sembra che questo rappresenti un elemento di riflessione, che ci responsabilizza ancora di più e che dà il senso della revisione del Piano con l'obiettivo chiaro di puntare al miglioramento della qualità della spesa, per intercettare la crescita e creare le condizioni per poter dare una risposta anche sul fronte del rientro del debito. Infatti, a fronte di 194 miliardi di euro complessivi del Piano, dobbiamo ricordare che 122 sono a debito e che in questo contesto

al nostro Paese. Un altro elemento molto importante che nella relazione semestrale emerge e che penso sia doveroso sottolineare in modo ancora più specifico è quello collegato non solamente agli investimenti, che rappresentano

Anche su questo si è fatta spesso una polemica nel dibattito politico, ma le riforme che erano inserite all'interno del PNRR erano 59. Queste 59 riforme sono state non solo confermate, ma in molti casi integrate e rafforzate con degli obiettivi specifici. A questo va aggiunto che per scelta del Governo abbiamo messo in campo un aumento del numero delle riforme, perché la revisione ha comportato sette nuove riforme. Mi piace citarle perché sono sette riforme importanti che implementano l'azione e gli obiettivi del Piano, ma soprattutto sono collegate ad alcuni ambiti molto rilevanti e cinque sono collegate al REPowerEU. All'interno di queste riforme ne voglio citare due in modo particolare, perché sono molto importanti: la prima è il testo unico sulle rinnovabili, che dà coerenza anche agli obiettivi che mettiamo in campo sul fronte degli investimenti nell'ambito della politica energetica del nostro Paese e dell'efficientamento energetico. La seconda è quella delle competenze, perché è inimmaginabile pensare di poter avviare una fase di investimenti così rilevante senza mettere in campo un quadro di investimenti sul fronte delle riforme accompagnandole con le competenze. Questo riguarda le grandi transizioni, in modo particolare la transizione verde sul fronte dell'efficientamento energetico.

Un'altra riforma molto importante sulla quale stiamo lavorando in questi giorni, perché la nuova *milestone* prevede l'obiettivo dell'approvazione di un provvedimento legislativo entro fine marzo (quindi stiamo lavorando su questo in un gruppo di lavoro con le Regioni), è quella della politica di coesione. un altro elemento molto importante, che non rappresenta una scelta del Governo contro qualcuno: basta leggere l'ottavo rapporto sulla coesione della Commissione europea per capire quali sono i livelli di clamorosa criticità nella qualità, nelle modalità e nell'efficacia della spesa delle risorse europee della coesione. In questo contesto abbiamo messo in campo un'azione che punta a creare le condizioni perché ci sia un raccordo tra le diverse fonti di finanziamento, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (risorse nazionali), il Fondo di coesione (risorse europee) e il Piano nazionale di ripresa e residenza. La riforma punta però in modo molto chiaro a stabilire anche una metodologia sul fronte e sul terreno della *governance* per mettere in campo una *governance* che si avvicini agli obiettivi e alle modalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè *target* e *milestone*, ragionare e lavorare sapendo che bisogna raggiungere un obiettivo, sapendo che in assenza del raggiungimento di quell'obiettivo, non c'è la conseguente erogazione del finanziamento. Se questo è vero, come è vero, per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza con modalità che stanno comportando risultati oggettivi, è ancor più vero per quanto riguarda la politica della coesione, in cui, come affermato dalla Commissione europea, i dati e le *performance* non rappresentano certamente dei risultati positivi, per usare un eufemismo. In questo contesto mi piace richiamare tre aspetti molto importanti che nella relazione sono evidenziati e che hanno rappresentato i punti di forza del lavoro che è stato portato avanti in questo periodo. Il primo è la collaborazione con la Commissione europea. Voglio sottolinearlo perché abbiamo creato le condizioni per un livello di collaborazione molto positivo con la Commissione europea, che ha portato ai risultati che sono stati indicati nel percorso che ci ha condotto al raggiungimento degli obiettivi e al pagamento della terza e della quarta rata quarta rata e anche ad un altro aspetto molto importante. Abbiamo infatti raggiunto e presentato, primi in Europa, la richiesta di pagamento della quinta rata nell'ambito delle previsioni dei 52 obiettivi in essa contenuti, che abbiamo fatto entro dicembre dello scorso anno. anno. Questo ci porterà ora, e vi stiamo lavorando, alla definizione della verifica con la Commissione europea del raggiungimento degli obiettivi e all'erogazione, alla conclusione di questo percorso, della quinta rata, per un importo pari a 10,6 miliardi miliardi di euro. Abbiamo messo in campo lo stesso lavoro nell'ambito del 2024, con la prima cabina di regia che si è riunita con l'obiettivo di pianificare il lavoro comune per quanto riguarda la sesta e la settimana rata, che sono i due obiettivi

ci sono state molte dichiarazioni e molte polemiche sul modello di *governance* che il Governo decise di assumere ad inizio legislatura. Cosa abbiamo fatto con la *governance*? Non abbiamo stravolto nulla. Abbiamo esattamente predisposto un modello di *governance* analogo a quello della Commissione europea. Se è vero, come è vero, che la Commissione europea ha una *task force* presso la sua Presidenza, che si raccorda con tutte le direzioni generali per verificare l'attuazione e la capacità o meno degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi, noi abbiamo predisposto un meccanismo analogo con una struttura di missione presso Palazzo Chigi. Tale struttura non accentra nulla, ma serve a semplificare il lavoro, in perfetta sintonia con tutti gli enti attuatori, beneficiari dei finanziamenti, a partire da tutte le amministrazioni centrali che, come noto, sono organizzate con le unità di missione dedicate all'interno del proprio Ministero e con tutto il sistema delle autonomie locali, con le Regioni e gli altri enti attuatori. Tutto ciò al fine di mettere in campo un meccanismo che ha comportato degli effetti che rivendichiamo, perché hanno rappresentato rappresentano risultati oggettivamente positivi per il nostro Paese, ancor prima che per un Governo o una parte politica. Questo è il tema sul quale voglio soffermarmi cogliere il secondo elemento importante che ha rappresentato uno schema molto positivo di lavoro comune in questo periodo. All'interno della *governance* noi abbiamo previsto e rafforzato molto il ruolo della cabina di regia.

rispetto al decreto-legge n. 19, sull'attuazione del PNRR, con tutte le organizzazioni di categoria e le parti sociali abbiamo avuto un confronto preventivo, ascoltando precedentemente i suggerimenti. Anche le audizioni di questi giorni confermano questo lavoro molto positivo. La cabina di regia ha rappresentato e rappresenta un momento e un modello di lavoro molto positivo per rafforzare e anche per cogliere le criticità e correggerle in corso. È evidente infatti che il Piano nazionale di ripresa e resilienza non è uno strumento che può essere statico e che vede l'approvazione di un provvedimento. Noi ci rivedremo spesso, non solamente per le relazioni semestrali e per gli aggiornamenti, ma molto probabilmente per un aggiornamento complessivo. Questo perché un piano di tale rilevanza ha bisogno di un adeguamento costante in funzione di dati oggettivi, come ho fatto in riferimento alla grave crisi energetica, ma anche in base alle esigenze di adeguamento degli interventi finalizzati all'interno dei singoli programmi, soprattutto per la scelta che il Governo ha fatto, all'inizio della legislatura, di mettere in campo in modo coordinato le diverse fonti di finanziamento, e quindi il Fondo per lo sviluppo e la coesione del PNRR, che, nelle raccomandazioni di luglio, la Commissione europea ha indicato come una priorità agli Stati membri. A me fa piacere sottolineare che questa

al ruolo della cabina di regia, che ha rappresentato uno strumento importante e che sicuramente, nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, sarà molto rilevante. Anche all'interno del decreto-legge n. 19, infatti, abbiamo avuto modo di cogliere suggerimenti opportuni da parte del mondo delle categorie produttive e delle parti sociali e, all'interno del provvedimento, abbiamo ritrovato questi suggerimenti, così da migliorare la qualità e l'efficienza della messa a terra dei progetti. Infine, penso sia importante fare due ulteriori riflessioni. La prima è collegata al tema del confronto con gli altri Paesi, al quale facevo riferimento poco fa. Dal rapporto di medio termine che la Commissione europea ha presentato emerge, come fatto positivo,

non è solamente una presa d'atto positiva, ma è uno stimolo a proseguire in questa direzione. È la conferma che il lavoro che si è messo in campo fino ad oggi è positivo. Non è sufficiente, c'è da fare ancora molto e c'è da lavorare molto, ma c'è un altro aspetto che mi piace sottolineare, che evidenzia il miglioramento e il cambiamento di approccio e di *sentiment* intorno al PNRR italiano. Mi riferisco alla relazione della Corte dei conti dei giorni scorsi, dalla quale emerge in modo molto chiaro un elemento di grande novità. *(Applausi)*. È vero che abbiamo discusso per mesi della precedente relazione della Corte dei conti, ma con una omissione molto particolare, perché quella relazione si riferiva al primo semestre del 2023 e prendeva come riferimento i dati del febbraio 2023. Abbiamo aperto un dibattito su quella relazione, come se vi fosse una responsabilità da parte del Governo,

il raggiungimento dei *target* degli obiettivi all'interno del Piano viene riconosciuto in modo molto chiaro e si indica, sia nella parte conclusiva della relazione semestrale, ma anche nelle mie comunicazioni questa mattina, la parte relativa alla spesa. Anche in ambito, non possiamo ragionare in ottica di spesa del PNRR come se ci fossero condizioni differenti rispetto al pregresso. Facciamo una valutazione e una premessa di carattere generale: la spesa relativa ai primi due anni del Piano è stata pari a 24 miliardi di euro. La spesa del 2023 è stata superiore a 21 miliardi di euro.

facciamo poi un'altra considerazione molto importante e rilevante: all'interno della spesa vi sono due fattori molto rilevanti ed importanti. Il primo è quello collegato al fatto che, con il decreto-legge poniamo un rimedio importante in questo senso. Molti degli interventi che sono stati attivati non vengono caricati rapidamente o contestualmente all'interno della piattaforma ReGis. quindi verosimile pensare che, a fronte degli oltre 45 miliardi di euro di spesa, ci siano molti interventi che non sono conteggiati in tale cifra. Quanto Quanto previsto all'interno dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del corrente anno, cioè la responsabilizzazione collegata al rispetto dei termini e alla necessità di caricare i dati, notevolmente da qui a breve quella spesa. La seconda considerazione, molto importante, è collegata alle modalità di spesa. Se è vero che nei primi anni le spese erano individuate per obiettivi molto collegati a ciò che rappresentava un passaggio tra l'esperienza di Governo, i progetti in essere e ciò che era previsto all'interno del Piano, oggi invece andiamo su una spesa vera. Essa ha le sue complessità, non c'è dubbio, però è anche

ad esempio molti degli interventi infrastrutturali, soprattutto medi e grandi, hanno completato la fase di progettazione e di gara e inizieranno ad avviare una fase di spesa che sarà sicuramente maggiore rispetto a quanto previsto. È quindi evidente che in questo contesto

trarre utili spunti di valutazione anche rispetto alla valorizzazione del dato di spesa del nostro Paese. Detto questo, sottolineo che il decreto-legge n. 19 e la revisione del Piano puntano ad una forte accelerazione della spesa. spesa. Basti pensare alle risorse che abbiamo previsto sul fronte della revisione del Piano - oltre 12 miliardi di euro inseriti per il sistema delle imprese - o agli automatismi previsti, cioè il credito d'imposta nell'ambito della revisione e le misure sui contratti di filiera nel campo dell'agricoltura. Quella

Dobbiamo tener conto sempre di una scelta, ossia di aver utilizzato al cento per cento la quota a debito del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per poter rientrare, la qualità della spesa e la crescita sono elementi fondamentali. In questo contesto previsto all'interno della relazione semestrale una specifica valutazione di tutto ciò che è accaduto fino al momento dell'approvazione del decreto-legge È chiaro che la parte relativa a tale decreto, quindi alla copertura degli interventi usciti dal PNRR e a tutte le norme previste all'interno di questo decreto sul fronte dell'accelerazione della spesa, non è inserita all'interno della relazione semestrale, perché detto decreto è stato approvato successivamente alla predisposizione della relazione semestrale. È evidente che siamo in giornate nelle quali i due temi saranno inevitabilmente collegati: domani mattina sarò alla Camera per riferire anche in quella semestrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza e domani pomeriggio inizierà l'*iter* approvativo in Commissione bilancio alla Camera del decreto-legge di attuazione delle modifiche e della revisione del Piano. Mi Mi piace sottolineare un elemento importante. Per la predisposizione di questo decreto-legge abbiamo lavorato per individuare norme che venissero condivise non solamente con i principali attori e protagonisti del sistema istituzionale, sociale e imprenditoriale del nostro Paese. Abbiamo infatti svolto anche un lavoro preliminare di confronto con la Commissione europea. Voglio sottolinearlo anche in questa sede, perché ha rappresentato e rappresenta un metodo di lavoro che ci ha consentito fino ad oggi di raggiungere questi risultati e sono convinto possa essere un metodo molto importante e positivo anche per gli obiettivi successivi. In questo contesto penso che sia importante valorizzare i risultati raggiunti, che sono oggettivi; non adagiarsi su questi risultati; tenere molto alto il livello di tensione nella fase di attuazione del Piano; individuare con chiarezza gli obiettivi per tempo; lavorare non inseguendo il singolo obiettivo della singola rata a qualche giorno dalla scadenza, ma programmando per tempo. È quello che stiamo mettendo in campo sapendo che gli obiettivi complessivi, il raggiungimento della spesa e soprattutto la fase collegata alle riforme possono rappresentare per il nostro Paese, ancor prima che per il nostro Governo, una prospettiva sulla quale dobbiamo iniziare a interrogarci. Un altro elemento che inizia ad emergere, che abbiamo più volte sottolineato e che dev'essere oggetto del dibattito in atto sul PNRR, è che molte misure e molti investimenti sono stati previsti all'interno del Piano nazionale non hanno un dopo. È importante sottolinearlo, perché è fondamentale avere esattamente lo stesso approccio che abbiamo avuto per la correzione e la revisione del Piano e per la soluzione per il finanziamento degli interventi usciti dal Piano, anche rispetto a una serie di riforme e misure che hanno previsto la copertura finanziaria con le risorse del PNRR fino a giugno 2026. Questo vale per settori fondamentali, dalla giustizia alla sanità - per fare due esempi particolari - sui quali è necessario che questo Parlamento, oltre a questo Governo, partendo da una riflessione originaria, cioè da quando sono stati inseriti questi obiettivi, individui le soluzioni per dare stabilità e quindi rendere efficace il percorso di riforme e di investimenti che stiamo portando avanti.

positivo per il nostro Paese. Concludo questo mio intervento introduttivo con una considerazione che ho fatto più volte e che mi piace sottolineare: il PNRR italiano non è solamente il più grande PNRR d'Europa, anche la grande scommessa del Next generation EU. Se è vero, come lo è, che un PNRR così grande e così complesso ha l'obiettivo di dare una risposta all'attuazione del Next generation EU, vi è interesse analogo e fondamentale da parte della Commissione europea, perché la riuscita del PNRR italiano è la riuscita del Next generation EU e quindi di un modello di finanziamento sul quale nei prossimi mesi e anni si giocherà molto della prospettiva europea. In questo contesto, è molto importante però anche gli elementi di valutazione nazionali. Si sottolinea il fatto che ci sono 122 miliardi di euro a debito, cioè la quota totale quota totale del PNRR, e che al momento solo sette Paesi (tre inizialmente, gli altri a ridosso del REPowerEU) hanno individuato forme di finanziamento aggiuntivo con l'indebitamento: questo è un tema di riflessione - e non di polemica

oculatezza. Lo dico perché magari altri Paesi hanno fatto scelte completamente diverse e, più che convincerci che noi siamo stati più bravi di tutti, cerchiamo di interrogarci sul perché, per esempio, tutti gli altri Paesi non abbiano utilizzato questo strumento con tali modalità. Apriamo una riflessione serena, per cercare di capire come sia necessario il lavoro che abbiamo messo in campo per migliorare la qualità della spesa, tenendo a mente sempre la rilevanza e l'importanza di quella quota di debito. le condizioni sulle quali noi stiamo lavorando. Questi sono i temi che hanno visto l'impegno da parte del Governo; un impegno non semplice, ma che sono convinto abbia portato risultati molto importanti; un impegno al quale mi auguro che anche il dibattito odierno in questo Parlamento possa offrire spunti utili e positivi per migliorare ancora di più il nostro lavoro.

Ogni giorno leggiamo dati e notizie, anche da fonti accreditate, che certificano questo fallimento e, nonostante tutto, il Governo continua a fare solo propaganda, mentre la realtà parla di ritardi, buchi e continui rinvii. Recentemente anche la Corte dei conti, a proposito dell'attuazione

Dopo i tagli drammatici ai progetti per i Comuni, gli asili e la sanità, state insabbiando anche l'attuazione dei progetti ancora in essere. È notizia recente il grido di allarme lanciato dalle Regioni - unanime, al di là dell'appartenenza politica - perché a rischio ci sono i nostri ospedali. La Commissione salute della Conferenza delle Regioni ha chiesto un incontro urgente al ministro della salute Schillaci contro il taglio di 1,2 miliardi di fondi del PNRR relativi prevalentemente a opere per la sicurezza delle nostre strutture ospedaliere. *(Applausi)*. È un taglio definito inaccettabile. Gli assessori regionali sostengono - e li cito - che è surreale che dal PNRR che nasce dalla pandemia vengano tolti soldi alla sanità. Da settimane leggiamo di un nuovo decreto per accelerare la spesa delle risorse del Piano che non riesce a vedere la luce per incapacità e tensioni interne alla maggioranza. A causa di questo, l'Italia rischia di non riuscire ad attuare progetti già previsti per migliorare servizi essenziali come istruzione, sanità, trasporti e riqualificazione urbana. Sono mesi che i Comuni e gli enti locali attendono risposte precise, ad esempio sui 10 miliardi cancellati nell'ultima rimodulazione, mentre continuiamo a verificare dati sull'attuazione del PNRR davvero preoccupanti, che dimostrano come il Governo, fino a oggi, sia stato del tutto inadeguato al riguardo. Il 75 per cento delle opere monitorate dalla piattaforma ReGis registra un ritardo e solo il 7,4 per cento dei fondi del Piano previsti per il 2023 è stato correttamente utilizzato (sono dati Openpolis). Più va avanti la fase di messa a terra del *recovery*, più emergono lacune e incompetenze di questa destra che è capace di scaricare responsabilità sugli enti locali, peraltro sotto organico e senza le energie che servirebbero. *(Applausi)*. Per colpa del Governo - lo dico molto convintamente, Ministro - l'Italia rischia di mancare un'occasione storica. Mostrate continuamente quasi una sorta d'insofferenza antieuropeista alla gestione e all'attuazione del Piano. Ministro Fitto, glielo voglio ricordare sommessamente e in sintesi: oggi l'Italia ha a disposizione le risorse del Next generation EU non per meriti vostri. Avete creato un clima politico di sfiducia Avete creato un clima politico di sfiducia e tensione passando mesi non ad attuare il Piano, ma ad annunciare di volerlo cambiare, paralizzando così tante amministrazioni nazionali e locali. A questo caos politico avete aggiunto errori tecnici che hanno paralizzato l'attuazione, presi dall'ossessione dell'accentramento dei poteri e per lo smantellamento dei controlli esterni. Avete perso più tempo a centralizzare le gestioni delle riforme che ad accelerare la spesa delle risorse stesse e le conseguenze sono evidenti. L'esame della quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano non può certamente ritenersi concluso con le sue conclusioni di oggi, Ministro. Serve che il Governo e la maggioranza - e più nello specifico i Presidenti delle

addivenire all'espressione di un atto di indirizzo frutto di un approfondimento serio e rigoroso, che può avvenire solo a valle dell'esame della quarta relazione e non a monte, come si pretende di fare tramite la comunicazione del Ministro in Aula. Serve che gli esiti del lavoro delle stesse Commissioni siano sottoposti all'attenzione dell'Assemblea per dare spazio a un dibattito il più ampio e partecipato possibile, che dovrebbe interessare tutto il Parlamento. Questo vi chiediamo e questo era il percorso che era stato immaginato sin dalla fase di predisposizione del Piano, che è continuamente delegittimato. Se andiamo a vedere gli atti d'indirizzo presentati dai parlamentari di Fratelli d'Italia quando sedevano ai banchi dell'opposizione durante i Governi Conte II, prima, e Draghi, dopo, è paradossale notare come abbiano chiesto un sempre maggiore impegno da parte del Governo nel coinvolgere il Parlamento, che pure veniva già diffusamente coinvolto. Lo dimostrano le norme che tanto nel decreto *governance,* quanto nella legge di delegazione europea, prevedemmo a tutela del ruolo del Parlamento, che che l'opposizione dell'epoca giudicava evidentemente non sufficienti e delle quali oggi nessuna viene effettivamente garantita. Questo chiediamo al Governo a partire dalla nostra risoluzione: un impegno affinché le prerogative del Parlamento siano pienamente ed effettivamente prese

Parlamento per decidere quali progetti cancellare, quali mantenere e quali aggiungere, semmai anche facendo una valutazione di impatto su di essi. Concludo, signor Ministro, ribadendo con forza la convinzione che il PNRR sia non proprietà privata di una parte politica o di un Esecutivo, ma patrimonio dell'intero Paese. Quando lo sarà anche per tutta la destra, allora avremo compiuto finalmente quel passo significativo nell'interesse esclusivo dell'Italia e dei cittadini.

in Europa e per l'Europa, ed è l'elemento centrale della relazione del ministro Fitto, che ringrazio veramente in modo profondo anche per la sua partecipazione, anche attraverso il sottosegretario Siracusano, a tutti i lavori della Commissione e per la disponibilità a fornire sempre nuovi elementi con la sua *task force* ai lavori in Commissione e in quest'Aula. Le mie espressioni sono ancora più rimarcate, doverose e sentite dopo l'intervento che ho appena ascoltato da parte di un'autorevole senatrice del Partito Democratico, nei cui confronti - la senatrice Rojc lo sa perfettamente - nutro una sincera stima e

Questo è il senso. Il Senato è oggi chiamato a esprimersi, signor Ministro, sulle relazioni del Governo e quindi sulla proposta di risoluzione di maggioranza relativa allo stato di avanzamento del PNRR. Il presidente Giorgia Meloni, nella premessa alla relazione sullo stato di attuazione del PNRR, ha detto: «È un lavoro di squadra, che sarebbe impossibile senza la capacità, la determinazione e la competenza dei tantissimi servitori dello Stato che ogni giorno

nell'interesse della Nazione, per il progresso, il benessere, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini italiani. Nell'ottobre del 2023 questa difficilissima sfida, che è certamente definibile come epocale per uno Stato membro dell'Unione come il nostro, con un *record* non proprio smagliante nella gestione dei fondi comunitari, appariva a molti, dentro e fuori dai confini nazionali, come una sorta di missione impossibile a causa dell'asserita impreparazione del nuovo Governo, delle sue inadeguatezze, dei suoi rapporti inevitabilmente infelici con l'Europa, delle sue sbagliate impostazioni e delle sue divisioni di metodo e di volontà politica. Tutto il catastrofismo che sentiamo ancora oggi in quest'Aula si è rivelato assurdo e sbagliato nei fatti,

Non erano, quindi, questi catastrofismi che ci preoccupavano, perché anche per osservatori imparziali il PNRR rappresentava una terra incognita, dopo il Covid e la criminale aggressione russa all'Ucraina; era effettivamente una terra incognita per l'ampiezza degli interventi che dovevano concentrarsi in un arco temporale brevissimo, interventi anche finanziari e di vasta portata, con tutta una serie di riforme importantissime per il futuro del Paese, che lei, signor Ministro, ha appena descritto appena descritto nel dettaglio. L'Italia ha raggiunto a pieni voti il traguardo posto a metà del percorso, con la quinta rata sulle dieci previste, con l'acquisizione di 101,9 miliardi di euro su 194,4 e - non certo da ultimo - non certo da ultimo - con l'evidente e costante rafforzamento dei propri rapporti con l'Unione europea nel suo insieme e il continuo rafforzamento della propria credibilità, con la netta affermazione della fiducia che viene data al Governo Meloni a livello europeo e globale. Quello di oggi è un voto che impegna il Governo a procedere con determinazione e coerenza. L'abbiamo ascoltata, signor Ministro, e continueremo ad ascoltarla durante i lavori del Parlamento nei prossimi mesi.

ci siamo ritrovati ad avere costi triplicati, per di più con l'incremento delle materie prime. Come se non bastasse, a ciò si è aggiunta la consapevolezza di un enorme buco nero nella nostra economia e nel nostro bilancio, quello

o tre, ma addirittura quattro manovre finanziarie, quanto a dimensione dell'esborso che avrebbe comportato. È una mossa che ha alzato follemente i costi di costruzione, gravando ancor più di quanto si pensi sulla nostra economia. Il Governo Meloni, tuttavia, ha saputo rispondere prontamente: ha cercato nuove rotte per l'approvvigionamento dell'energia, diversificato le fonti, riconsiderato sussidi e *bonus* edilizi, promosso

di coesione, fondi europei e fondi del PNRR. Questi risultati ci portano a considerare l'impervia salita compiuta sino ad oggi se non come l'inizio di una facile discesa, perlomeno come la possibilità di avere davanti una pianura sulla quale procedere più celermente. Ieri il presidente del Consiglio Meloni ha ricordato a Bolzano l'importanza dello strumento parallelo al PNRR, i fondi di coesione, fondamentali per alleviare disparità fra Nord e Sud e interne a ciascuna Regione. Basti un dato: per il ciclo di programmazione 2014-2020 erano disponibili 126 miliardi di euro; in quei sei anni, su 126, ne sono stati spesi soltanto 47, nemmeno la metà. E poi ci vengono a raccontare che le nostre politiche aumentano la disparità e le diseguaglianze fra Nord e Sud. Il Governo italiano, dal primo giorno del suo insediamento, ha avviato un dialogo costruttivo con tutte le Regioni italiane e questo è stato un altro elemento che lei ha appropriatamente valorizzato: il cambio di metodo non soltanto con l'Europa, ma con tutte le realtà, gli enti locali, le Regioni, i Comuni e gli ambienti imprenditoriali e sindacali, con i quali si è proceduto a creare una dinamica veramente nuova e positiva. Sedersi costruttivamente al tavolo dei Consigli dei ministri dei vertici europei e avere il coraggio di riformare incisivamente il PNRR: è stata questa la chiave del successo.

per l'attualità di quello che è il PNRR oggi. In effetti, la Corte dei conti in alcuni passaggi definisce virtuoso il percorso compiuto, quindi erano indispensabili quest'ampio processo

nella ricerca e nella scuola, per portare veramente un'Italia nuova nell'Europa e credibilità e fiducia solide per il percorso che abbiamo davanti. Vi ringrazio quindi, signor Ministro e sottosegretario Siracusano,

come più volte ribadito da Italia Viva, il PNRR non appartiene a una maggioranza, ma è stato aggiudicato da precedenti Governi con altri Presidenti del Consiglio, in particolare il presidente Draghi, e sarà gestito in gran parte

Lei, per esempio, ha ricordato prima che nei due anni precedenti sono stati spesi 24 miliardi e 21 nel 2023, forse perché nei due anni precedenti c'era la parte di progettazione e oggi è arrivato il dunque,

estremamente mortificato dalla pandemia, che aveva dimostrato carenze strutturali pazzesche. Non sono fondi comuni e non sono neanche i fondi europei che siamo abituati a vedere. Sono fondi che servono a rilanciare economicamente un Paese:

Quando lei dice che abbiamo rimandato indietro alcuni progetti e alcuni fondi e li sostituiamo con altri fondi europei non è la stessa cosa, innanzitutto perché gran parte dei fondi che voi avete rimandato indietro riguardano per esempio la transizione ecologica. Noi possiamo anche discutere e convenire con voi che probabilmente alcuni dei progetti e delle visioni europei del *green new deal* erano eccessivi; però rimodificare la rete energetica e dare un ampio respiro alla transizione energetica del nostro Paese, che ha dimostrato la sua insufficienza proprio con la crisi in Ucraina e con il caro energia, fa bene al Paese. Far ritornare indietro quella parte di fondi, come tutta la parte sul dissesto idrogeologico, ci ha profondamente colpito. Rimaniamo però nei temi che lei ha sottolineato con grande vigore.

vengono spese le risorse. Sarò rapida nel concludere i miei cinque minuti di intervento. Voi avete cambiato la *governance* del PNRR, assumendovene la responsabilità. Secondo me, non è stata accelerata la messa in campo dei progetti, ma si è complicata e sono stati allungati i tempi. Soprattutto però è vero che storicamente le Regioni non riescono a spendere i soldi europei

è molto di più; è la nostra mappa per rinnovare l'Italia, puntando su riforme e investimenti che cambieranno il nostro domani, ed è la testimonianza dell'impegno del nostro Paese a rinnovarsi, a investire nel suo futuro e a promuovere una crescita sostenibile. Anche secondo Gentiloni, il Piano europeo, di cui il nostro PNRR è buona parte, potrebbe far crescere il PIL fino all'1,4 per cento. È un'opportunità d'oro per la nostra economia. Ministro Fitto, lei oggi ci ha aggiornato sul cammino fatto e su quello che ci aspetta. Parliamoci chiaro: chiaro: ha detto che, senza le scelte strategiche fatte da questo Governo, certi traguardi del PNRR sarebbero stati irraggiungibili. Abbiamo affrontato un mondo che cambiava velocemente, passando dalla pandemia fino alle crisi energetiche, alle guerre e alle tensioni geopolitiche e siamo stati all'altezza delle situazioni. Rimodulare il PNRR è stata non una passeggiata, ma una risposta coraggiosa che ha mantenuto l'Italia sulla strada dello sviluppo. La Corte dei conti - come lei sottolineava certificato i risultati. Abbiamo raggiunto gli obiettivi, abbiamo firmato convenzioni con i soggetti attuatori ed effettuato anche i trasferimenti di somme a titolo di anticipazioni; un lavoro prezioso per il futuro dell'Italia. È stato evidenziato dalla stessa Corte dei conti

dalla senatrice Fregolent - ma addirittura sono state facilitate tutte le operazioni. Questo processo di revisione è un chiaro esempio di un Governo che non solo reagisce alle sfide, ma addirittura le anticipa anticipa e che ha operato scelte decisive affrontando con coraggio anche e soprattutto lo scetticismo. Quando è stato chiaro che alcuni progetti non sarebbero stati realizzabili nei tempi previsti, si è presa la decisione strategica di riallocarli, garantendone comunque il finanziamento attraverso altri canali. Questa mossa non solo ha salvaguardato l'efficacia del PNRR, ma ha anche consentito di non sprecare un euro delle risorse a nostra disposizione. Le somme non sono tornate indietro - come diceva la collega Fregolent ma addirittura siamo riusciti ad utilizzarle tutte, anche quelle che purtroppo saranno a debito per l'Italia, senza sprecare un euro. Molto utile è stata in questo senso la creazione di sinergie tra il PNRR e altri strumenti finanziari europei, come il Fondo sociale europeo e il Fondo per lo sviluppo e la coesione, per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili. Lo stesso presidente dell'ANCI Decaro qualche giorno fa ha espresso la soddisfazione dei Comuni per il decreto PNRR che recepiva tutte le richieste, assicurando che nessun cantiere ci fermerà: quindi approvazione dei finanziamenti per il rinnovo degli asili nido, digitalizzazione e avanzamento dei lavori in molte delle città metropolitane come segni di progresso. Abbiamo anche imparato a essere più flessibili: tagliare la burocrazia, per finire in tempo i lavori. Una delle nostre maggiori vittorie - come sottolineava anche lei - è il dialogo aperto con l'Unione europea, che ha portato ad un incremento significativo delle risorse finanziarie disponibili, con l'aggiunta di circa tre miliardi, successivamente arricchite anche di altri 3,5 miliardi con il recente decreto. Questi numeri sono la prova tangibile della fiducia riposta in noi dall'Europa e anche della nostra determinazione a utilizzare queste risorse per il bene del Paese. Il Sud ha ricevuto una particolare attenzione nel Piano. La sua sensibilità verso le Regioni meridionali, ministro Fitto, ha ispirato azioni concrete, volte a ridurre il divario di sviluppo e a promuovere un'equità territoriale, con l'obiettivo di trasformare il Mezzogiorno in un terreno fertile per l'innovazione, l'istruzione e lo sviluppo sostenibile, investendo in infrastrutture digitali e salute, per garantire che il Sud possa sfruttare appieno il suo potenziale. La creazione della zona economica speciale (ZES) unica rappresenta un passo fondamentale verso l'integrazione e lo sviluppo economico di quelle Regioni. Investimenti mirati, infrastrutture rinnovate e rilancio dell'industria locale sono solo alcuni dei benefici che la ZES porterà, promuovendo l'equità territoriale ed offrendo nuove opportunità di crescita. La modernizzazione del Paese è in pieno svolgimento, con progetti che spaziano dal digitale all'istruzione, all'energia verde. Questi sforzi sono il fulcro di una strategia che vede il PNRR non solo come un piano di recupero, ma anche come un trampolino verso il futuro dell'Italia. Anche i Ministri di Forza Italia sono stati molto interessati stimolati da quello che è previsto nel PNRR, rilanciando anche i suoi campi, con riforme ordinamentali. Tuttavia, la strada verso la completa attuazione del PNRR non è esente da ostacoli, fra cui la necessità di superare l'eccessiva burocrazia e di garantire una gestione efficace e trasparente dei fondi con la concreta realizzazione delle opere, perché, ad oggi, abbiamo solo le anticipazioni. La risposta a queste sfide si manifesta attraverso misure concrete, come il potenziamento dei controlli, l'eventuale commissariamento dei Ministeri in ritardo con le opere e l'introduzione di sanzioni per evitare ulteriori ritardi. So che c'è scetticismo: molti hanno detto che non ce la faremo e che è tutto un *bluff*, invece guardate dove siamo; abbiamo superato le tappe richieste dall'Europa, abbiamo già ricevuto 102 miliardi dei 194 previsti e siamo addirittura i primi Di fronte allo scetticismo e alle sfide, il Governo ha risposto con risultati concreti. Finora l'Italia è riuscita a centrare e persino a superare le aspettative dell'Unione europea, ottenendo ulteriori finanziamenti,

L'azione del Governo nel contesto del PNRR è una dimostrazione di *leadership* e responsabilità, perché il Piano non è solo un piano di finanziamenti, ma è anche una visione per il futuro dell'Italia. Non è un mucchio di carte, ma è una cosa viva, che sta cambiando il nostro Paese in meglio. Il lavoro svolto sta fornendo inoltre un modello replicabile per la gestione efficace dei fondi europei nel futuro, con particolare attenzione alla trasparenza, all'efficienza e alla partecipazione Guardiamo al futuro. Il PNRR non è - come diceva prima una collega - proprietà privata. Abbiamo nelle nostre mani un'occasione d'oro ed è il momento di mettere da parte le divisioni, di unirci e di spingere tutti nella stessa direzione. Questo Piano è la nostra *chance* per rilanciare l'Italia, per renderla un Paese dove ognuno può trovare le opportunità per realizzarsi, dove l'innovazione e l'inclusione sono non solo parole, ma anche fatti. Dobbiamo prendere questo momento, farlo nostro e lavorare insieme con passione e determinazione per il bene dell'Italia e di tutti i cittadini. Andiamo avanti insieme, signor Ministro, per scrivere questa nuova pagina nella storia del nostro Paese.

perché, effettivamente, il PNRR è una risorsa non di questa maggioranza, ma una risorsa fondamentale per il Paese, che oltretutto è arrivata grazie al presidente Giuseppe Conte, quindi lo sentiamo come una nostra responsabilità ed è per questo che ci rendiamo conto di quanto sia delicata la sua realizzazione e di quanto sia fondamentale, *in primis*, non sprecare neanche un centesimo e, in seconda battuta, che tutto venga realizzato nei tempi e nei modi previsti. Su questa seconda parte mi spiace dover constatare che siamo ben lontani dal punto in cui dovremmo essere. Mi spiego meglio.

dopo gli effetti devastanti sull'economia italiana dovuti al *lockdown* e alla pandemia. Siccome la più grave fragilità che avevamo notato - e che penso fosse sotto gli occhi di tutti - era era l'inadeguatezza del nostro sistema sanitario nazionale, si è deciso di investire una gran parte delle risorse proprio per rafforzare le strutture prevalentemente territoriali, che erano state l'anello debole della catena durante la pandemia. Purtroppo, già nella stesura successiva, i 20 miliardi previsti divennero poco più di 15,5. Va bene, possiamo anche capire il perché,

tutti. Noi siamo sinceramente preoccupati, ma vedo un po' meno preoccupazione da parte di chi invece in questo momento ha l'onere e l'onore di mettere a terra tali A luglio dello scorso anno avete fatto una rimodulazione del Piano dovuta parzialmente all'aumento dei costi di energia e materie prime. Delle case di comunità, degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali che dovevano essere realizzati con quei 15 miliardi, avete tolto 76 centrali territoriali, 96 ospedali di comunità e 414 case di comunità.

Voi dite che le Regioni non mettono a terra i progetti per i nuovi ospedali, per le ristrutturazioni e via discorrendo. In parte avete ragione, però quelle Regioni in gran parte le amministrate voi e non da ieri, ma da qualche anno, quindi, se avete un problema a usare i soldi,

ma soprattutto l'ha detto la 10a Commissione del Senato, che si occupa di sanità, con un atto approvato all'unanimità da tutti, in cui si riconoscono le difficoltà e la farraginosità dell'utilizzo delle risorse,

lenta, lunga e complicata da utilizzare *(Applausi)*, ossia: come fare per non fare niente. Qualche mese fa c'è stato un incendio in un ospedale a Tivoli.

Che fa la Commissione sanità del Senato, che responsabilmente si occupa del problema? Fa un provvedimento, con l'unanimità di tutti i Gruppi parlamentari, per stabilire che le Regioni dovrebbero fare celermente un piano straordinario di ammodernamento della rete ospedaliera, usando i fondi in maniera snella, magari sul modello del PNRR (se funzionasse, ma abbiamo visto che le realizzazioni sono solo proprio per evitare di incorrere nuovamente in incidenti di questo genere. Si utilizza quindi l'articolo 20 per fare nuovi ospedali (che sono in programma da parte di tutte le Regioni, ma che non riescono a farli), per fare case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali (che non facciamo più col PNRR) e per mettere a posto

le ultime revisioni che ci avete sottoposto e che emergono nella relazione, abbiamo ben pensato di poterci far rientrare anche altri interventi che dovevano essere fatti nell'ambito del PNRR. Mi domando se secondo voi questo articolo 20 sia un pozzo senza fondo e la soluzione a tutti i problemi della sanità italiana. *(Applausi)*. Ci sentiamo dire in continuazione che la sanità non può essere un pozzo senza fondo, quindi abbiamo spostato questa bella frase: la sanità non può essere il pozzo senza fondo della finanza italiana, invece l'articolo l'articolo 20 può essere il pozzo senza fondo dove andare a infilare tutto quello che non riuscite a fare con i soldi che avete già a disposizione. Ci sarebbe da ridere, se non mi venisse da piangere, perché tutto questo non riguarda qualcosa di eccezionale e superfluo, di cui potremmo anche fare a meno, ma riguarda la salute di tutti noi. Infatti, negli ospedali, quando abbiamo difficoltà, ci andiamo tutti, anche noi. noi. Non è la sanità privata quella che poi risolve i problemi reali del Paese. Se avete voglia di spendere utilmente del tempo per farvi un po' di cultura sulla sanità italiana, guardate la puntata di «Presa diretta» che è andata in onda lunedì sera e fatevi venire qualche dubbio su dove stiamo portando il nostro sistema sanitario. *(Applausi)*. Il quadro sarebbe già abbastanza fosco così, se non ci fosse un'altra ciliegina sulla torta, giusto per far capire agli italiani quanto vi interessa la loro salute. Ebbene, tra tutte le misure inserite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in merito alla sanità, c'era un capitolo molto importante, relativo all'ammodernamento tecnologico delle grandi apparecchiature del sistema sanitario nazionale:

anche qui avete fatto bene i compiti a casa e il termine per l'acquisto delle nuove apparecchiature è slittato a giugno 2026. Ma sì, tanto che differenza fa una mammografia fatta adesso o a giugno 2026? Solo la morte. Certo, ma a voi che ve ne importa? Chissà cosa ve ne importa mai della salute dei cittadini italiani, del fatto che con apparecchi mammografici più efficienti si possano fare migliori diagnosi precoci e più mammografie nello stesso tempo rispetto agli apparecchi più vecchi, si possano dare alle donne cure adeguate

Sicuramente i risultati conseguiti hanno riguardato, tra l'altro, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la modernizzazione dell'industria cinematografica e le riforme degli appalti pubblici e del processo civile e penale. Per quanto riguarda la transizione ecologica, l'Italia ha mostrato un impegno notevole verso il raggiungimento di una mobilità sostenibile e la promozione di fonti energetiche rinnovabili, come evidenziato dagli investimenti in idrogeno verde e nell'infrastruttura di ricarica elettrica. Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci chi siamo e non dobbiamo dimenticare che tutto il dimenticare che tutto il settore *automotive* italiano contribuisce all'emissione di CO2 nel mondo solo per lo 0,4 per cento. Qualcuno a Bruxelles ha pensato a una direttiva che dal 2035 mette fuori mercato le auto a benzina e *diesel* e mantiene il solo elettrico. Questa non è sostenibilità ambientale, ma è il suicidio di un intero comparto economico e industriale senza alcuna motivazione ambientale. Questo la Lega lo sostiene e lo ribadisce da sempre ed ecco perché, nel momento in cui vogliamo utilizzare i fondi del PNRR per la transizione ecologica, non dobbiamo non pensare invece a sostenere anche il sistema industriale collegato e favorire solo ed esclusivamente la Cina. decreto-legge cosiddetto PNRR del 2 marzo 2024, attualmente in discussione alla Camera, contiene misure urgenti in diversi settori nevralgici per l'economia nazionale, finalizzate a garantire gli obiettivi del nuovo PNRR italiano. Infatti, a fine 2023 è stato rinegoziato e sono stati ottenuti ulteriori fondi per quanto riguarda il REPowerEU, per altri 2,9 miliardi di euro. Tuttavia, all'articolo 1 del decreto si legge che si interviene al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, abrogando le disposizioni introdotte dal decreto del 6 maggio relativamente al finanziamento di investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria in considerazione del perdurare dei valori limite delle polveri sottili PM10 (materiale particolato) e del biossido di azoto (NO2) in determinati territori del Paese. Nonostante sia condivisibile l'obiettivo del decreto in discussione, si ritiene necessario garantire al Paese, e in particolare ai territori interessati dal superamento del valore limite della qualità dell'aria, le risorse necessarie a garantire gli interventi a breve e lungo termine, intesi a ridurre le concentrazioni in aria dei principali inquinanti atmosferici, *in primis* il PM10 e il biossido di azoto,

per ottenere misure di risanamento atmosferico efficaci ed efficienti per la salute di tutti i cittadini. Questo abbiamo scritto nella risoluzione: chiedo pertanto al ministro Fitto, per suo tramite, Presidente, di tener conto anche delle osservazioni che allora sono state fatte. che allora sono state fatte. C'è poi un altro problema riguardante il Fondo complementare al PNRR, che molti colleghi hanno già evidenziato. Si tratta di una decisione che farà mancare circa 700 milioni di euro già finanziati per la sanità. In particolare, oltre mezzo miliardo viene meno nel programma verso un ospedale sicuro e

Le Regioni lamentano possibili problematiche relative agli investimenti già programmati. Vogliamo e chiediamo quindi, direttamente al ministro Fitto per suo tramite, signor Presidente, la garanzia del rispetto del finanziamento del programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile». La Corte dei conti, invece, critica la frammentazione degli investimenti da parte di numerosi enti attuatori, la presenza di progetti non ammissibili, la scarsa capacità amministrativa dei Comuni e il drastico aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Sicuramente per assicurare il PNRR sarà decisivo rafforzare la capacità amministrativa degli enti. È vero che la revisione del piano di indirizzo sembra quella di ridurre il coinvolgimento dei Comuni, tuttavia, se ciò fosse confermato nel futuro *trend* di sviluppo del Piano, il loro ruolo rimarrebbe comunque centrale nella realizzazione degli obiettivi. È quindi cruciale che si implementino altri interventi per integrare nelle amministrazioni comunali le competenze necessarie a sostenere i processi amministrativi e burocratici richiesti.

Ci arrivano note dai nostri sindaci che stanno costruendo scuole e palestre in cui ci dicono che i Ministeri chiedono documenti su documenti e molto spesso, anche quando vengono loro forniti, non rispondono per settimane e i lavori sono fermi. Non è colpa del Governo, perché questo problema esisteva anche prima. Personalmente, mi occupavo di finanziamenti europei per la ricerca e l'innovazione e non ho mai avuto problemi su progetti con fondi diretti dell'Europa, con procedure semplici, chiare, snelle e pagamenti tempestivi. I fondi indiretti, invece, ricevuti tramite bandi nazionali e regionali, prevedevano sempre tempi lunghi nelle risposte, compilazione di miriadi di documenti, non solo *online*, ma soprattutto cartacei, e continue richieste degli uffici, in fase sia istruttoria sia di rendicontazione. Alla fine tutto questo, se non semplificato, ci si ritorce contro. Come prima non spendevamo i fondi europei indiretti, figuriamoci i fondi del PNRR. Tutte le risorse a tutti i livelli, dal locale al nazionale, devono lavorare tempestivamente e proficuamente alle procedure che sono loro affidate, comprese le varie *task force* che dovrebbero facilitare questo lavoro e non sparire senza fare relazioni o non rispondere agli enti locali realizzatori, specialmente se sono gli enti locali.

insieme alla sua abilità politica, che gli ho sempre riconosciuto e che gli voglio riconoscere anche questa mattina, confeziona sicuramente una narrazione sull'azione del Governo che, se ci fermiamo agli *slogan*, per quello che ci riguarda è ineccepibile. Se ci fermiamo agli *slogan*, però, perché il Ministro giustamente ha detto che ci sono un prima e un dopo, che la revisione è stata necessaria per allineare i dati oggettivi con i cambiamenti

dalla capacità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che come lei ha ricordato è il più importante in Europa. Non a caso, la Commissione europea ci dice che siamo i primi: è il Piano più importante che che abbiamo consolidato e progettato con Next generation EU proprio per rilanciare lo sviluppo economico e la crescita, per ridurre le disuguaglianze e i divari territoriali, mettere in sicurezza e soprattutto per progettare il futuro economico e sociale di questo Paese. Tuttavia, Ministro, lei sa bene che non si genera lavoro

Paese. Quando dico che voglio proporle un salto di qualità nelle relazioni tra Governo e Parlamento, intendo che non possiamo lasciare il Parlamento nelle terze e quarte relazioni. Abbiamo bisogno di un monitoraggio reale dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo spazio per le parole, per le relazioni e per i comizi comincia cioè a ridursi, anche perché i tempi di attuazione di questo Piano sono relativamente brevi. Infatti, chi ha una minima competenza nel rapporto con la pubblica amministrazione sa bene che gran parte del successo di questo Piano dipenderà dalla capacità degli enti locali, dei Comuni e delle stazioni appaltanti di dare attuazione ai progetti, cantierarli e realizzarli.

Credo che ormai il Governo, dopo un anno e mezzo, non possa limitarsi a guardare ad un colpevole, ad una responsabilità al passato, premesso che noi ci sentiamo i protagonisti di Next generation EU e dunque, inevitabilmente, di questo Piano nazionale di ripresa e resilienza.

d'accordo, se è possibile conoscere con quali alleanze l'Italia stia lavorando in Europa per garantire un futuro a Next generation EU, per garantire una stagione nuova di investimenti a debito comune nella dimensione europea.

Ho apprezzato le considerazioni finali che ha fatto nella sua relazione, cioè cominciando ad ipotizzare che, se riusciremo a dare attuazione concreta al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'obiettivo dell'Italia, e dunque anche del nostro Governo, diventerà garantire una misura strutturale agli investimenti nella dimensione europea appoggiata sul rendere e consolidare in maniera definitiva investimenti indispensabili. Diciamoci la verità: l'Europa, per non rimanere un mercato mercato e per continuare ad essere un luogo in cui la produzione industriale e lo sviluppo economico abitano e costruiscono le radici per il futuro, ha bisogno di più investimenti, di nuovi investimenti.

se siamo consapevoli che il successo del PNRR dipende dalla capacità di spesa dei Comuni, cioè se siamo consapevoli di avere 41 miliardi appoggiati al sistema delle autonomie locali,

abbiamo una situazione molto complessa, anche nella dinamica territoriale: ci sono le città metropolitane, i grandi centri urbani, il Nord e il Sud, ma ci sono tante e purtroppo sempre più crescenti aree interne nel Mezzogiorno e nel Nord del Paese.

al dimensionamento delle stazioni appaltanti e alla necessità cioè di avere una nuova riforma della pubblica amministrazione che investa nella parola «pubblica» che - glielo ricordo - non è brutta, ma è l'essenza fondamentale di un'idea di comunità, perché l'attuazione di questo Piano, purtroppo, impatta su divari delle stazioni appaltanti pericolosissimi. C'è un intero Mezzogiorno che, nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rischia di

pensi ad esempio a come garantire più crescita economica in questo Paese. Uno degli obiettivi fondamentali del Governo dovrebbe essere quello delle politiche di genere, perché lei sa

per consentire a questo Paese di recuperare i livelli occupazionali, che ovviamente sono da terzo mondo, non da *leader* in Europa, per quello che riguarda la dimensione femminile, ancora oggi, anche se sono migliorati. Le voglio ricordare che occorrerebbero il salario minimo, i congedi paritari, gli asili nido e i servizi, cioè occorrerebbe un'infrastruttura di questo Paese adatta a quella sfida, che a quel punto garantirebbe più crescita economica, non *una tantum*, ma strutturale. Ho fatto l'esempio degli asili nido perché poi tutto è appoggiato sulla capacità di dare attuazione e concretezza, ma potrei allargarlo ancora alla dimensione sanitaria. Alcune colleghe mi hanno preceduto in questo, lo voglio dire con grande chiarezza: noi avevamo impostato il Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla dimensione sanitaria, perché quella era il pilastro di un'idea di riforma del sistema sanitario. Noi parliamo di tutto in Parlamento, ma non ho visto da parte di questo Governo portare in questa sede un'idea della riforma del sistema sanitario italiano: c'è la medicina territoriale; invece, ho visto purtroppo atterrare sul bilancio dello Stato tagli, non investimenti. Ecco che vedo una contraddizione tra l'aver voluto abbandonare la stagione delle riforme, quelle che servono, e l'aver introdotto nella maggioranza e dunque nell'azione di Governo controriforme che servono probabilmente a rafforzare il vostro consolidamento di equilibri interni, ma che sono dannose all'idea dello sviluppo economico di questo Paese.

Manca. MANCA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, i ritardi su questo pilastro sono elementi che riducono le capacità espansive della crescita economica in questo Paese. Voi avete fatto controriforme, state abbattendo nel sistema giudiziario la certezza della pena e state facendo un'operazione a nostro avviso sbagliata anche sul sistema fiscale, che abbatterà la progressività fiscale, quando invece pagare le tasse è indispensabile per garantire il diritto alla salute e il diritto all'istruzione. Aprite la stagione delle riforme vere e portateci in Parlamento un monitoraggio, perché vogliamo aprire i cantieri per garantire un futuro economico a questo Paese.

la quarta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, approvato in cabina di regia il 22 febbraio scorso, illustra il lavoro svolto dal Governo nel secondo semestre del 2023 per raggiungere tutti gli obiettivi programmati e per completare, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, il processo di revisione del Piano, ottenuto nonostante le forti perplessità di molti esponenti delle opposizioni. L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si concluderà nel primo semestre del 2026, ha rappresentato per il Governo e per questa maggioranza, anche grazie alle modifiche apportate allo stesso ed approvate dall'Europa, una priorità ed una sfida fin dall'avvio della legislatura. Il Governo ha svolto fin dal suo insediamento un'intensa attività di verifica dell'effettiva corrispondenza tra i cronoprogrammi originariamente previsti per gli investimenti e le riforme inserite nel PNRR e i cronoprogrammi aggiornati. Il 2026 è una data rigida per permettere la realizzazione di tutti gli impegni ed è stato serio riconsiderare alcuni progetti non più suscettibili di realizzazione. La rimodulazione è stata necessaria ed i motivi anche geopolitici sono noti a tutti, anche e perché, in mancanza di un tempestivo intervento di tipo correttivo, si sarebbe prodotta l'inevitabile conseguenza di non ottenere da parte dell'Unione europea il trasferimento delle risorse collegate al raggiungimento delle *milestone* e dei *target* del PNRR, con un evidente e grave pregiudizio degli equilibri di bilancio. L'intensa e complessa attività di negoziato con la Commissione europea per la revisione del Piano ha consentito di garantire, da un lato, la destinazione delle risorse e gli interventi più utili per il Paese e, dall'altro, di assicurare la realizzazione dei progetti nei tempi previsti. Quest'attività si è conclusa l'8 dicembre scorso con una decisione del consiglio Ecofin, con la quale la dotazione finanziaria complessiva del Piano è stata incrementata di circa 2,9 miliardi di euro, dei quali sono contributi aggiuntivi a fondo perduto, assegnati all'Italia per l'iniziativa REPowerEU. Il Governo ha saputo dimostrare che il PNRR non è una strada rigida e immutabile, ma piuttosto un percorso che poteva e doveva essere adattato alle reali esigenze e priorità del nostro Paese. È un segno di saggezza e lungimiranza e ciò che è stato realizzato fino ad ora merita il nostro plauso e il nostro sostegno. Anche la Corte dei conti nei giorni scorsi ha sottolineato l'importanza delle modifiche apportate dal Governo alla struttura iniziale del PNRR allo scopo di superare le difficoltà legate alla realizzazione di alcune riforme o investimenti nella loro configurazione originaria. A pochi mesi di distanza possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che quelle promesse sono state mantenute. Il PNRR, signori, non conosce soste: soste: insieme alla relazione, infatti, il Governo ha adottato anche il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, ora all'esame della Camera, con il quale, sul fronte delle misure escluse dai fondi del PNRR, ha stanziato le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti. prevede inoltre la copertura finanziaria relativa anche agli investimenti aggiuntivi previsti dal nuovo PNRR, assicurando altresì la perdurante applicazione agli interventi non più finanziati delle misure acceleratorie e di semplificazione previste per il Piano, ivi comprese quelle relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa e all'utilizzazione delle risorse del fondo per le opere indifferibili già assegnate. Anche il presidente dell'ANCI Decaro, nonostante i problemi che la sua Bari vive in questo momento, ha dovuto dichiarare la sua soddisfazione e riconoscere che tutti i finanziamenti sono stati recuperati e che quindi nessun cantiere, in nessuno degli 8.000 Comuni italiani, dovrà fermarsi, così come da noi già dichiarato in quest'Aula il 1° agosto 2023. Certo, sappiamo bene che non

altri fondi. Chiediamo al Ministro di prestare però la massima attenzione su questi temi e sul lavoro che stanno facendo le Regioni, alcune in particolare, come la mia, la Campania, che è indietro su tutti gli obiettivi della sanità e nella quale abbiamo un Presidente che si preoccupa di fare manifesti e dire che è il Governo che chiude i pronto soccorso, dimenticando che in quel caso la competenza è regionale e quindi è sua. *(Applausi)*. Non dobbiamo però fare polemica, perché siamo nell'Aula del Senato e non su un palcoscenico dove incentivare le *performance* cabarettistiche. Ad oggi, grazie al pieno e tempestivo conseguimento degli obiettivi e traguardi previsti, l'Italia ha ricevuto 102 miliardi di euro sui 194 che costituiscono la dotazione complessiva del Piano. Di questi, 41 sono a fondo perduto. Quello appena trascorso è stato un semestre di intensa attività; strategie ben pianificate e interventi mirati hanno consentito al nostro Paese di ottenere risultati tangibili e, al tempo stesso, straordinari. L'Italia è il primo e unico Stato membro dell'Unione europea ad aver ricevuto, il 28 dicembre, la quarta rata dei finanziamenti. Il Governo, forte dell'attuazione degli obiettivi previsti, il 29 dicembre ha già richiesto l'erogazione della quinta rata. Con l'approvazione della richiesta di pagamento di questa rata, pari ad oltre 10 miliardi, l'Italia avrà conseguito 113 miliardi di euro, pari al 58 per cento dei 194 miliardi stanziati in sede europea per il PNRR. Si tratta di un risultato straordinario e dobbiamo ringraziare il Governo, il signor Ministro e la presidente Meloni, che si stanno impegnando a fondo, rispettando gli impegni europei. L'azione determinata e incisiva del Governo, con il contributo e il solido sostegno del Parlamento, ha consentito di dimostrare, con la forza dei fatti, la capacità del nostro Paese e di questa maggioranza di mantenere gli impegni assunti. Grazie ad una visione chiara e al lavoro di squadra è stato possibile affrontare al meglio le numerose sfide che si sono presentate nell'ambito dell'attuazione del Piano. Non dobbiamo però accontentarci dei successi finora raggiunti. È nostro dovere continuare a lavorare con determinazione, affinché l'Italia prosegua nel cammino di crescita e sviluppo che abbiamo intrapreso. Nella risoluzione che ci accingiamo ad approvare ci sono poi tutta una serie di impegni per il Governo che danno la misura della nostra serietà nel perseguire gli obiettivi che ci siamo posti e nel rispettare anche gli accordi con i *partner* europei. Il Governo Meloni sta realizzando un progetto importante come il PNRR, che vale a costruire anche un metodo di lavoro per noi e per l'Unione europea. In vista delle prossime elezioni europee possiamo dire che l'Italia sta facendo tanto, smentendo tutti i critici e dando una dimostrazione che la serietà e la concretezza pagano e danno risultati a beneficio di tutti. Onorevoli colleghi senatori, nel concludere il mio intervento, desidero sottolineare nuovamente l'importanza fondamentale del Piano, così com'è stato modificato, come strumento per investire nel futuro e nella crescita del nostro Paese. L'instancabile impegno del nostro Governo ha reso possibile il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati, con progetti in corso che promettono di trasformare e rinvigorire l'economia e la società italiana. Tuttavia, non possiamo ignorare le sfide che ci attendono e la responsabilità, in capo ad ognuno di noi, di fare il massimo per il bene della nostra Nazione. In questo contesto, ritengo essenziale sottolineare l'importanza dell'unità nazionale di fronte ad un piano di investimenti di tale portata. È inaccettabile che le opposizioni, per dare legittimazione alle loro campagne denigratorie contro il Governo, tifino addirittura contro gli interessi nazionali, sperando che l'Italia fallisca gli obiettivi previsti e perda i finanziamenti e le risorse previsti dal Piano. È sconcertante che per alcuni sembri più importante che il Governo commetta errori piuttosto che l'Italia apra le porte al suo futuro. confido nelle nostre capacità e nella capacità del Parlamento italiano di superare tali divisioni e di unirci nell'interesse superiore del Paese. Solo lavorando insieme, Governo, opposizione e società civile, possiamo garantire il successo del PNRR e il rilancio dell'Italia verso un futuro prospero e sostenibile. L'approccio basato sul dialogo, a livello sia comunitario sia interno, è molto apprezzato ed ha già dato i suoi frutti. Per me vi sono temi che trascendono i colori politici. L'interesse nazionale ed il benessere dei cittadini dovrebbero sempre prevalere sulle faziosità di parte. Desidero esprimere la mia fiducia nella *leadership* della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale, con la sua guida determinata e visionaria, saprà condurre l'Italia verso un nuovo orizzonte di libertà e di crescita. In conclusione, signor Presidente, richiamare una citazione di Abraham Lincoln, che incarna perfettamente lo spirito che il nostro Governo sta dimostrando: «Il **miglior modo** di **prevedere il futuro è crearlo»**. È quello che stiamo facendo: stiamo dimostrando, con azioni concrete, come tradurre la nostra visione di Italia in realtà. Con unità, dedizione e fiducia nel futuro, possiamo costruire finalmente un'Italia migliore per tutti, creando oggi il futuro di domani.

I testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

Lo voglio dire partendo dal primo intervento, quello della senatrice Rojc: utilizzare le parole "fallimento" e "propaganda" sinceramente lo trovo un po' eccessivo, me lo consenta; possiamo anche non essere d'accordo, ma parlare del lavoro fatto come di un fallimento obiettivamente mi sembra assolutamente sopra le righe sotto tutti i punti di vista.

ascoltato con molta attenzione e glielo dico perché il decreto è in Aula alla Camera e in Commissione si sta discutendo. Dico queste cose perché penso che non faccia bene al nostro dibattito avere un approccio di questo tipo. più utile magari anche inserire elementi di contrapposizione e di divisione, ma oggettivamente su alcune questioni penso che ci sia bisogno di avere un approccio anche

alcuni dei quali voglio tornare per approfondire. Il tema che in più interventi è tornato, quello della Corte dei conti, dobbiamo leggerlo per quello che è: la Corte dei conti - lo ribadisco perché evidentemente non sono stato chiaro nel mio primo intervento compreso - nella sua prima relazione, che si riferiva al primo semestre del 2023, quindi fino a giugno 2023, ha indicato con i dati del febbraio 2023 un giudizio con una serie di criticità che risentivano della valutazione a quella data. La relazione che la Corte dei conti ha presentato alcuni giorni fa, che si riferisce all'intero 2023, rappresenta un quadro completamente differente. Perché non dirlo? Perché dire che la Corte dei conti ha espresso un giudizio negativo? A cosa serve? Sono dati oggettivi. La Corte dei conti ha espresso valutazioni di preoccupazione sull'andamento della spesa - è un tema sul quale ho parlato e farò ancora ulteriori

ha previsto una rimodulazione con lo spostamento fuori dal Piano di alcuni interventi, che non sono stati rimandati indietro. L'articolo 1 del decreto-legge n. 19, che è in discussione in queste ore (e domani pomeriggio ore (e domani pomeriggio sarò presente in Commissione bilancio per illustrare la posizione del Governo), prevede l'intero finanziamento di questi progetti. Non si può parlare quindi di progetti mandati indietro:

Abbiamo trovato all'interno del Piano una serie di progetti che vi erano stati inseriti. Prima ho fatto un esempio che voglio ribadire ancora di più: i sei miliardi di euro per piccole e medie opere sono di un programma del 2019 che è stato inserito all'interno del Piano, senza tener conto delle condizioni Se noi non avessimo fatto questa operazione, avremmo inseguito il taglio delle rate di volta in volta. *(Applausi)*. Avremmo mancato gli obiettivi, perché i progetti ai quali facciamo riferimento - e questo non l'abbiamo deciso noi, ma l'abbiamo condiviso con la Commissione europea - non erano rendicontabili, non erano ammissibili il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo voglio sottolineare perché è importante che su questi aspetti ci si intenda. Occorre intendersi sul fatto che questi interventi sono stati rifinanziati - quindi non mandati indietro - al punto che - lo ribadisco ed è stato detto anche durante il dibattito - il presidente Decaro, in una dichiarazione, ha espresso l'apprezzamento dell'ANCI perché è stata mantenuta fede all'impegno che il Governo aveva assunto di rifinanziare tutti i progetti. *(Applausi)*. Non c'è quindi alcun definanziamento. Lo dico perché di questo tema si è parlato per mesi. Si è raccontato che noi avevamo fatto dei tagli. Nessun taglio: abbiamo riprogrammato e garantito gli interventi. Lo dico anche in riferimento a un altro tema, che è stato oggetto di diversi interventi. Penso alla questione collegata alla sanità,

In riferimento alle questioni oggetto di critica, vorrei ricordare che ci sono dati che spesso non vengono considerati.

diversi miliardi di euro non ancora impegnati. Per questa ragione, all'interno del decreto-legge n. 19 del 2024 troverete una norma specifica che individua lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo per avviare una velocizzazione nella spesa delle risorse assegnate per gli investimenti nel campo sanitario. Sono queste le considerazioni oggettive rispetto al lavoro che si sta facendo. Penso che non sia utile che questi temi diventino oggetto di polemica. Ascolto ogni volta - e lo rispetto, ma mi consentirete di non condividerlo il richiamo al risultato raggiunto, in termini di merito, sull'importo del Piano. Vorrei ricordare che il Next generation EU e il conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza sono oggetto di finanziamenti collegati a tre fattori, non al merito. Con esso, si dava una risposta alla crisi del Covid-19 e l'Italia ha avuto quell'importo perché è uno dei Paesi con la popolazione più ampia, popolazione più ampia, che nella fase Covid-19 ha avuto la peggiore *performance* in termini di crescita del prodotto interno lordo e ha avuto una delle peggiori *performance* in assoluto sul fronte dell'occupazione. Queste sono le ragioni che hanno determinato quell'importo. All'interno di quel Piano, però, i 68 miliardi di euro a fondo perduto,

debito. La dimensione del Piano è quindi determinata da una scelta che altri Paesi (quasi tutti) non hanno fatto, come ho ricordato. Non è una polemica: è un rimettere in ordine i vari passaggi e dire le cose come stanno. stanno. Non è un caso che, per esempio, la Spagna - cito un Paese con un Governo certamente non in linea con il nostro, di colore politico completamente differente e alternativo - abbia scelto di utilizzare la quota a debito collegata al piano di investimenti sul REPowerEU, cosa che non aveva fatto prima. È evidente che la valutazione sulla possibilità o meno di andare a indebitarsi sia stata fatta nel momento in cui è sorta un'esigenza alla quale dare una risposta strutturale sul fronte degli investimenti. È per questo che noi, non avendo

grattacapi e problemi e coprendo con quelle risorse interventi che non avevamo nel Piano e che altri Paesi stanno utilizzando. Il tema delle risorse assegnate alle imprese - penso alla transizione energetica - è fondamentale, perché consente

importante esprimere qualche altra valutazione su alcune considerazioni. La collega Murelli ha posto il tema delle risorse per la qualità dell'aria, che è collegato non alla relazione, ma al decreto-legge all'interno del quale si è compiuta un'operazione

le finalità della legge. Condividendo pienamente la valutazione che è stata fatta, è impegno del Governo recuperare quell'importo e quelle risorse, come ho avuto già modo di dire in via informale e come emergerà nell'ambito della discussione che faremo sia sul decreto-legge PNRR, sia sul successivo decreto-legge collegato al procedimento

nei decreti-legge che stiamo discutendo troveremo certamente la garanzia rispetto a questo tema. Mi piace sottolineare anche il tema della capacità amministrativa, che è stata più volte sollevata nei vari interventi. Il riferimento è a un'iniziativa che il Governo ha assunto e che era all'interno del decreto Sud e coesione varato lo scorso anno. Al suo interno, oltre a una serie di scelte che sono state citate - penso al tema della zona economica speciale, così come al meccanismo dei nuovi accordi di coesione che sono in linea con l'approccio e con la *governance* della spesa rispetto alla responsabilizzazione dei diversi livelli istituzionali - abbiamo individuato, con il Programma coesione 2021-2027 (*CapCoe*), una prima importante risposta per una parte del Paese, se è vero, com'è vero, che con l'utilizzo di risorse europee, cogliendo questa opportunità, finanziamo un programma di assunzione di 2.200 persone all'interno della pubblica amministrazione, l'85

le scelte sul fronte delle aree interne. E, sempre per la prima volta, un Governo si sta ponendo il problema di dare risposta a una delle questioni fondamentali per il futuro del nostro Paese, se è vero, come lo è, che se da una parte c'è una strategia sulle grandi aree metropolitane e sulle città metropolitane, dall'altra c'è l'esigenza, dal punto di vista non solamente demografico, ma anche della garanzia dei servizi,

delle polemiche rispetto alle scelte che stiamo facendo in termini di rimodulazione. Su questo vorrei fare una considerazione di carattere più generale, cui ho accennato poc'anzi, che cambia completamente l'approccio. Qui non si può dire: c'è questo intervento, lo state togliendo. Bisogna capire perché un intervento è stato inserito all'interno del PNRR e se rispetta i *target* e le *milestone* per i quali è stato inserito. inserito. Se non dovesse succedere questo e non dovessimo fare quello che abbiamo già fatto e che continueremo a fare, vi daremo la possibilità, in quest'Aula, di dire: avete perso la rata, vi stanno tagliando le risorse, non state raggiungendo gli obiettivi. *(Applausi)*. un interesse comune evitare tutto questo e dovrebbe essere una delle principali strategie lavorare insieme perché ci possano essere obiettivi da raggiungere che siano coerenti e in linea con quanto previsto all'interno del Piano. Questo riguarda tutte le questioni che sono state indicate all'interno del dibattito. Voglio dirlo anche rispetto ad alcune considerazioni sul fatto che si proceda per *slogan* o con dichiarazioni generiche da comizio. No, mi dispiace: l'azione del Governo su questo è sempre stata e continua ad essere molto puntuale e, anche nell'ambito di questa replica, mi fa piacere confermare

tra il prima e il dopo, che è stata più volte evocata. Se avessimo voluto fare una polemica tra il prima e il dopo, avremmo avuto tanti argomenti per incendiare il dibattito parlamentare, ma non ce n'è bisogno, non serve a nessuno. Serve un approccio corretto e coerente rispetto al fatto che dev'esserci una continuità istituzionale, ma ci dev'essere anche una valutazione attenta dei progetti e delle iniziative che devono essere messe in campo. E soprattutto c'è bisogno di un lavoro che all'interno di questo Parlamento trovi, anche nel riscontro del pregresso, lo stesso approccio. Penso sia utile allargare il ruolo del Parlamento, trovare delle formule. Non so se i tempi ce lo consentiranno, ma in alcune proposte di risoluzione si parla della necessità di dare un maggior ruolo al Parlamento sul fronte della rendicontazione dei progetti. Io penso che i progetti non possano essere oggetto di questa valutazione, perché sono oltre 254.000. Vogliamo pensare di poterlo fare? Penso di no.

Lo dico perché è evidente che in questo contesto, se la richiesta è creare le condizioni per avere un momento di confronto ulteriore con il Parlamento che vada anche oltre le previsioni normative,

spesso detto, anche con forme di critica, noi siamo nelle condizioni di poter dire con chiarezza che, rispetto alle questioni sollevate, ogni volta che c'è stata l'esigenza di un confronto con il Parlamento, lo abbiamo garantito

Sospendo la seduta per dieci minuti,

parere è favorevole sul punto 5 del dispositivo con la seguente riformulazione: «ad assumere ogni iniziativa necessaria per assicurare la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e in particolare di quelle ad alta velocità nei territori delle Regioni Calabria e Sicilia». 7 del dispositivo si propone la seguente riformulazione: «ad assumere ogni iniziativa necessaria ad assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del dissesto idrogeologico con particolare riguardo ai territori caratterizzati da maggior rischio».

«a garantire, nel rispetto della pertinente normativa, la tempestiva trasmissione al Parlamento di tutte le informazioni occorrenti per valutare lo stato di avanzamento del PNRR a livello di ciascuna misura e submisura, nonché ad assicurare la presenza dei Ministri, qualora chiamati in audizione in Parlamento, per fornire informazioni dettagliate e i chiarimenti necessari sull'attuazione del PNRR relativamente alle riforme e agli investimenti

Signor Presidente, voglio cogliere l'occasione di confronto tra il Governo e il Parlamento che il ministro Fitto ci dà oggi con le comunicazioni sul PNRR. Signor Ministro, ha detto che questa può essere un'occasione per fare una verifica sugli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere nelle rate successive. Voglio prendere questo impegno metodologico proprio per fare ciò che Azione fa sempre, ossia entrare nel merito delle questioni. Lei ha ricordato alcuni passaggi importanti della negoziazione con la Commissione europea. Per esempio, è partito dalla rimodulazione della quarta rata per introdurre un precedente per la rimodulazione complessiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ha citato alcuni eventi, quali la guerra in Ucraina, la crisi energetica e l'aumento dei prezzi, per ricordarci che il programma REPowerEU, di fatto, ci aiuta a sterilizzare l'aumento dei prezzi e dà un'accelerazione per favorire l'indipendenza energetica. Signor Ministro, voglio dirle con molta franchezza e molta sincerità che in questi mesi si è dimostrato un eccellente negoziatore con la Commissione europea. Cosa non ci convince della riformulazione o della revisione del Piano? Il fatto che lei proceda con una gestione commissariale: in che senso, «commissariale» verso chi? Verso chi ha avuto scarsa capacità di spesa. Nella comunicazione ha citato i tanti progetti, ad esempio sotto i 100.000 euro, quindi le difficoltà della pubblica amministrazione. Sarebbe forse opportuno ricordare che la scarsa capacità di spesa, con risultati ben sotto la media, ha riguardato non solo i Comuni piccoli, ma in primo luogo i Ministeri. Il Ministero del lavoro ha speso lo 0,6 per cento dei fondi; il Ministero del turismo il 2,8 per cento; il Ministero dell'agricoltura il 3 e il Ministero della salute il 4

vi sia una gestione commissariale delle spese del PNRR. Azione è e sarà sempre a favore del PNRR. Lo saremo anche questa volta, perché chi scommette contro il PNRR non scommette sul fallimento del Governo, ma scommette sul fallimento dell'Italia e dell'Europa e noi non scommetteremo mai sul fallimento dell'Italia e dell'Europa. Quella che vogliamo offrire è una chiave di lettura diversa per valutare il successo o l'insuccesso del Governo sul PNRR. Se lo valutiamo dal punto di vista delle negoziazioni delle rate, dobbiamo ammettere che il Governo, sia nella quarta rata sia nella gestione della quinta rata, sta procedendo bene, in modo positivo. Questa può essere però l'unica chiave di lettura per analizzare il successo del Governo nella gestione del PNRR? A nostro avviso, no. Ve ne sono almeno altre due. La prima è la capacità di spesa.

Rispetto alla stima iniziale di 86 miliardi di euro entro la fine del 2023 è stato speso poco più della metà dei fondi disponibili. Se questo è il tema, non possiamo ritenerci soddisfatti. Sapevamo però che le difficoltà del nostro Paese non riguardano né questo Governo né il prossimo, ma il sistema Paese in quanto tale.

pubblica amministrazione, giustizia, sanità, istruzione. *(Applausi)*. Nella sua comunicazione, oltre alla contabilità sui progetti e sulle rate, ci aspettavamo da lei un intervento su alcuni aspetti essenziali. Uno: quali riforme trasversali sono state realizzate e quali non sono state ancora realizzate? Due: quali spese hanno avuto un effetto moltiplicatore sugli investimenti? Le ricordo - lo sa benissimo - che il PNRR non è fatto per la spesa corrente, ma dev'essere un volano degli investimenti. In

Il primo: abbiamo bisogno di un vigoroso piano di stimoli sugli investimenti. Lo ripeteva ieri il presidente di Confindustria noi di Azione lo stiamo dicendo da inizio legislatura: ripristinate integralmente le misure di Industria 4.0 ed estendetele

per pagare adeguatamente medici e infermieri significa che le strutture della medicina territoriale e le case della salute rischieranno di diventare scatole vuote, se non ci mettiamo dentro infermieri e medici.

- per questo si chiama Next generation EU - a poter beneficiare delle riforme che devono essere fatte verso la transizione ecologica e verso la transizione digitale. *(Applausi)*. Noi ci asterremo, ma se

nuova finestra"). Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Aldo Moro» di Montesarchio, in provincia di Benevento, che assistono ai nostri lavori.

il ministro Raffaele Fitto che, da quando si è insediato l'Esecutivo, ha lavorato con grande impegno e determinazione nell'interesse esclusivo del Paese. Lo dico perché tante volte, purtroppo, abbiamo assistito a un triste copione delle opposizioni: sperare che l'Italia non faccia una bella figura in Europa, cosa che non è avvenuta. Ciò vuol dire non volere il bene dell'Italia e soprattutto degli italiani, che viene prima di qualsiasi cosa. Ce lo ricorda La proiezione sulla crescita del PIL nel 2026, quando il PNRR sarà completato, sarà dell'1,4 per cento in media europea. Per Paesi come l'Italia, questo tasso di crescita della nostra economia, secondo queste proiezioni, salirà del del 2-2,5 per cento, quindi la potenzialità dello strumento è fondamentale, ma soprattutto grazie a questo Governo e a lei, Ministro, siamo il primo Paese in Europa per obiettivi realizzati nell'ambito del PNRR. Non siamo stati noi a promuoverci, ci mancherebbe. Siamo i più virtuosi, con 178 obiettivi raggiunti sui 527 originari. Lo ha certificato la Commissione europea, che ha pubblicato qualche settimana fa la valutazione di medio termine dei piani. L'Italia è prima in Europa. Il Piano va avanti. Certamente ci sono ancora tante tappe da compiere. Siamo consapevoli che si tratta di un percorso lungo e complesso, ma di certo siamo sulla strada giusta. Anche la Corte dei conti, come diceva signor Ministro, alcuni giorni fa ha espresso, fra l'altro, un giudizio totalmente positivo sullo stato di attuazione del PNRR nel 2023. È un altro segnale positivo e incoraggiante, così come positive e incoraggianti sono state le valutazioni della Corte sulle modifiche apportate al Piano. Da più parti si diceva che, se avessimo tentato di rinegoziarlo, avremmo rischiato di perdere le risorse. Noi abbiamo sempre ritenuto che dovesse essere rinegoziato, quando è stato scritto la realtà era diversa: non c'era la guerra in Ucraina, non c'era il conflitto in Medio Oriente, non c'era stata una crisi energetica significativa, che ha portato al capitolo importante del REPowerEU e al piano Transizione Transizione 5.0, su cui giustamente c'è grande attenzione da parte delle imprese e del mondo produttivo. Sono risorse centrali per favorire la doppia transizione digitale ed ecologica. Abbiamo il dovere di non deludere le attese di chi, come le nostre aziende, rappresenta il motore socioeconomico dei territori. n. 19 sul PNRR, recentemente emanato dal Governo, ha cominciato il suo *iter* alla Camera di deputati, nella Commissione bilancio. Il decreto-legge, come diceva proprio lei, Ministro, consente lo sblocco di 6,3 miliardi di euro di crediti d'imposta per la transizione *green* e digitale delle imprese. è importante, a nostro avviso, che sia stata aumentata la dotazione finanziaria nell'ambito del settore agricolo, con interventi pari a circa 3 miliardi L'agricoltura è vita ed è essenziale investire su questo settore, che non a caso viene chiamato primario, perché primaria è la sua funzione per la vita di tutti noi. Lo abbiamo fatto, come ha ricordato lei, a dicembre e non a seguito delle proteste dei trattori che abbiamo visto nei giorni scorsi. Riteniamo essenziale garantire una spesa efficiente dei fondi europei e nazionali, per dare corso a tutta una serie di interventi indispensabili per la sicurezza idrogeologica dei nostri territori, a partire dalla realizzazione dei bacini di laminazione. Le risorse sono strumenti che devono essere adeguati al mutare del contesto. La revisione del PNRR, come ha evidenziato anche il presidente Meloni, è stata la cosa giusta da fare. Occorre quindi continuare a lavorare affinché si raggiungano i *target* previsti nel 2024 per ottenere la sesta e la settima rata del PNRR. L'Italia ha il PNRR più grande; abbiamo ricevuto lo stanziamento maggiore, pari a 194,4 miliardi di euro (e, a seguito della revisione, gli importi sono stati addirittura incrementati), di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni. Nel 2023, grazie al buon governo del centrodestra, abbiamo presentato gli obiettivi e ottenuto il pagamento della terza e quarta rata. Le somme erogate ammontano a 101,9 miliardi 101,9 miliardi di euro. Non solo: siamo stati la prima Nazione europea a presentare gli obiettivi per la quinta rata e abbiamo rinegoziato gli obiettivi del PNRR, cosa che si poteva e si doveva fare. Insomma, tutto tutto questo ci dice una cosa, cari colleghi: la maggioranza che c'è in Parlamento ha nel suo DNA politico la cultura del fare. Oggi, in quest'Aula, chiediamo al Governo di proseguire sulla buona strada, per mettere a terra le risorse europee, proseguendo le interlocuzioni con la Commissione e soprattutto coinvolgendo le Regioni e gli enti locali. Gli enti territoriali svolgono una funzione essenziale per vincere la sfida del PNRR e, in questa fase delicata, hanno bisogno di tutta la nostra attenzione. Già, perché il successo e la buona riuscita del *recovery plan* dipendono dal dialogo tra centro e periferia e dalla sinergia fra tutte le istituzioni, a tutti i livelli. Ecco perché

Partiamo dalla semplice veste grafica della relazione di accompagnamento, che è corposa, di 700 pagine. Gli Uffici l'hanno fatta girare e non l'hanno neanche stampata in copie per tutti quanti i senatori (giustamente, perché avrebbe rappresentato uno spreco enorme di carta).

in parte perché venivano da altre programmazioni e progettazioni che secondo lei non erano coerenti con le linee del PNRR, in parte perché erano interventi sotto i 100.000 euro e lei ha considerato una frammentazione della spesa che avrebbe rallentato la rendicontazione, in parte per altri motivi, perché non pensava che potessero raggiungere e rispettare le *milestone.* Più o meno queste sono state le motivazioni che nel tempo le abbiamo sentito dire.

In questi otto mesi, però, gli enti locali e i sindaci, che erano gli unici che avevano realmente rispettato le scadenze, avevano pubblicato le gare e avevano anche aggiudicato i lavori, sono rimasti bloccati con le imprese che hanno cominciato a sollecitare le consegne delle opere per avviare i lavori e con le Ragionerie degli enti locali che hanno cominciato a temere che si creasse un debito fuori bilancio. Questo perché? Lei viene

è considerato come un'entità. Che cos'è? È il PNRR, ma noi sappiamo bene che il Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'insieme di una serie di progetti, azioni e obiettivi che devono servire a riprendere, rilanciare e sviluppare l'economia nazionale e fare questa famosa transizione energetica. Pertanto, la mancanza di concretezza e dettaglio delle sue relazioni purtroppo ci ostacola o comunque rende difficile poter esprimere un apprezzamento compiuto sulla sua attività.

tutte le risorse che potevano essere utilizzate per lo sviluppo e la coesione e per le infrastrutture territoriali finiranno per essere portate sulle opere che dovevano essere finanziate con il PNRR.

l'approvazione e il pagamento delle rate. Benissimo, questo lo accredita sicuramente come un abile negoziatore, ma non lo accredita altrettanto bene come un abile amministratore. Mi dispiace, ma questo lo dobbiamo dire chiaramente. *(Applausi)*. Lo dico perché, ottomesi per capire che poi questi progetti di rigenerazione urbana andavano finanziati con i fondi nazionali sono troppi, lo si poteva dire anche prima e ci si sarebbe arrivati lo stesso. Inoltre, nella nuova rimodulazione del PNRR che il Ministro presenta

possibilità di avere servizi e si colpisce sempre la sanità pubblica, perché mi dispiace, ma la verità è che quella che viene sempre sistematicamente colpita è la sanità pubblica.

ma poi non sappiamo esattamente quali sono o comunque leggendo la relazione apprendiamo che la maggior parte sono obiettivi amministrativi, di digitalizzazione, di servizi,

sono stati stralciati quattro miliardi di euro per il finanziamento del terzo valico ferroviario. Dove sono queste somme? Quando si faranno queste opere? Possiamo temere di restare senza il terzo valico? Poi che cosa faremo?

ma poi alla fine bisogna ottenere un risultato concreto, che sono le infrastrutture. Facendo un rapporto costi-benefici, avremo anche avuto tante risorse, ma evidentemente non le sappiamo ancora spendere e continuiamo a non spenderle adeguatamente e gli unici che avevano dimostrato di saperle spendere, che erano i sindaci, per otto mesi li abbiamo fatti stare fermi e adesso gli abbiamo detto che devono usare le risorse che avrebbero dovuto utilizzare per altre attività. Il PNRR è sicuramente innovativo, non soltanto per le sue finalità, ma anche per la sua impostazione, è un piano cosiddetto per *performance* e per *performance* il Ministro ha voluto trasformare anche il Fondo per lo sviluppo e la coesione, perché quando lo ha modificato con il decreto cosiddetto Sud ha voluto trasformare anche questo fondo in un piano per *performance.*

Questa impostazione, ovviamente, intrinsecamente è anche corretta, ma diventa sbagliata quando poi non si danno le capacità alle amministrazioni di raggiungere gli obiettivi quando poi non si fa veramente una riforma della pubblica amministrazione e quando ci si limita a dare le risorse per fare assunzioni a tempo determinato e poi trasformarle a tempo indeterminato. In questo modo, certamente la spesa non si libererà e non riusciremo a raggiungere gli obiettivi. Questo - si badi bene - non lo diciamo con compiacimento, al contrario lo diciamo con grande preoccupazione, perché non torneranno più risorse così ingenti da parte dell'Europa per l'Italia e il nostro dovere è vigilare, stare attenti, suggerire,

vanno raggiunti, ma senza lasciare indietro nessuno, non con rinegoziazioni a discapito delle attività e delle realtà territoriali, ma a vantaggio delle stesse, mettendo le risorse anche per far raggiungere i risultati attesi.

quindi ogni anno dobbiamo raddoppiare la spesa rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Come pensiamo di poter velocizzare la realizzazione dei progetti, se continuiamo a non voler investire sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione? Chi farà questo lavoro? Vi sono poi settori in cui siamo davvero solo all'inizio. Dalla relazione emerge che gli investimenti diretti in opere pubbliche sono fermi all'11

idrogeologico: in sostanza si confermano scelte politiche regressive del Governo nei confronti del Mezzogiorno, che contribuiranno ad ampliare i divari

sanitario universale, tanto che nel piano di revisione del PNRR il Governo ha operato un taglio di 510 strutture tra ospedali e case di comunità. Tuttora il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi territoriali,

non possono essere immobili vuoti, ma bisogna fare in modo che ci siano persone che operano e siano in grado di intervenire, quindi siamo di fronte a una situazione del tutto inadeguata quanto al modo in cui affrontare questo tema. Per non parlare poi

Anche in materia di mobilità sostenibile, il PNRR di fatto è inadeguato: ad esempio, si prevede l'acquisto di 3.400 autobus elettrici, a fronte di un fabbisogno che è più del doppio; sono eliminati i finanziamenti all'Alta velocità nel Mezzogiorno. Si parla del ponte di Messina, però non si fanno i collegamenti all'interno del Mezzogiorno, in cui si tagliano addirittura 787 787 milioni di finanziamento. Il Governo fa un gioco del tutto opaco, tra definanziamento e finanziamento, che sostanzialmente coinvolge senza coinvolgere le parti sociali e gli enti locali, tant'è che le Regioni in questi giorni stanno predisponendo un documento unitario che lamenta la sottrazione di 700 milioni di finanziamento alla sanità. Tutto questo mentre si azzerano le risorse del Fondo di perequazione infrastrutturale, che costituisce la premessa di un riequilibrio del Paese, anche dal punto di vista geografico. Il Mezzogiorno continua a pagare un prezzo più alto in termini di desertificazione industriale, produttiva, sociale e demografica. Concludo con un cenno alla questione che per me è più rilevante, quella che, al di là dei ritardi, è davvero gravissima: la totale assenza di una visione di prospettiva e di programmazione del futuro. Questo è il dato fondamentale: è del tutto assente un'idea di politica industriale. Il PNRR dovrebbe essere una grande occasione per realizzare una riconversione ecologica dei settori produttivi del nostro Paese, ma in esso manca l'impegno di risorse significative in nuove tecnologie, nella ricerca di soluzioni innovative, nei processi produttivi e nei nuovi prodotti da immettere sui mercati nazionali e internazionali. È sbagliato e miope affrontare il Piano separando la questione della transizione ecologica da quella industriale, perché dovrebbe essere esattamente il contrario:

Una parte importante del nostro sistema produttivo, prima o poi, si troverà di fronte a un bivio: delocalizzare nelle aree del mondo a basso costo, seguendo il vecchio modello dell'economia fossile, oppure cambiare facendo leva, con il tempo necessario, sugli investimenti necessari che far decollare la transizione ecologica. Ecco, questo Governo - lo conferma la sua relazione, Ministro - nega la crisi climatica, taglia le risorse al PNRR sulla transizione ecologica, spinge per il rafforzamento degli investimenti e le infrastrutture legate a fonti fossili e rallenta tutto sul versante delle rinnovabili,

che vorremmo ospedali fantastici e avere infrastrutture realizzate, salvo il fatto che poi quelli che le auspicano sono coloro che fanno i comitati per dire «no» pure a un'antenna del telefono, non dico a qualche opera pubblica più importante. Veniamo ai dati che fanno da sfondo a questa fase, in cui il ministro Fitto, accogliendo giustamente l'ennesimo invito del Parlamento, ha annunciato una sua presenza continuativa su una vicenda che accompagnerà per molti anni l'Italia e l'Europa. Lo *spread* è sceso a 130 punti di base, una cifra tra le più basse degli ultimi anni, pari a meno della metà

Abbiamo oggi 700 miliardi di titoli pubblici di Stato in mani italiane; ciò vuol dire avere anche una capacità di controllo all'interno dei nostri confini di una parte importante del debito. È migliorato il clima di fiducia dei consumatori, gli occupati sono aumentati di 362.000 unità in un anno rispetto

Prima si faceva assistenzialismo e non sviluppo; e ancora, l'inflazione ha avuto un regresso importante; il PIL ha comunque un segno positivo: vorremmo tutti di più, ma altri Paesi europei, anche quelli tra i più importanti,

nel corso dello scorso anno, abbiamo avuto 24 miliardi di recupero di evasione fiscale. Eppure siamo un Governo di centrodestra che non vuole essere un governo di tagliagole fiscali; vogliamo che si paghi il giusto, vogliamo che, per esempio, paghino i giganti della rete. Leggevo poco fa il pessimismo di Giorgetti rispetto

per proseguire interventi che non erano più finanziati dal PNRR. Ci sono problemi di misure che non potevano essere finanziate perché non c'erano i progetti. È stato spiegato decine di volte. Non si può lasciare un appostamento di cifra, se non c'è il progetto. Si sospende quel finanziamento, si accantonano delle cifre, si trovano altri fondi, si fa un'azione combinata tra fondi di coesione e altre voci per massimizzare gli effetti. È inutile lasciare una cifra, se non c'è il progetto fatto casomai da un sindaco o da un presidente di Regione che fa il corteo a Roma, invece di stare a casa sua a spendere le cifre adeguate. Dirò poi qualcosa su quel presidente di Regione. Voglio anche ringraziare i ministri Zangrillo e Bernini, ma anche tutti gli altri Ministri, compresi quelli di Forza Italia, che nei loro capitoli di competenza danno un contributo efficace e serio. Riteniamo che ci siano anche riforme che vengono sollecitate attraverso il PNRR, che riguardano l'ordinamento, il territorio e le infrastrutture. Quelli che fanno una descrizione fantasiosa di un fallimento dicono bugie, ma il Paese se ne accorge. Se ne accorge in Abruzzo e se ne sono accorti pure in Sardegna, dove i voti delle nostre liste

mi mette di buon umore leggere fantasia. Penso che sia importante quello che è stato fatto anche l'8 dicembre presso l'Ecofin, dove l'Italia ha ottenuto altri 2,9 miliardi, arrivando a 194,4 miliardi di euro, anche con REPowerEU. Abbiamo avuto poi la criticità della mancanza di progetti sul territorio talvolta, ma il Governo sta affrontando anche questo aspetto. Tutto questo viene fatto alla luce del sole, con informazione e L'Italia ha portato sostanzialmente a casa 102 miliardi sui 194 previsti, ma forse la mia stima non è nemmeno adeguata, perché, mentre si discute, le famose rate arrivano e vengono erogate. Si va a Bruxelles e si dimostra la correttezza dell'operato. Il nostro ruolino di marcia è quindi rispetto. Bisogna evitare sprechi e sperperi, non finanziare misure che non si fanno, finanziare quelle che si fanno e stimolare tutti a fare e ad agire. Non voglio qui ricordare i meriti storici del presidente Berlusconi e di Forza Italia rispetto a questo progetto, che nasce dal disastro del Covid-19 e dall'emergenza, ricordare gli errori dei Governi guidati da Conte, che erano stati rimandati con perdite, perché mandavano carte, ma non progetti seri. Devo riconoscere che anche il Governo tecnico segnò un miglioramento, ma questo attuale Governo politico di centrodestra ha migliorato molto le cose e le carte, anche rispetto al al Governo tecnico e a Draghi (sicuramente persona migliore di Conte, ma non è che ci volesse molto per essere migliore di Conte). Credo pertanto che tutti questi indicatori economici che ho citato si colleghino a tutto ciò. I piani andranno oltre il 2026

(dove De Luca imita Crozza, che imita De Luca, che imita quell'altro e non si capisce più; a volte, l'imitazione di Crozza che imita De Luca è migliore del De Luca originario o anche di Crozza senza la parrucca; insomma, non si capisce più dove siamo).

però, non ci sono progetti, mentre il Governo sta girando l'Italia per firmare accordi con le Regioni. Il ministro Fitto accompagna, per le sue competenze, il presidente del Consiglio Meloni dal Nord al sud, da Presidenti di Regioni che la pensano in un modo o in un altro. Non ci sono distinzioni, ma accordi che vengono firmati.

sono voluti il Governo Meloni, il centrodestra e i nostri Ministri, che ci vanno sempre. Lui si offende, ma voi andate a fare fatti. Lui ha lasciato il degrado in quelle zone. *(Applausi)*. Questo è il bilancio, quindi, prima di fare lezioni o di andarvene offesi,

forse anche i tecnici devono imparare un po' da una politica che ha saputo negoziare - e nemmeno ci ispireremo al disastro della Regione Campania. Il nostro voto quindi, attraverso la risoluzione che ho sottoscritto a nome del Gruppo Forza Italia, è convinto, di apprezzamento all'azione del ministro Fitto e di tutto il Governo, che saprà affermarsi in Europa nel difendere anche l'economia

Non me ne voglia il ministro Fitto, ma desidero che l'Italia esca vincitrice da questa grande sfida chiamata PNRR. Intanto, anticipo subito il voto contrario del Gruppo che rappresento, il MoVimento 5 Stelle. All'inizio, mi ero preparata un intervento, ma poi mi sono fatta prendere da quello da quello del ministro Fitto e volevo dunque argomentare la dichiarazione di voto contraria proprio su alcuni passaggi che ha sottolineato nella sua informativa. Ministro, ripete - l'ha detto anche la presidente Meloni in campagna elettorale in Sardegna e abbiamo visto anche delle faccine un po' particolari - che la rimodulazione del Piano sia stata una cosa impossibile, che tutti abbiamo contrastato. Non credo che le opposizioni di questo Parlamento abbiano contrastato ciò che è previsto dai regolamenti comunitari, perché la rivisitazione del PNRR è prevista da un articolo dei regolamenti comunitari, nel caso in cui ci siano cause oggettive che

Entro il 31 agosto 2023 tutti i Paesi membri dell'Unione hanno ripresentato il PNRR rimodulato. C'era una data stabilita e addirittura noi siamo stati un po' in ritardo. Ricordo ancora le parole del ministro Fitto, che diceva di avere ancora tempo fino al 31 agosto. Quindi qual era questa missione impossibile?

la questione in Commissione. Lei, Ministro, poco fa diceva di non avere memoria di questo coinvolgimento del Parlamento. Ebbene, nella scorsa legislatura proprio la Commissione bilancio ha dedicato mesi a valutare le schede di progetto del PNRR, perché si tratta di programmazione unitaria e il Parlamento ne dovrebbe essere sempre a conoscenza, conoscenza, visto che è lo strumento per eccellenza di indirizzo e controllo di questo e di qualsiasi altro Esecutivo. Signor Ministro, non so se abbia avuto questa nota, ma il 3 agosto ho scritto ai Presidenti delle Commissioni

anche parlato del fatto che nel corso del 2023, proprio per la proficua interlocuzione avuta con la Commissione europea - e di questo le dobbiamo dare atto, ma credo che qualsiasi Governo nel momento *clou* dell'attuazione del PNRR non potesse che interloquire

il decreto-legge citato, per tappare alcuni buchi, ne abbiamo aperti altri tre o quattro. Mi riferisco ad esempio a quei famosi 13 miliardi di euro di progetti definanziati dal PNRR che adesso vengono coperti per intero.

potuto affrontare il definanziamento, senza trovare altre coperture? Lei doveva governare questi processi. Anche se gli errori forse non sono imputabili a questo Governo, sicuramente i Comuni non potevano essere lasciati da soli, perché avremmo visto il loro dissesto immediatamente. Va bene quindi che abbiamo trovato le risorse,

Con la rimodulazione avete letteralmente fatto finta di disegnare un nuovo piano Transizione 5.0 per le imprese. Questo nuovo piano prevede che i relativi crediti d'imposta non saranno cumulabili con nessun altro incentivo, a partire proprio da quelli legati alla ZES unica del Mezzogiorno. Come ben sanno le aziende, questa non cumulabilità finirà per penalizzare soprattutto il Sud, visto che finora le stesse imprese meridionali potevano sommare i crediti d'imposta Transizione 4.0 a quelli del Mezzogiorno, arrivando a coprire anche l'80 per cento delle spese per gli investimenti in risparmio energetico, beni strumentali e transizioni varie. Per non parlare poi del fatto che già i crediti d'imposta per la ZES unica, così come stabiliti dal Governo, hanno tetti che escludono la possibilità di accesso alle piccole e medie imprese del Sud. Di fronte a questa politica economica disastrosa, siamo sicuri che le imprese di tutta Italia non si faranno prendere in giro in modo così smaccato dall'Esecutivo. Si accorgeranno, per esempio, che 6,3 miliardi di euro spacciati dal Governo come investimenti aggiuntivi nel nuovo piano Transizione 5.0 sono tutt'altro che soldi nuovi: rappresentano, invece, il residuo delle risorse già presenti nel PNRR per il piano Transizione 4.0 lasciato in eredità dal Governo Conte II ma non spese dall'attuale Esecutivo, perché ha inizialmente tagliato e affossato quel piano, salvo poi rendersi conto che andava immediatamente reintrodotto. Chiedo però al Ministro nel frattempo quanto tempo abbiamo perso: perso: quanto tempo avete fatto perdere al tessuto produttivo? Se il Paese è a crescita zero e ha undici mesi consecutivi di calo della produzione industriale, si deve a queste gravi manifestazioni di incapacità e incompetenza economica. Tuttavia, un merito oggi al Ministro poco fa ha detto, nella sua relazione, che il credito d'imposta rappresenta per il tessuto imprenditoriale crescita e investimento.

senza considerare il fatto che questo accentramento non è che faccia bene all'Italia, perché prima o poi i nodi verranno al pettine. Magari, con un maggiore coinvolgimento del Parlamento, alcuni nodi potremmo risolverli insieme. Mi riferisco alle entrate minori rispetto alle rate che avremo ora nel 2024, che causeranno qualche problema nella tenuta dei conti pubblici, o anche

alla Transizione 4.0, strumenti messi in campo dal Governo Conte II. *(Applausi)*. Ministri, membri del Governo, colleghi, ieri «Il Sole 24 Ore» ha pubblicato dati inediti di Eurostat e della Fondazione Edison, con tanto di tabella.

Paesi europei, nonostante siamo l'unico Paese ad aver sofferto di un profondo calo demografico. Lo so, è dura accettarlo e ascoltarlo, ma il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 sono gli anni del superbonus, di Transizione 4.0, del potenziamento del Fondo centrale di garanzia delle PMI, del reddito di cittadinanza e del decreto-legge dignità, tutte misure del Governo Conte II.

il PNRR è una grande occasione per l'Italia. Finora le cose stanno andando bene e le battaglie le abbiamo vinte, però bisogna vincere la guerra. Il buon utilizzo dei fondi europei, che - lo ricordiamo - sono nostri, perché l'Italia è da sempre contributore netto, cioè dà più di quello che riceve - quindi è una restituzione di fondi che fanno il giro e tornano

ci sia una forte innovazione nel settore digitale e in particolare i giovani sono molto forti in tale ambito. È quindi importante spendere bene queste risorse e per l'Italia è doppiamente importante, soprattutto soprattutto per l'entità delle risorse che abbiamo chiesto, che ci sono state concesse in massima parte a debito (123 miliardi circa) e vanno restituite. Stiamo già pagando gli interessi: 504 milioni quest'anno, 714 l'anno prossimo, poi via via crescendo e infine arriverà la quota di capitale. Ciò impegnerà tantissimo i bilanci nei prossimi anni, quando, tra l'altro, abbiamo già

Ebbene, è fondamentale che, per riuscire a restituire questi fondi, le risorse vengano spese bene,

quindi restituire queste rate e aver creato uno sviluppo tale da non dover tagliare altra spesa importante, altrimenti avremo fatto una bella frittata.

con soldi presi a prestito, e contemporaneamente tagliare una spesa già adesso. Per tradurre: se nella rimodulazione

utilizziamo in maniera giusta le risorse che ci vengono date a prestito. Cosa succede però dei 10 miliardi che abbiamo tolto? Non li togliamo semplicemente, li rifinanziamo. Perfetto, ma come li rifinanziamo? Lo facciamo tagliando altra spesa già adesso. Allora qui bisogna stare particolarmente attenti e faccio riferimento soprattutto a due fondi che vengono tagliati: i fondi per gli ospedali e i fondi per la qualità dell'aria del bacino padano. Nella replica, il Ministro ha dato risposte che non convincono fino in fondo: c'è un impegno a trovare una soluzione per questi due temi, ma era meglio metterlo nell'atto formale. Resta un impegno importante, era meglio metterlo nell'atto che votiamo. Per esempio, il fondo degli ospedali, che si intitola «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», viene tagliato e il Ministro ci dice che non c'è problema, perché, anziché usare quel fondo che viene tagliato, si usa il suddetto articolo 20, cioè il fondo dell'edilizia sanitaria che c'è ed è finanziato. Fin qui tutto bene, ma c'è un piccolo, grande problema: che succede alle Regioni che hanno già usato la quota di quel fondo? Dove prendono le risorse? Restano a bocca asciutta. Qual è la loro colpa? Aver speso i fondi nei tempi e aver rispettato il piano d'investimento: per questo non avranno i fondi. Per capirci, quelli che rispettano la regola del PNRR, cioè una spesa per investimento da fare nei tempi, restano a bocca asciutta. Non può funzionare così. C'è un impegno a trovare una soluzione e ci auguriamo di trovare nel decreto-legge che è in discussione alla Camera la copertura che trovi questa soluzione,

le Regioni coinvolte le conosciamo tutti: Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia, le quali fanno investimenti per evitare di pagare la sanzione, perché siamo già in infrazione. La sanzione è sospesa, perché si fanno questi investimenti,

l'ammontare delle sanzioni, che aumentano in maniera importante: dai 7,5 milioni base al giorno si passa a quasi 10 milioni al giorno. Quella è la base, diventa molto più alta per infrazioni che riguardano la salute, come nel caso specifico. Parliamo di miliardi di euro di potenziale sanzione. se il Ministro si impegna a trovare una soluzione, siamo tutti d'accordo. Era meglio metterlo nell'atto formale, perché almeno era un atto formale. Abbiamo un impegno - va bene - e ci auguriamo di trovare nel decreto-legge che è in discussione alla Camera la copertura di questo tema, altrimenti resta il taglio.

Il difficile - ahinoi - viene adesso e questo riguarda tutti. Fin qui è programmazione, adesso le cose vanno fatte, i cantieri vanno fatti e bisogna stare nei tempi. Faccio un esempio che è emblematico, Caput mundi. Non so se ve lo ricordate. Nel PNRR c'è un progetto, Caput mundi: mezzo miliardo di euro, 500 milioni di investimenti da fare nel Comune di Roma.

Il difficile, quindi, viene adesso. Finora abbiamo vinto le battaglie, dobbiamo vincere la guerra. Siamo consapevoli che il difficile viene adesso e noi daremo tutto il supporto possibile e immaginabile per arrivare in fondo e spendere benissimo le risorse.

a costruire, ma anche a definire le linee guida del Next generation EU a livello europeo. La grande innovazione di chi crede nell'Europa è stata quella di investire sul debito comune. Era il sogno di Romano Prodi, degli eurobond per finanziare politiche che rispondessero alle grandi sfide che noi, come singoli Stati, non siamo più in grado di portare avanti. Ecco, mi fa piacere oggi sentire le parole del ministro Fitto, che porta la destra sovranista e la destra populista su posizioni pro-Europa. *(Applausi)*. È un passo in avanti e noi apprezziamo questa nuova maturità.

interessava, perché, avendo BBB di *rating*, ci costava molto di più e abbiamo sostituito tutta una serie di progetti con il debito che arrivava fortunatamente dall'Europa. Questo il ministro Fitto non lo dovrebbe spiegare guardando dalla nostra parte, ma dall'altra parte, visto che la Lega ha pur sempre grandi difficoltà ad accettarlo. *(Applausi)*. Anche in prospettiva, se noi vogliamo investire sugli interessi del nostro Paese, abbiamo interesse che quel debito comune e quei tipi di programmi, come Next generation EU, diventino strutturali.

affrontare e sostenere la politica industriale in un momento di grande trasformazione dal punto di vista ecologico e digitale delle nostre economie. Allo stesso modo, il nuovo Sure è stato fondamentale per sostenere la cassa integrazione e la sostenibilità del nostro *welfare* in quel passaggio e, in su uno Sure per quanto riguarda la transizione ecologica, che di certo non sarà un pranzo di gala e sarà davvero complicata. Da questo punto di vista, speriamo di poter investire in questo senso sul debito comune con posizioni pro-Europa.

quanto avvenuto nel 2023 emerge il generale raggiungimento degli obiettivi procedurali consistenti nell'adozione di provvedimenti amministrativi, pubblicazioni di avvisi, stipula di convenzioni con soggetti attuatori ed emanazioni di decreti direttoriali. Tuttavia, sono risultate situazioni di ritardo negli interventi

penso sia importante fare anche un'operazione di chiarezza. Spesso ce la prendiamo con i Comuni, che in molti casi hanno già fatto l'aggiudicazione, hanno aperto i cantieri, hanno firmato i contratti e hanno fatto la revisione dei prezzi delle materie

Noi siamo contenti che il ministro Urso abbia speso il 70 per cento delle risorse, ma sono *bonus*. Il Ministero delle infrastrutture deve costruire infrastrutture ed è molto più complicato. Vogliamo metterli sullo stesso piano? De Luca ha gli stessi problemi che ha il ministro Salvini. Allora, se vogliamo essere seri, dobbiamo raccontare le cose in Fare un'infrastruttura è maledettamente più complicato che fare un bando e assegnare *bonus*: queste mi sembra siano informazioni di base. Dal punto di vista del rifinanziamento delle coperture per i Comuni, siamo arrivati un po' in ritardo, ministro Fitto. il rapporto con ANCI si è chiuso, fortunatamente, con una copertura e un ritorno sui bandi precedenti, però lei sa meglio di me che, rispetto alle linee di bilancio iniziali, passare alle regole del PNRR e poi ritornare indietro non è così facile per i Comuni.

quindi che tutto è ad invarianza. Rimangono gli stessi soldi, ma gli obiettivi al ribasso sono stati mantenuti. Se avessimo voluto mantenere lo stesso livello di ospedali, di comunità e di case di comunità, avremmo dovuto mettere soldi aggiuntivi. Questo lo dico per amore di verità.

funzione, chiediamo di garantire una costante trasmissione al Parlamento di tutte le informazioni necessarie a valutare lo stato di avanzamento del PNRR a livello delle singole schede di progetto, al fine di favorire l'esercizio delle attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

alla Commissione europea. È una cosa che voi non avete mai fatto. Addirittura Fazzolari, Ciriani, l'ex Capogruppo all'interno di Fratelli d'Italia chiedevano di seguire negli stati di attuazione le stesse procedure che si

Non abbiate paura della trasparenza, perché noi, che più di altri abbiamo fortemente voluto questo Piano, siamo interessati al fatto che abbia successo, e al successo la massima trasparenza non ha mai portato danno.

che magari non oggi, ma in futuro possiate accettare di andare incontro alla trasparenza, che è uno degli elementi fondamentali perché il PNRR possa essere attuato negli interessi degli italiani, delle imprese e delle famiglie.

è la seconda volta che ho l'onore di esprimere il voto del nostro Gruppo a seguito di un suo intervento e non le nego che questo mi fa molto piacere, perché il suo compito non era facile. Il suo compito era ed è molto complesso: riuscire a coniugare gli interessi economici connessi al PNRR le possibilità che esso rappresenta per l'Italia in un momento geopolitico complesso, con il vento del disfattismo alimentato da tutta l'opposizione che le soffiava dietro le spalle. Non sarà stato facile tradire le aspettative, riuscire a trasmettere sicurezza, dialogare e convincere tutta l'Europa che che i rappresentanti dell'Italia oggi sono altra cosa rispetto al passato, e i risultati lo dimostrano ampiamente. Nel 2023 l'Italia ha rispettato tutti gli obiettivi della terza rata ereditati dal precedente Governo. Abbiamo presentato gli obiettivi della quarta rata e ottenuto il suo pagamento. Siamo la prima Nazione in Europa ad aver presentato gli obiettivi della quinta rata. *(Applausi)*. Tutto questo è stato fatto mentre si riorganizzava il PNRR e lo si ridisegnava per un semplice motivo: il precedente Piano era stato scritto in un contesto diverso, quindi non poteva tenere in considerazione alcune emergenze che oggi stiamo affrontando, come quelle generate dal conflitto russo-ucraino. Il PNRR è uno strumento e gli strumenti vanno adeguati al mutare del contesto. Sentiamo ancora i profeti di sventura, i nostri avversari politici e i giornali della sinistra dire: non ce la faranno mai; perderanno i soldi del PNRR; sarà un *flop*. Tutti quei signori sono stati smentiti dalla forza dei fatti, dei suoi fatti, signor Ministro, e di questo Governo. È un dato chiaro e oggettivo. I fatti danno ragione a questo Governo che, con la *leadership* di Giorgia Meloni e grazie al ministro Fitto in tema di PNRR, ha instaurato una collaborazione diretta e stretta con la Commissione europea.

Oggi nasce il nuovo Piano di ripresa e resilienza italiano, che è stato rivisto e integrato in stretta collaborazione con la Commissione europea e con tutte le amministrazioni titolari per rafforzarne l'efficacia, per favorire la crescita economica, la tutela dell'ambiente, la coesione sociale e l'efficienza energetica. Il Piano è stato modificato e adattato con il metodo del dialogo. C'è chi preferisce fare piazzate, urlare *slogan* e c'è chi invece lavora in laborioso silenzio cercando di dare risultati alla Nazione e a tutti. Ricordo che il Governo ha assicurato la massima condivisione con le parti sociali, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito della cabina di regia che si è riunita venti volte da settembre. Il nuovo Piano, superando le numerose criticità attuative, consentirà al Governo di sostenere la crescita economica attraverso un più incisivo percorso di riforme e investimenti. Abbiamo liberato 21 miliardi di euro di risorse (in pratica, una seconda manovra economica), in gran parte destinati allo sviluppo e alla complessità del tessuto produttivo. Mi consenta per il suo tramite, Presidente, di sottolineare che

Parliamo di 12 miliardi di euro per gli incentivi alle imprese, di cui oltre sei in Transizione 6.0. Ci sono poi le risorse per gli agricoltori: tra contratti di filiera e di voltaico siamo passati da 5 a 8 miliardi di euro, abbiamo lavorato sull'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese e destinato quasi un miliardo di euro alla alla sanità. Abbiamo quindi adattato il Piano per dare risposta alle esigenze reali del Paese, mentre la maggioranza di sinistra e socialista d'Europa ha approvato misure contro gli agricoltori, svendendoli come i grandi inquinatori da punire. *(Applausi)*. La nostra Nazione ha stanziato risorse aggiuntive per il PNRR, per sostenerli e per sostenere la produzione e il *made in Italy*. Sappiamo tutti che il Piano ha scadenze nette, occorre completare i progetti per un *timing* determinato e si rischia la perdita dei fondi. Da qui ho apprezzato il pragmatismo del ministro Fitto. Alcuni progetti irrealizzabili o non ammissibili sono stati modificati; in particolare, alcuni affidati agli enti locali e che rischiavano di non essere realizzati nei tempi, saranno finanziati tramite altri programmi europei e nazionali invece che con il PNRR, che avrebbe avuto tempistiche molto più stringenti. Le missioni del Piano salgono da sei a sette, con l'introduzione del capitolo REPowerEU. Le riforme, parte essenziale del PNRR e del percorso di modernizzazione della Nazione, passano da 63 a 66. Le sette nuove riforme, cinque delle quali relative al capitolo REPowerEU, includono, tra le altre, il riordino degli incentivi alle imprese, con l'obiettivo di razionalizzare e fornire alle imprese strumenti semplici ed efficaci, politiche di coesione per estendere alle politiche di sviluppo e coesione l'approccio orientato ai risultati del PNRR. Su questo punto, consentitemi un piccolo inciso: l'ottavo rapporto della Commissione europea ci dice che, in materia di politiche di coesione, l'Italia è il primo Paese europeo per ottenimento di risorse, ma il peggiore per le *performance,* sia in termini di qualità sia di quantità della spesa. La riforma delle politiche di coesione non è più rinviabile. Inoltre, avremo un Testo unico per le procedure in materia di energie rinnovabili, per razionalizzare e semplificare il quadro normativo e autorizzativo e si procederà con una riqualificazione dei lavori pubblici e privati per l'innalzamento delle competenze in materia di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. Si introdurranno anche strumenti per le imprese per ridurre il rischio finanziario legato all'acquisto di energia da fonti rinnovabili. Oggi abbiamo la conferma di aver fatto un lavoro di cui l'intera Italia può essere fiera. *(Applausi)*. Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso. Siamo scesi nel concreto, verificando le criticità e le abbiamo superate, facendo in modo che tutti i soldi del PNRR venissero spesi nei tempi e quindi abbiamo concentrato le risorse sulla crescita e sulla modernizzazione della Nazione. Il risultato, sul quale in pochi scommettevano, dice che non era una scelta sbagliata. un Piano finalmente concreto e realizzabile, che ci permetterà di non perdere neanche un centesimo. Questa sfida sullo spendere bene e sullo spendere subito la stiamo vincendo insieme come Nazione e questo può e deve essere un elemento di orgoglio a prescindere da quale casacca politica si indossi, perché stiamo rafforzando i territori e stiamo destinando risorse alla competitività del nostro sistema e delle nostre imprese. Il Governo è impegnato a raggiungere tutti gli obiettivi previsti dalla quinta rata entro la fine dell'anno. Questo risultato si basa anche sulla logica vincente di mantenere un approccio basato sul dialogo, ma molto apprezzato a livello di Unione europea, che sta dando i suoi frutti, restituendo una paventata da chi prefigurava un'Italia isolata a livello europeo e internazionale. Il dialogo viene mantenuto anche a livello interno, con un Governo impegnato nel coinvolgimento di associazioni, enti territoriali, sindacati e portatori di interesse e per noi parlamentari che rappresentiamo proprio le istanze dei nostri collegi elettorali dei territori è un dato di assoluto valore. Il nostro plauso va quindi al ministro Fitto per il lavoro fin qui svolto e all'interno Governo Meloni per una gestione del Piano efficace ed efficiente. La strada è tracciata. Da qui al 2026, l'Italia farà grandi passi in avanti e potremo dire di lasciare al termine del nostro mandato di Governo, che - assicuriamo a tutti i gufi - durerà durerà tutta la legislatura, un'Italia migliore rispetto a quella che ci hanno lasciato i precedenti Governi. Per questo motivo, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Avverto che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto, ha espresso parere contrario sulle premesse ed in parte favorevole, previa riformulazione, sugli impegni della proposta di risoluzione n. 1; parere

necessaria per assicurare la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e in particolare di quelle ad alta velocità nei territori delle Regioni Calabria e Sicilia». Sul punto 7 del dispositivo si propone la seguente riformulazione: «ad assumere ogni iniziativa necessaria ad assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del dissesto idrogeologico

Allegato B)*. Abbiamo così concluso il dibattito sulle comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Come da intesa, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 16.

avente ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 7 del 29 gennaio 2024, indicato in titolo, come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla 1a Commissione nel corso dell'esame in sede referente. L'articolo 1, che è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione, detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione nell'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative. In particolare, il comma 1 dispone che, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024 le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. Nello il comma 2 disciplina le operazioni di votazione delle consultazioni europee, prevedendo che le stesse si tengano nella giornata di sabato dalle ore 15 alle ore 23 e di domenica dalle ore 7 alle ore Il comma 3 detta norme per il caso di abbinamento delle consultazioni per le elezioni europee con un turno di elezioni amministrative o con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali elettorali o referendarie. In tutti questi casi si prevede lo svolgimento delle votazioni nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e di domenica, dalle ore 7 alle ore Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976. In relazione a questa norma segnalo al Presidente e ai colleghi che la Commissione aveva votato all'unanimità un emendamento per incrementare

della Costituzione. Il comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, rinvia al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di Provincia e dei consigli provinciali in scadenza nello stesso anno. La disposizione si applica esclusivamente alle Province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell'intera Provincia. La durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo. L'articolo 1-*bis,* inserito nel corso dell'esame in Commissione, specifica che i funzionari statali, da nominare componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, possono essere sia in servizio sia a riposo. L'articolo 1-*ter,* inserito nel corso dell'esame in Commissione, introduce in via sperimentale una disciplina di esercizio del voto da parte degli studenti fuori sede, con riferimento alle elezioni europee del 2024. Ad essere disciplinato è quindi il voto, per l'elezione nel 2024 dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, degli elettori che, per motivi di studio, si trovino ad avere un temporaneo domicilio per un periodo di almeno tre mesi in un Comune italiano situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. La previsione differenzia il caso in cui il temporaneo domicilio si situi in un Comune diverso da quello di iscrizione elettorale e in una Regione diversa, ma entro la medesima circoscrizione elettorale, dal caso in cui il temporaneo domicilio si situi in un'altra e diversa circoscrizione elettorale. Qualora la circoscrizione elettorale sia la medesima, il voto è esercitabile nel Comune di temporaneo domicilio.

Il voto è esercitato in tal caso presso sezioni elettorali speciali per le liste dei candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore. L'esercizio del voto fuori sede è su domanda, può essere presentata, ai sensi del comma 4, secondo una triplice modalità: personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici. La domanda deve essere indirizzata al Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti almeno trentacinque giorni prima della data di svolgimento della consultazione elettorale ed è revocabile con la stessa modalità entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stessa del voto. Nei successivi commi sono disciplinate nel dettaglio le modalità di esercizio del diritto di voto dei fuori sede e le operazioni di scrutinio. Il comma 22 reca, infine, la quantificazione degli oneri, pari a circa poco più di 614.000 euro, ovviamente per l'anno 2024, in quanto la norma fa riferimento in via sperimentale soltanto all'anno 2024. 2024. L'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. In tal senso, il comma 1 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), intervenendo in particolare sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione dell'anagrafe della popolazione residente e alla determinazione della popolazione legale. Il comma 2 prevede l'adozione di un apposito regolamento governativo volto a modificare le disposizioni del vigente regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989), collegate all'esecuzione del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'Istat. L'articolo 2-*bis*, introdotto sempre in Commissione, prevede che la registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico, o di marche comunque contenenti parole, figure o segni con significato politico, non rilevi ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste, nonché della propaganda elettorale. L'articolo 3, rubricato «Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione», intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di Provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità dell'amministrazione provinciale, sia con riferimento al sistema elettorale applicabile agli stessi. Nello specifico, il comma 1 dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i Comuni capoluogo di Provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, sia quello previsto dagli articoli 72 e 73 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Quindi, si applica sempre il sistema previsto per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il Consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco simbolo si dà luogo a un turno di ballottaggio, qualora nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti. comma 2 introduce una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria. Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della Provincia sia costituita da nome di più Comuni, stabilendo che, in tal caso, il capoluogo sia individuato in ciascuno dei Comuni medesimi. Il comma 4 precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici. L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del Consiglio comunale. 1 modifica l'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, prevede l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.000 a 15.000 abitanti, eliminando al contempo ogni limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Il comma 2, in deroga all'articolo 71, dispone che, per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Si prevede altresì che, qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nella lista elettorale del Comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'AIRE, che non esercitano il diritto di voto. Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i Comuni possono beneficiare delle risorse del Fondo per l'incremento delle indennità dei sindaci. L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, modifica la disposizione vigente in materia di esenzione di firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni europee. In particolare, si prevede l'esenzione dalla sottoscrizione per i partiti o gruppi politici costituiti in Gruppo parlamentare nella legislatura in corso o al momento della convocazione dei comizi, anche in una sola delle due Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale, o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Altresì, l'esenzione vale anche per un partito che abbia ottenuto con il suo contrassegno almeno un seggio nelle ultime elezioni europee, a condizione che sia affiliato a un partito politico europeo, costituito in un Gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che la disposizione che stabilisce l'ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti della Regione per rispettivo Consiglio si applichi esclusivamente ai dipendenti della Regione che svolgano, al momento della candidatura, funzioni e attività amministrative. amministrative. L'articolo 4-*quater*, introdotto sempre nel corso d'esame in Commissione, estende alle firme per le proposte di *referendum* in ambito locale la normativa vigente sulla semplificazione nella raccolta delle sottoscrizioni, consentendo, per esempio, che l'autenticazione possa essere eseguita da avvocati iscritti all'albo che abbiano dato la propria disponibilità. L'articolo 4-*quinques*, introdotto anch'esso durante l'esame in Commissione, prevede che non siano soggetti a ripetizione i trattamenti relativi ad aspettative, permessi ed indennità degli amministratori delle forme particolari più accentuate di decentramento istituite dai Comuni, ai sensi del comma 5, articolo 17, del decreto legislativo n. 267, come determinati dal Comune medesimo e riconosciuti ai componenti componenti delle medesime forme di decentramento fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Altresì si rimette a un decreto interministeriale del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato, città e autonomie locali, la fissazione dei criteri e delle modalità in base ai quali i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari più accentuate di decentramento, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinano una spesa superiore a quella che il Comune può sostenere applicando le tipologie di indennità ai tetti di spesa previsti per gli amministratori delle predette forme di decentramento. L'articolo 4-*sexies,* introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che siano esentate dalla raccolta delle firme per la presentazione alle elezioni regionali le liste che siano espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai Gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento. L'articolo 5 reca la copertura finanziaria. L'articolo 6 attiene infine all'entrata in vigore del provvedimento. **Saluto

in piccola parte - a nostro avviso - condivisibili, in larga parte non condivisibili. Ci sono delle considerazioni di principio che si impongono a mio giudizio, ma anche a giudizio

La prima ha a che vedere con il carattere eccessivamente eterogeneo che in partenza il decreto-legge presenta. Questo aspetto va contro una buona prassi che tutte le forze politiche e tutti i Gruppi parlamentari dovrebbero avere interesse ad affermare perché contribuirebbe a rendere più sana, leggibile e trasparente la nostra attività all'interno delle istituzioni. Troppo spesso ci troviamo di fronte a provvedimenti che nascono iper eterogenei e che escono dal Parlamento ancor più eterogenei. Quindi, durante la conversione parlamentare il problema originario viene aggravato rende più opaco il processo legislativo e ciò contribuisce a ridurre la credibilità del Parlamento. Mi pare che troppo spesso non ci sia sufficiente consapevolezza della gravità di questo problema che, invece, io penso vada sottolineato ogni volta che ci troviamo di fronte alla conversione di un decreto-legge che ha queste caratteristiche. La seconda questione di principio su cui

Quindi, si sta parlando di elezioni che distano, dal momento in cui discutiamo di queste norme, meno di tre mesi. Con il decreto si interviene a operare un accorpamento, condivisibile e del tutto logico, tra elezioni amministrative ed elezioni europee, cosa che, peraltro, è stata fatta per quasi tutte le elezioni europee precedenti e che quindi ormai è una tradizione. Questa operazione la si fa anche per cambiare le regole di eleggibilità. Penso, per esempio, alla possibilità di essere eletti sindaco, che viene modificata per decreto a tre mesi dalle elezioni. Vedremo poi come anche questo si presti a

con un confronto ampio in Parlamento e senza la tagliola che in qualche modo il decreto-legge rappresenta, un intervento organico: non un intervento che sembra calato dall'alto, imposto e quindi avente le caratteristiche quasi di una forzatura, che viene portata avanti senza tener conto a sufficienza delle prerogative del Parlamento. Ci sono nel provvedimento, ovviamente, delle misure che riteniamo giuste. Ho parlato dell'accorpamento della data delle elezioni amministrative con le elezioni europee.

di legge sui fuori sede il suo percorso naturale in tempo utile. Ma è comunque giusto il tentativo di dare una prima risposta alla questione del voto per chi si trova, per ragioni di studio, lontano dalla Regione di residenza e, in molti casi, sostanzialmente impossibilitato a votare. Si fa un primo tentativo, dandogli però la caratteristica di una sperimentazione. Quindi, benché non possiamo certamente dirci contrari a questa scelta, dobbiamo sottolinearne il carattere estremamente asfittico, perché è una scelta che non ha nessun respiro, che non ha nessuna organicità, che si riferisce soltanto al Parlamento europeo. Non si capisce, infatti, perché questo diritto lo si possa affermare solo per il Parlamento europeo e non anche per le elezioni di Camera e Senato e per i *referendum*. *(Applausi)*. Non si capisce perché debba valere soltanto per gli studenti e non anche per chi si trova lontano dalla Regione di residenza per ragioni di lavoro e di cura. Si dice che è una misura sperimentale, ma non va bene. Qui c'è veramente poco da sperimentare: qui c'è una vergogna da sanare, e non delle invenzioni da fare. Cosa dobbiamo sperimentare? In tanti altri Paesi questo problema è pacificamente risolto con mezzi collaudati. Non si capisce perché in Italia dovrebbe essere difficile e meritevole di chissà quale sperimentazione una misura che potrebbe andare avanti sostanzialmente *de plano*. Una questione che, invece, ci convince molto poco, e anzi che riteniamo pericolosa per il nostro sistema istituzionale, è l'intervento che è stato fatto sui limiti di mandato dei sindaci per quanto riguarda i Comuni sotto i 5.000 abitanti. Qui si pone un problema di merito e di principio. Il problema di merito che si pone è il seguente. Come possiamo pensare che possa funzionare nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, e quindi in territori dove il contatto tra amministrati e amministratori è molto stretto e dove le possibilità di condizionamento di chi esercita il potere sono massime, si possa avere l'elezione diretta ad una carica monocratica di governo sostanzialmente un numero infinito di volte? Sostanzialmente, si può fare il sindaco a vita: dove sta la logica di tutto questo? Guardate che chi chi fa questo pensando di rafforzare l'elezione diretta del sindaco, nella quale dal 1993 in tanti hanno creduto e in cui anche noi continuiamo a credere, in realtà non si accorge che sta portando argomenti

Il Ministro ora è al telefono. Siccome sto parlando di una cosa importante, mi fermerei in attesa che finisca la telefonata. Ripeto, è una cosa importante. a noi suscita molta inquietudine il fatto che, nonostante i nostri appelli, si sia deciso deciso di andare avanti con l'approvazione di una norma, ossia l'abolizione del limite dei mandati nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, che è in palese contrasto con una recentissima sentenza della Corte costituzionale. Mi riferisco, signor Ministro, alla sentenza n. 60 del luglio 2023. Mi domando come si possa intervenire con un decreto-legge in materia sapendo che c'è una sentenza della Corte costituzionale che dice che assolutamente l'elezione diretta di un organo monocratico di governo deve avere un limite di mandati. La sentenza della Corte non dice il il numero del limite, che lascia alla discrezionalità politica, ma dice che la limitazione dei mandati è un temperamento di sistema necessario a fronte dell'elezione diretta. A nemmeno un anno di distanza, il Parlamento si trova di fronte a un decreto-legge del Governo che fa finta che questa sentenza della Corte costituzionale non esista e che legifera in maniera incostituzionale. Lo voglio dire a quelli che oggi voteranno a favore *(Applausi)*: è palese che questa norma è incostituzionale. Basta leggere la sentenza, che non è del 1973: è la n. 60 del 2023. Quindi la maggioranza oggi e chi, insieme alla maggioranza, voterà questo provvedimento si assumerà la responsabilità di legiferare in maniera incostituzionale, nonostante gli avvertimenti dati dall'opposizione e sapendo che probabilmente questa norma sarà portata da un giudice all'attenzione della Corte costituzionale e sarà dalla stessa cassata. Devo dire che questo non è il modo di onorare il lavoro nelle istituzioni e nemmeno la credibilità L'ultima cosa che dico riguarda un fatto del quale siamo venuti a conoscenza pochissimi minuti fa. Mi viene detto che c'è un emendamento - ora siamo in discussione generale e torneremo sul tema in occasione della discussione

a tre mesi dalle elezioni si interviene in maniera unilaterale - primo problema - per decreto-legge, secondo problema. Il terzo problema: con un emendamento che non è stato presentato in Commissione e che viene depositato *in extremis* in Aula alla chetichella e surrettiziamente, in modo da impedire ogni seria discussione. Con questo emendamento si stravolge una legge elettorale, quella del 1993 sui sindaci, che nei trentuno anni dalla sua approvazione ha sempre goduto di uno *status* privilegiato, ossia il seguente: non è mai stata modificata da nessuna maggioranza *pro tempore* in maniera unilaterale.

Vi invito caldamente a fermarvi, come già altri hanno fatto in questi minuti. Sappiate che, se questa cosa non viene stoppata, siamo di fronte non ad una forzatura, ma a un vero e proprio colpo di mano antidemocratico *(Applausi)*, perché non si cambiano le regole del gioco gioco in questa maniera e con un modo di agire fraudolento, furbacchione e disonorevole per il Parlamento, in cui questo tentativo si consuma, e per chi ci mette le impronte sopra.

oggi convertiamo in legge il decreto-legge n. 7 del 29 gennaio 2024 riguardante le disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali del 2024, le revisioni delle anagrafi delle popolazioni residenti e la determinazione della popolazione legale. Questo provvedimento è stato esaminato nella Commissione affari costituzionali di cui faccio parte. Il decreto si compone di sei articoli e l'intervento normativo ha l'obiettivo di definire alcuni aspetti tecnici, ma soprattutto ha la responsabilità

È previsto un allungamento per le operazioni di voto anche nella giornata di lunedì, per le europee l'anticipazione è al sabato; è previsto il differimento delle elezioni dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali al 29 settembre 2024 nelle Province in cui il numero dei Consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell'intera Provincia. Sono disciplinate le revisioni delle anagrafi delle popolazioni residenti, è prevista la registrazione dei simboli politici come marchi di impresa, sono previste norme elettorali applicabili ai capoluoghi di Provincia e relativa denominazione, ulteriori disposizioni in materia di elezioni di sindaco e consigli comunali. È prevista anche l'esenzione delle sottoscrizioni di firma per le elezioni europee per il partito che abbia ottenuto con il suo contrassegno un seggio nelle ultime elezioni europee. Viene introdotta l'ineleggibilità di dipendenti della Regione alla carica di consigliere regionale per il rispettivo Consiglio, ove svolgano funzioni ed attività amministrative e in ambito di proposte referendarie viene estesa l'applicabilità della disposizione che individua una serie di soggetti ulteriori rispetto ai notai per l'autenticazione delle firme. Noi parlamentari abbiamo il dovere di arricchire la legiferazione e approvare i provvedimenti finali, senza dimenticare però di inserire misure utili ed efficaci che impattano nel quotidiano degli italiani. Mi soffermo, quindi, su un tema importante: il voto degli studenti fuori sede. La destra giovanile e Fratelli d'Italia sono stati sempre sensibili al tema. L'onorevole Fabio Roscani, che è anche presidente di Gioventù Nazionale, ha dialogato con i comitati degli studenti, ha spiegato loro le tante criticità tecniche, ma ha assunto un impegno che oggi onoriamo. Vorrei ricordare che il problema è stato posto sin dal 2009 e che i vari Governi precedenti nulla hanno fatto sino ad oggi. Prima di illustrare l'emendamento votato in Commissione, ci tengo però a spiegare un passaggio precedente. Alla Camera, a luglio scorso, è stato approvato un disegno di legge che conferiva una delega al Governo da esercitare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Il tema è la disciplina del voto degli elettori che per motivi di studio, di lavoro e cure mediche si trovano in un Comune diverso da quello di residenza. In Senato, abbiamo cominciato l'*iter* a gennaio e il Presidente della Commissione ha incardinato il provvedimento e fissato subito le audizioni a tempi di *record.* Abbiamo ascoltato tutte le criticità emerse, soprattutto quelle illustrate dal prefetto Angelo de Prisco, direttore per i servizi elettorali, vice capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Abbiamo ascoltato i comitati degli studenti e proprio per non deludere loro abbiamo preferito, senza illuderli, preparare un emendamento al decreto elezioni, così da mettere in atto un sistema sperimentale che consentirà già dalle europee 2024 almeno ai giovani di poter votare. Questo metodo sarà applicato per chi, per motivi di studio, è temporaneamente domiciliato per un periodo di almeno tre mesi in un Comune italiano situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Il voto è espresso per le liste dei candidati della circoscrizione di appartenenza, la domanda è presentata trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle consultazioni ed è revocabile entro venti giorni prima delle consultazioni; in ogni capoluogo di Regione saranno istituite sezioni speciali elettorali; presso ogni sezione è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori. Per votare, oltre al documento di riconoscimento valido e alla tessera elettorale, occorre l'attestazione di ammissione al voto. Pertanto, gli elettori studenti fuori sede hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal Comune di domicilio al capoluogo di Regione e ritorno per l'esercizio del voto.

Ringrazio la Commissione affari costituzionali per il lavoro svolto e tutti i Gruppi politici che hanno votato e posto la firma sull'emendamento proposto da Fratelli d'Italia. Prima di concludere il mio intervento, signora Presidente, per amore della verità e soprattutto per correttezza e onestà intellettuale rispetto ai giovani che sono il nostro futuro, ci tengo a rispondere ai colleghi delle opposizioni che in Commissione questo passo e pochi minuti fa il collega Parrini lo ha definito una vergogna. Signora Presidente, per il suo tramite ringrazio il collega Parrini per questa affermazione, perché innanzitutto è un'ammissione di immobilismo dei Governi precedenti di cui un po' tutti hanno fatto parte, soprattutto il PD. Lo ringrazio perché in realtà con questa affermazione si conferma che il primo passo importante verso le esigenze dei giovani lo fa il Governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni. Pertanto, siccome su ogni provvedimento, su ogni iniziativa portata avanti da questa maggioranza c'è una narrazione creativa, smettiamola di giocare e strumentalizzare i giovani: le matite per votare per le europee 2024 per gli studenti fuori sede sono pronte grazie alla concretezza e alla determinazione di Fratelli d'Italia.

sopraggiunta negli ultimi minuti. Sono molto colpito da questo nuovo tentativo, che c'era già stato alcuni mesi fa quando discutevamo del ritorno al voto popolare nelle Province,

Non voglio nemmeno affrontare una discussione di merito, anche se sono profondamente contrario nel merito a questo emendamento; desidero però dire che in questo caso sono davvero particolarmente colpito

il Presidente e anche i colleghi della Commissione, io sono uno di quelli che, fortunatamente non da solo, in questi mesi portano avanti in quella Commissione battaglie politiche su questioni di prima grandezza, come l'autonomia differenziata e il premierato. Ciò nonostante, ho sempre riconosciuto, in particolare alla Presidenza, ma anche ai colleghi e alle colleghe che ne fanno parte, un senso delle istituzioni significativo e comunque il tentativo di stare sempre nel merito delle questioni. Siccome parliamo di questioni rilevantissime

fosse un luogo dentro al quale è possibile sviluppare una discussione seria. Il fatto che un punto così serio, che riguarda un cambiamento davvero di non poco conto dell'assetto istituzionale dei Comuni, non sia stato affrontato in queste settimane in Commissione e

come ritengo, i presupposti per considerare inammissibile questo tipo di emendamento che è stato presentato. Naturalmente non è mio mestiere parlare di questo, almeno in questa sede. Ancora, sugli elementi di criticità, vorrei dirlo con vorrei dirlo con grande chiarezza: condivido molte delle riflessioni che ha fatto il collega Parrini pochi minuti fa. Lo dico affinché resti agli atti: noi come Gruppo, o meglio come componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, ma in ogni caso come sensibilità politica dell'Alleanza Verdi e Sinistra,

che quasi solennizza la possibilità di avere sindaci a vita. Mi sembra davvero il retaggio di un tempo che fu, che non vorremmo che mai si ripetesse. Devo dire che sono anche molto critico rispetto all'ipotesi di allargare il numero dei mandati da due a tre nella fascia di Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Penso che due mandati consecutivi sia invece una norma democratica che serva a tenere il sistema. Penso che sia completamente campato in aria il paragone tra i parlamentari e i sindaci, non foss'altro per il fatto che i sindaci sono evidentemente organismi monocratici, differentemente dai parlamentari. Penso che quando si parla di organismi monocratici, vale per il *Premier*, se dovesse passare - naturalmente spero di no - la riforma del premierato e vale per i sindaci, quello di due mandati consecutivi sia un giusto limite. Ancora, molto rapidamente, perché vedo che sto finendo il tempo, sui fuori sede penso che si potesse fare meglio. Credo anche che il lavoro che è stato fatto, secondo me molto importante, delle associazioni dei fuori sede, che si sono mobilitate nel corso di questi mesi per chiedere la rapida approvazione di questa norma, abbia comunque obbligato le forze politiche e il Governo a venire incontro a quelle richieste giuste e sacrosante. Penso sinceramente che si potesse fare meglio, sia nel senso di favorire una maggiore praticità, perché il meccanismo di partecipazione al voto per gli studenti fuori sede - mi pare di poter dire - è leggermente farraginoso, per usare un eufemismo; penso anche che sarebbe stato giusto, come peraltro chiediamo in una serie di emendamenti che tutte le forze di opposizione hanno tutte le forze di opposizione hanno presentato, estendere questa possibilità che viene data, anche se in maniera ancora troppo limitata, ai fuori sede, anche ai lavoratori, ai pazienti

conclusione, trovo eccessivamente restrittiva - l'ho detto tante volte in Commissione e anche su questo ho presentato un emendamento - la normativa che ridisegna la possibilità di presentarsi alle elezioni europee. La considero sbagliata nel metodo e nel merito: nel metodo, perché credo che sia sbagliato cambiare le norme a pochi mesi o addirittura a poche settimane dal voto; nel merito, perché penso che sia troppo ristretta la possibilità di presentarsi alle elezioni, soprattutto per chi è fuori dal Parlamento. Vedo che c'è un emendamento che riduce il numero delle firme: questo mi sembra comunque un passo in avanti positivo, ma anche su questo probabilmente si doveva evitare una forzatura che nel corso delle giornate passate c'è stata

nel provvedimento al nostro esame ci sono delle forti criticità che non possono restare nell'ombra, soprattutto se le guardiamo in un contesto più ampio. Un contesto in cui si stanno delineando indirizzi politici che sembrano voler rafforzare il potere nelle mani di poche persone, escludendo dalla partecipazione democratica i cittadini. In questo decreto-legge si interviene sul terzo mandato, togliendo il limite del secondo mandato nei Comuni che hanno meno di 15.000 abitanti, non si prevede alcun limite di mandato nei Comuni che hanno meno di 5.000 abitanti e si legittimano di fatto anche le assunzioni preelettorali perché viene sostanzialmente bocciato un emendamento del MoVimento 5 Stelle che voleva contrastare questo fenomeno evidentemente di natura propagandistica, che possono adottare i sindaci uscenti.

il rafforzamento delle cariche monocratiche, a partire dal sindaco, creando una sorta di figura rafforzata del sindaco, per arrivare poi ai governatori delle Regioni. Magari per questo non vi siete messi d'accordo in maggioranza, però già con l'autonomia differenziata qualche potere in più glielo state conferendo. Arrivate poi, alla fine, all'idea del premierato. premierato. Presidente, questi super sindaci, però, almeno considerando le esternazioni di un deputato della Lega, insieme ai loro assessori e a qualche loro amministratore, saranno gli unici a potersi candidare alla Camera dei deputati perché volete vietare ai cittadini di candidarsi se non hanno già precedentemente svolto il ruolo di sindaci, di assessori o di amministratori locali.

un attacco alla democrazia e allo Stato di diritto. State modificando l'impianto dei valori della nostra Costituzione, una bomba atomica nell'assetto istituzionale, e lo fate in vari provvedimenti, a partire da questo decreto-legge. Vogliamo parlare anche di cosa stiamo facendo parallelamente. Questo infatti è ciò che stiamo facendo in Commissione affari costituzionali, ma parallelamente a questo rafforzamento dei super sindaci, c'è anche il progetto di riforma sul premierato.

sotto lo *slogan* che esso sarà eletto dai cittadini, tacendo che però sarà un Presidente del Consiglio che non è quello che siamo abituati a vedere oggi. Sarà infatti un Presidente del Consiglio che potrà fare il brutto e il cattivo tempo, potrà fare ciò che vuole, potrà tradire le promesse elettorali e nessuno lo potrà sfiduciare. Cosa ancor più grave, perché io vorrei parlare proprio delle linee politiche che si stanno seguendo e non limitarmi soltanto a questo decreto-legge, parallelamente a tutto questo, c'è anche un attacco alle alte cariche istituzionali. Si stanno facendo provvedimenti che diminuiscono i poteri del Presidente della Repubblica e si stanno togliendo poteri al Parlamento. Ditemi voi che cosa potrà fare il Parlamento. Vi siete anche rifiutati di approvare un emendamento sull'articolo 77 della Costituzione che cercava almeno di porre a freno la sistematica usurpazione del potere legislativo. Ditemi voi che cosa potrà fare un Parlamento che non potrà sfiduciare il *premier* eletto; cosa potrà fare un Parlamento che già oggi si occupa solo di decreti-legge oppure di disegni di legge di natura governativa. Ci sono già solo in Senato quasi mille disegni di legge di origine parlamentare e non c'è spazio perché si possa sperare che vengano esaminati, entrando a far parte del dialogo democratico. Presidente, la democrazia è fatta di equilibri. Nel mondo del diritto esiste un simbolo che è quello della bilancia. Nel mondo politico e nel sistema democratico dovremmo immaginare di poter prendere a prestito quel simbolo. La bilancia serve proprio per misurare i pesi e i contrappesi e vedere se esiste davvero un equilibrio tra i poteri dello Stato. Se l'ago della bilancia non si trova al centro, non possiamo parlare di democrazia, perché la democrazia si regge sulla divisione dei poteri. Lo Stato di diritto si regge sulla divisione dei poteri.

Il mito dell'uomo forte non deve essere un vanto. Sì, posso capire che sia molto seduttivo. L'uomo forte è chi rassicura; è chi ci protegge. Ci toglie la libertà, ma ci dà sicurezza. Rispecchia un po' l'archetipo del padre che abbiamo interiorizzato e che, se da un lato ci comanda, dall'altro ci dà questo senso di protezione. Ma questa è una debolezza. Se abbiamo bisogno dell'uomo forte, dobbiamo interrogarci sulle nostre fragilità interne. Noi rinunciamo alla nostra libertà per consegnarci all'uomo forte, che rappresenta in qualche modo il padre. Ma siamo o non siamo un popolo di maggiorenni? O abbiamo ancora bisogno di un padre, dell'uomo forte, del sindaco forte, del *premier* forte? forte? Se non riusciamo ad emanciparci da questa idea e continuiamo a insistere con il rafforzamento delle cariche monocratiche, almeno cerchiamo di capire quali possono essere i rischi della concentrazione del potere. Cerchiamo di capire quali sono i rischi che ci ha insegnato anche la storia. Nessuno può dare la garanzia che un sindaco eletto, un governatore eletto o un Presidente del Consiglio eletto corrispondano realmente all'immagine che hanno dato di sé. Esistono tecniche di manipolazione delle masse contro le quali non abbiamo ancora acquisito gli anticorpi. Oggi vanno di moda le promesse elettorali su cose che si sa benissimo

Hitler e alla sua ascesa al potere. Potevano riconoscerlo? Sì. Bastava andare a un comizio di Hitler per rendersi conto che parlava di razza ariana, di eroi alti, biondi e muscolosi:

Colleghi, io credo che il problema della democrazia oggi sia un altro. Noi non dobbiamo rafforzare il potere, dobbiamo arginarlo; perché il potere monocratico si sta espandendo, sta togliendo potere ai cittadini, sta togliendo potere a chi rappresenta i cittadini in quest'Aula. Ci si sta sottraendo al dialogo democratico. Colleghi, propongo Non parliamo di democrazia, perché quella che state disegnando è soltanto una democrazia di facciata. Dietro questo disegno, alla fine, si nasconde una modalità autoritaria, che non disdegna neppure il manganello, quando serve, e che preferisce l'uomo forte e l'autoritarismo rispetto al dialogo democratico, al confronto e a ciò che dovrebbe rappresentare oggi la democrazia. È iscritto a parlare il senatore De Priamo. con questo decreto, relativo alle consultazioni elettorali per l'anno 2024, si prevedono una serie di interventi che sono tutti legati da un comune denominatore, che è quello di estendere la partecipazione democratica, in particolar modo per quanto riguarda le consultazioni dell'anno in corso, a partire anche dall'estensione, per quanto riguarda le elezioni europee, del voto al sabato, che sicuramente consente una maggiore partecipazione. Così come vi sono altri provvedimenti, come quello di proroga del voto per le Province, che sono legati al buon senso e alla razionalizzazione degli appuntamenti elettorali, anche se nel caso delle Province, ad oggi, attraverso una forma indiretta.

rispetto all'inserimento in questo come in altri provvedimenti di norme ulteriori attraverso il lavoro di Commissione e attraverso la presentazione di un emendamento. Non da oggi ma da molti anni, sicuramente con delle ragioni, si critica l'eccesso di decreti.

che in questa legislatura, con questo Governo e con questa maggioranza, vi è assoluta attenzione alle istanze che provengono dal Parlamento. In questo provvedimento lo si vede in modo plastico.

per Comuni sempre di piccole dimensioni. Eppure lo stesso Partito Democratico presenta documenti, fa riunioni e agenzie che chiedono addirittura il terzo mandato per i governatori delle Regioni. Quindi ci chiediamo se il Partito Democratico che dice certe cose in 1a Commissione sia lo stesso Partito Democratico che ne dice altre alle agenzie. O è un caso di omonimia oppure c'è una certa schizofrenia politica. Oltre a ciò, in questo provvedimento ci sono altri interventi, anche attraverso l'attività emendativa, sicuramente interessanti e validi, come ad esempio quello sul tema del decentramento

il Parlamento sarà coinvolto a fare. Cito inoltre le norme per la semplificazione delle firme per le elezioni europee, sulle quali il collega Lisei ha fatto un attento lavoro emendativo. Indubbiamente, come è stato già detto dalla collega Spinelli, quello che dà un forte significato politico a questo provvedimento è l'inserimento, per la prima volta nella storia repubblicana, del voto dei fuorisede alle prossime elezioni europee.

forse pensava che fosse una sorta di trappola per il Governo, per poter poi dire: abbiamo votato tutti insieme alla Camera, ma voi non siete stati in grado di consentire il voto ai fuorisede. Ci dispiace se qualcuno pensava che il Governo cadesse in questa trappola. Il Governo invece è riuscito alla grande a conseguire questo obiettivo e quel mezzo milione di giovani elettori potrà votare, potrà aumentare la partecipazione democratica e il protagonismo dei giovani nella nostra Repubblica. Di ciò va dato atto al grande lavoro che ha svolto il Governo, in particolar modo con la sottosegretaria Wanda Ferro, che va ringraziata (lo ha fatto già la collega Spinelli), con il presidente Balboni, con un lavoro di tutti, di squadra e della Commissione. consentito di raggiungere questo obiettivo; un lavoro serio e approfondito, con il coinvolgimento degli uffici, affinché fosse realmente raggiungibile

fare qualcosa di concreto per aumentare e far tornare la passione politica e la passione civica, e combattere quello che di fatto era un astensionismo involontario, quello di migliaia e migliaia di giovani studenti universitari che oggettivamente avevano una difficoltà reale a compiere viaggi della speranza di migliaia di chilometri o centinaia di chilometri semplicemente per poter esercitare un loro diritto. Certo non era un obiettivo facile da raggiungere, ma questo Governo e questa maggioranza ci sono riusciti. Avviandomi a concludere l'intervento, ci viene anche da sorridere quando alcuni esponenti, in questo caso di tutti i Gruppi di opposizione, invece di essere contenti, di mostrare soddisfazione per il grande obiettivo che abbiamo raggiunto, ci dicono che però si doveva estendere questo diritto anche ai lavoratori e ai malati. ci faccia sorridere perché non sia un obiettivo giusto, anzi ci lavoreremo, ci stiamo già lavorando e sicuramente è un altro obiettivo da raggiungere. Ma questo atteggiamento ci ricorda un po' quelli che a Roma vengono soprannominati i più uno, cioè quelli che rilanciano sempre, ma sempre quando sono gli altri a dover fare. *(Applausi. Voi rilanciate, noi agiamo e scriviamo una grande pagina per favorire la partecipazione e il protagonismo dei giovani nella vita politica. A voi lasciamo tranquillamente il ruolo del più uno. Noi continuiamo a governare l'Italia con il massimo dell'impegno e della responsabilità. *(Applausi)*.

Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, nell'esaminare questo provvedimento credo che sia utile partire dal suo titolo: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale». un provvedimento che avrebbe, dunque, la funzione di fissare alcune disposizioni essenziali, la data delle elezioni e la revisione dell'anagrafe della popolazione e che invece, oltre che venire adottato con un decreto-legge di cui non si comprendono né la necessità, né l'urgenza, viene utilizzato per introdurre norme del tutto eterogenee che introducono, appunto, modifiche strutturali del sistema di governo degli enti locali, le quali invece richiederebbero un ampio e approfondito dibattito parlamentare. Questo, dunque, è il punto di partenza. Ancora una volta la maggioranza ignora il richiamo reiterato della Corte costituzionale alla necessaria omogeneità dei decreti-legge e al dovuto rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Ancora una volta questa maggioranza non ascolta le parole del presidente Mattarella, che in numerose occasioni ha invocato la necessità di attenersi al Dettato costituzionale al fine di preservare l'equilibrio delle istituzioni alla base della nostra democrazia parlamentare. Questo provvedimento, in realtà, è un ulteriore tassello alla vostra ormai costante tendenza ad alterare l'equilibrio delle istituzioni e nelle istituzioni, a giocare con le istituzioni, in altri termini. Mi riferisco anzitutto alle modifiche relative al limite dei mandati, che viene del tutto abolito per i sindaci dei Comuni sotto i 5.000 abitanti e portato a tre dai due attuali per i sindaci dei Comuni sotto i 15.000 abitanti. Mi chiedo e vi chiedo quale sia il senso di un intervento così parziale, che rischia di alterare un equilibrio che finora è stato assai efficiente. L'indicazione programmatica che si legge dietro queste modifiche è chiara ed è opposta rispetto alle esigenze di funzionalità democratica delle istituzioni locali e di rispetto dell'equilibrio dei poteri. Ciò che vorreste approvare, infatti, è semplicemente l'allentamento di un limite a una fortissima concentrazione di potere in capo a cariche monocratiche, ovvero i sindaci; un un limite che trae origine dalla legittimazione, appunto fortissima, che il rapporto immediato - nel senso letterale del termine, senza mediazioni tra elettori ed eletti - conferisce ai sindaci. Per questa esigenza di temperamento di sistema, per citare la Corte costituzionale, esiste il limite dei mandati, senza il quale o attenuando il quale si producono effetti del tutto negativi, a maggior ragione in contesti piccoli o piccolissimi: concentrazione di potere, clientelismo, effetti distorsivi sulle elezioni successive. Sono parole che ha usato il Consiglio di Stato già nel 2008 e più di recente la Corte costituzionale ha ribadito gli stessi concetti con la sentenza n. 60 del 2023. Non è difficile prevedere - lo diceva prima il collega Parrini - che la Corte costituzionale sarà chiamata a ribadirlo quando chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale di questa norma che elimina del tutto il limite dei mandati per i sindaci dei Comuni sotto i 5.000 abitanti. La realtà è che - come fate da mesi con autonomia differenziata e premierato - avete usato questo provvedimento per i vostri giochi politici. Mi riferisco, in particolare, al balletto sul terzo mandato, che si riferisca ai sindaci o ai Presidenti di Regione; un balletto sulla pelle delle istituzioni, nel quale dietro ogni proposta c'erano e ci sono un nome e un cognome, un partito, una corrente di partito. Su questo tema anche il partito di cui faccio parte, il Partito Democratico, ha avuto e ha una discussione che è approdata a un punto chiaro. Primo: occorre discutere in maniera organica le possibili modifiche e i possibili miglioramenti al testo unico degli enti locali; secondo: si può discutere sul limite dei mandati se si ridiscute il tema dell'elezione diretta. Lo dico per come la vedo io: il limite dei mandati si può attenuare, si può persino abolire, se e solo se si elimina l'elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti di Regione. Queste sono le ragioni per cui, in queste condizioni e a legislazione vigente, il nostro è un no netto al terzo mandato. Dal mio punto di vista, credo che occorra fare molta attenzione a toccare un modello, in particolare quello dell'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, disegnato dalla legge Ciampi del 1993, che funziona molto bene. I cittadini eleggono il sindaco e i consiglieri comunali e hanno chiari i meriti e le responsabilità di chi è chiamato a governare, di chi hanno scelto per governare. Certo, è un meccanismo che può essere migliorato, in particolare sotto il profilo del peso sempre più ridotto che hanno assunto e assumono le assemblee elettive. Dunque, qual è la linea di tendenza che dovremo adottare nell'aggiornamento dei meccanismi elettorali e delle regole relative al governo di Regioni e Comuni? A mio avviso, è necessario non alterare i meccanismi che danno stabilità, rafforzando al contempo il peso delle assemblee elettive, dei consigli comunali e dei consigli regionali, elementi chiave per assicurare la rappresentanza e il pluralismo politico, sociale e territoriale. Voi, invece, cosa fate? Come dimostra l'impostazione che date alla riforma costituzionale sul cosiddetto premierato, voi, questa destra al potere, avete in mente un potere sempre più concentrato su una persona, su un capo tendenzialmente assoluto. In questo Parlamento è evidente a tutti che il problema è lo svuotamento di poteri e di funzioni dei rappresentanti dei cittadini: di noi parlamentari e del Parlamento come tale. Occorrerebbe allora intervenire per superare questo limite, sia nei rapporti tra Governo e Parlamento, sia intervenendo sulla legge elettorale che può conferire più o meno forza in questo momento pochissima forza - ai rappresentanti del popolo. Occorrerebbe al contempo rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio nell'ambito della forma di Governo parlamentare. Voi, al contrario, volete stravolgere l'attuale forma di Governo (parlamentare, appunto), concentrando tutti i poteri in capo al Presidente del Consiglio e annullare sostanzialmente il potere del Presidente della Repubblica, la sua di garante dell'unità nazionale. È un progetto pericoloso, che noi stiamo contrastando qui in Senato giorno per giorno e che, ne sono certo, se non muterà radicalmente, i cittadini considereranno per quel che è: un pericolo per la nostra democrazia, perché non aumenta l'efficienza delle istituzioni, ma semplicemente comprime oltre ogni limite il peso del Parlamento e del Presidente della Repubblica e, dunque, dei cittadini medesimi. il mio intervento su una nota positiva. Sebbene si tratti di un intervento sperimentale e per larghi tratti insufficiente, il provvedimento in esame istituisce per la prima volta il diritto degli studenti fuori sede di votare laddove studiano. È una battaglia che, insieme ai comitati come "Voto dove vivo", "The good lobby" e altri, combattiamo da molti anni. Io oggi ho trovato una mia proposta di legge, presentata alla Camera nel gennaio 2014 e sottoscritta insieme a me dai deputati che allora erano i più giovani di quel Parlamento, Anna Ascani, Enzo Lattuca, c'era qui anche il più o meno giovane collega Lorenzo Basso insieme ad altri colleghi. Fu una battaglia che non ebbe successo in quella legislatura e neppure in quella successiva (la scorsa). Il fatto che oggi si segni un primo punto, che si istituisca questo diritto che ampia gli spazi della democrazia e della partecipazione, ci deve far riflettere sulla circostanza che nell'attività parlamentare le buone battaglie possono richiedere anche molti anni; ma, se giocate con tenacia e con pazienza, possono essere coronate da successo e quando lo sono, come oggi, si prova una grande soddisfazione. Certo, ci sono molti limiti nella norma che viene proposta alla nostra approvazione, rispetto alla quale noi presentiamo degli emendamenti migliorativi. Penso, anzitutto, al fatto che si applica solo alle elezioni europee, mentre potrebbe estendersi anche le elezioni politiche e in seguito anche alle elezioni regionali e comunali. In secondo luogo, penso al fatto che, se si è domiciliati fuori dalla propria circoscrizione, si può votare solo nel capoluogo di Regione e ciò renderà complessa l'operazione. Infine, un altro limite è rappresentato dal fatto che la misura - per questo presentiamo specifici emendamenti - non si estenda alle persone che vivono lontano dal luogo di residenza per ragioni di lavoro o di cura. Come dicevo, in questa sede abbiamo presentato emendamenti che speriamo siano approvati, ma continueremo comunque a lavorare - lo ha fatto in questi anni, in particolare, il collega Andrea Giorgis, sia nella scorsa che in questa legislatura - per estendere i diritti dei cittadini e delle cittadine a partecipare col voto alla vita democratica, contrastando così l'astensionismo. Ad ogni modo quella di oggi è una bella pagina per la nostra democrazia, collega De Priamo. Quindi, non critico questa norma: è una bella pagina per la nostra democrazia e per le nostre istituzioni, di cui sono particolarmente felice e orgoglioso. Purtroppo, questa pagina si inserisce all'interno di un provvedimento che altera l'equilibrio dei poteri nell'ambito dei Comuni. C'è anche il pericolo che vengano discussi emendamenti totalmente fuori contesto, che alterano persino il *quorum* per l'elezione al primo turno dei sindaci. Lo diciamo chiaro: si tratta di un tentativo gravissimo di modificare le regole del gioco in un provvedimento con il quale questa norma non ha alcuna attinenza. Noi ci appelliamo al presidente La Russa, perché impedisca questo scempio e, se necessario, lo faremo anche con il Presidente della Repubblica. Non siete i padroni delle istituzioni, non siete i padroni di questo Parlamento che noi abbiamo il dovere di difendere, come difendiamo con tutta la nostra fermezza le regole della nostra democrazia. Purtroppo questo è un provvedimento segnato dal fatto che, appena passa una legge decreto-legge da convertire, nel quale voi potete inserire questa vostra visione della concentrazione del potere su una sola persona, allora cercate di farlo al fine di alterare l'equilibrio dei poteri e l'efficienza democratica delle nostre istituzioni. Queste sono le ragioni per cui noi non potremo che votare contro la

che ringrazio sentitamente per aver espresso la sua soddisfazione e aver detto testualmente che è una bella pagina, di cui essere tutti orgogliosi, l'inserimento in questo disegno di legge di conversione della norma per il voto agli studenti fuori sede. La ringrazio due volte, senatore Meloni, perché, avendo ascoltato anche l'intervento del suo collega di partito, senatore Parrini, mi era sembrato di aver colto da parte del suo partito un ben altro atteggiamento e un ben altro giudizio; al punto che il senatore Parrini si è addirittura spinto a dire che noi avremmo inserito questa norma nel disegno di legge in esame, perché non abbiamo avuto voglia - testualmente di concludere l'esame del provvedimento avente lo stesso oggetto che ci era arrivato dalla Camera, quando invece tutti i colleghi componenti della 1a Commissione hanno potuto constatare di persona quanto questo Presidente si sia impegnato, anche personalmente, affinché sull'argomento si potesse arrivare almeno a un primo passo. È un primo passo importante, di cui credo che sia giusto che quest'Assemblea, dopo che lo ha fatto la Commissione, si intesti tutta insieme un passo avanti nella democrazia, nel consentire a tutti coloro che non sono in grado di farlo - non perché non vogliano farlo, ma perché sono obbligati a rimanere lontano da casa - di esercitare il diritto-dovere di voto. Ringrazio in questo senso la senatrice Spinelli e il senatore De Priamo per avere sottolineato questo aspetto. Penso di poter dire su questo punto, collega Meloni, senza volermi attribuire eccessivi meriti, che se il sottoscritto non avesse sollecitato in modo pesante i propri colleghi di maggioranza e il Governo a fare almeno questo primo passo, probabilmente oggi non saremmo nemmeno nelle condizioni di esprimere la soddisfazione che lei ha espresso e per la quale, ancora una volta, la ringrazio. Abbiamo ascoltato tutti in audizione i tecnici esprimerci una serie molto rilevante e complicata di problemi, per superare i quali ancora c'è bisogno di tempo. Consentire almeno agli studenti di poter esprimere il loro voto

soluzione. D'altronde, cari colleghi, se fosse stato così facile dare il voto ai fuori sede, la domanda

Sul tema del ballottaggio eventuale 40 per cento, introdotto per la prima volta in Assemblea da un emendamento dei colleghi della Lega, nel merito sono d'accordo. Non credo sia un attentato alla Costituzione. È già in vigore in Sicilia, è stato approvato nei giorni scorsi in Friuli-Venezia Giulia. Evidentemente è un sistema che ha la sua dignità come altri.

sull'opportunità di inserirlo in questa sede, in questo momento; certamente un intervento così rilevante, che cambia così profondamente le regole che sono in vigore nel 70 o 75 per cento dei Comuni italiani, in tutti tranne che la Sicilia e il Friuli-Venezia Giulia, avrebbe avuto bisogno di un maggior approfondimento e di un maggior confronto. Pur essendo io personalmente d'accordo con questa norma norma - come tutti sanno, ormai è sempre più frequente il caso di un sindaco che vince al ballottaggio con meno voti di quanti ne ha presi il suo avversario al primo turno - sono anche d'accordo con quanti sottolineano

che ledono la dignità del nostro lavoro, perché - secondo me - definire vergognosa la presentazione di un emendamento non ha nulla a che fare con il legittimo esercizio dell'attività che tutti quanti stiamo svolgendo. *(Applausi)*.

i colleghi che sono intervenuti e i senatori tutti. È stato un lavoro proficuo che certamente ha visto visioni differenti e spesso non trovare una comune intesa, una comune visione. Sarà comunque un lavoro proficuo anche rispetto a quella che è stata la volontà di estrapolare tanti emendamenti che non hanno trovato accoglimento, non soltanto in alcuni casi per aspetti puramente tecnici, ma anche

dal punto di vista legislativo, come il TUEL, che ha oltre trenta anni di vita e che oggi necessita di una revisione rispetto ai grandi temi degli enti locali. degli enti locali. Ho ascoltato molti interventi, alcuni interessanti e alcuni - come sicuramente ha stigmatizzato molto bene il presidente Balboni

Tra queste, ovviamente si è parlato delle proposte emendative riguardanti gli interventi di modifica a regime nel Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, compresa la legge Delrio sulle Province e la normativa statale concernente i principi fondamentali in materia di elezione del Presidente, degli organi elettivi delle Regioni e della legge elettorale europea.

e a me, onestamente, interessa sottolinearlo nuovamente in questa sede. È un lavoro, predisposto rispetto al Testo unico degli enti locali, che è in dirittura d'arrivo, che troverà un giusto confronto con tutti i Gruppi politici, con tutte le parti politiche il Parlamento, soprattutto attraverso gli incontri che si sono riaperti con gli attori principali. Penso ai Ministeri coinvolti, che non sono soltanto

di valutare diverse proposte da voi fatte, non soltanto dalle opposizioni, ma anche dalla stessa maggioranza, in sede di discussione di quel disegno di legge delega, anziché intervenire con misure scollegate, a macchia di leopardo, nell'ambito di un provvedimento finalizzato a disciplinare le consultazioni elettorali per l'anno 2024. La rimozione del limite del mandato, di cui ho sentito parlare dal collega Parrini, che riguarda i sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti e la possibilità per il terzo mandato per i Comuni che arrivano al tetto dei 15.000 abitanti, è un intervento che il Viminale ha adottato non ascoltando soltanto la voce dei tanti singoli amministratori. Voglio qui ricordare anche le sollecitazioni che sono arrivate

da parlamentare della Repubblica, che mi è sembrata un po' forzata rispetto a una sentenza che riguarda una legge della Regione sarda. Per quanto mi riguarda, essa potrebbe anche sancire quell'uniformità sul territorio nazionale del limite ai mandati dei sindaci, che giudica in qualche modo quella legge sarda. Soprattutto, credo il principio del limite dei mandati possa essere in qualche modo bilanciato attraverso la possibilità, sancita anche dalla Cassazione, quale temperamento di sistema rispetto all'introduzione dell'elezione diretta e della loro elezione; quindi, con quel bilanciamento rispetto al principio di eguaglianza all'accesso alle cariche elettive. Per quanto riguarda la situazione ben diversa delle Regioni, che hanno un potere, non soltanto di amministrare, ma anche un potere legislativo, sul tema del terzo mandato, voglio chiarire e lo voglio fare da rappresentante di questo Governo. Non c'è alcuno scontro nella maggioranza, ma c'è un dibattito sereno; un dibattito sul sul piano parlamentare su un tema su cui non c'era stato accordo precedente rispetto ai tanti punti d'intesa del programma della coalizione, ma che vedrà, in altre sedi, sicuramente la giusta attenzione e il giusto approfondimento. La nostra posizione è che la proposta debba essere valutata all'interno sempre della revisione del Testo unico degli enti locali, in modo da poter essere approfondita in tutte le sue sfaccettature. Ho sentito parlare anche di un disallineamento per quanto riguarda chi vuole rimuovere un limite ingiustificato verso chi ricopre ruoli di responsabilità all'interno della Regione per eventuali candidature. candidature. Per quanto riguarda la parte dei Comuni e delle Province, sempre per quel filo conduttore che riguardava la revisione del TUEL, abbiamo rinviato questo ad un successivo approfondimento, rispetto al parere che è stato dato

in una effettiva posizione di conflitto è fortemente limitato. Questo chiarisce quel disallineamento che più volte avete sollecitato sia in sede di Commissione e oggi in Aula per quanto riguarda la disciplina applicata per i consiglieri provinciali e comunali. Il tema della retroattività della norma - lo vogliamo ribadire anche in Aula - non si pone. È sufficiente ricordare come le diverse sentenze da parte della Corte costituzionale abbiano osservato che il principio di non retroattività della legge va inteso come fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo per quanto riguarda la materia penale (articolo 25 della Costituzione), ma anche in altri settori dell'ordinamento. Ciò vale ancora di più quando l'intervento legislativo incide su giudizi ancora in corso, in ossequio dei princìpi costituzionali relativi al rapporto tra il legislatore Arriviamo ad un punto che avete sollevato. La raccolta delle firme per le elezioni europee europee è già iniziata e i partiti hanno termini più stretti per raccogliere le firme nel numero previsto per legge. Ciò ha visto da parte della maggioranza la volontà di questo taglio di oltre il 50 per quella volontà di chi sempre e comunque rispetta credo la politica e che ha trovato accoglimento da parte del Ministero dell'interno. Abbiamo parlato più volte - lo hanno detto molti colleghi anche della maggioranza, ma ho visto oggi arrivare altri testi a firma dei Gruppi di opposizione - anche della responsabilità dei sindaci e degli amministratori. Anche quella ovviamente è una partita fondamentale nella nella futura revisione del TUEL che troverà i giusti approfondimenti, come del resto ha trovato l'accoglimento un ordine del giorno della Commissione.

del voto a distanza per quanto riguarda le europee per gli studenti fuorisede. Esso è in linea con gli impegni assunti dal Governo anche con i comitati degli studenti - questo lo voglio ribadire - diretti a favorire la giusta partecipazione alla vita democratica attraverso soluzioni tecniche. Ho sentito molte volte ripetere in Commissione, quasi come un mantra, che il Governo ha cambiato idea, che il ministro Piantedosi la pensava in un modo e quant'altro.

l'idea era quella di una buona legge, di una sperimentazione con voto valido che desse la possibilità agli studenti fuori Regione di poter votare e di mettere alla prova un sistema in termini di sicurezza, di trasparenza e di segretezza del voto. Questo

mandato, in 1a Commissione alla Camera parlare di tante promesse fatte e mai mantenute. Oggi è arrivato il momento di mantenere le promesse. Lo abbiamo fatto attraverso anche una sperimentazione alla quale abbiamo invitato i comitati. Si tratta della sperimentazione del voto digitale per gli italiani all'estero e oggi vedo parecchi di questi emendamenti con delle problematiche rispetto ai pareri che servivano del MEF e del MAECI. Questo ovviamente ha dato un riscontro positivo rispetto al voto, poiché c'è stato un aumento del 20 per cento; ma vi sono stati oltre 9.000 tentativi di hackeraggio e di intrusione che non sono riconducibili a gruppi, ma che certamente

che possano consentire l'emissione della famosa tessera elettorale, che ognuno potrà scaricare o che potrà visionare rispetto alla propria posizione da elettore attraverso

Credo che si sia fatto tanto, tanto ancora c'è da fare, ma certamente sento di poter dire che questo Governo a guida Meloni, di cui mi onoro ovviamente di far parte, gli impegni assunti li ha mantenuti. Qualcuno diceva che solo le persone assurde non cambiano le proprie opinioni; noi le opinioni le cambiamo rispetto ad un percorso di serietà, di leggi rispetto alle quali troppe volte si è dovuti tornare indietro con problemi molto difficili da risolvere. Noi auspichiamo di lasciare traccia, ma soprattutto di fare piccoli passi, che però possano rimanere nella storia del buon Governo.

Gli italiani residenti in uno Stato membro possono optare di votare per il candidato locale oppure votare un candidato italiano nel seggio aperto presso i nostri consolati. Questa legge interessa 2.095.000 italiani, solo una parte, quindi, dei circa sei milioni di italiani residenti all'estero e iscritti nell'anagrafe AIRE. Si tratta praticamente della seconda Regione italiana per numero di residenti. Gli italiani iscritti nei Paesi europei che non fanno parte dell'Unione non hanno la possibilità di votare, a meno che non tornino in Italia a spese proprie. La stessa cosa si applica per gli italiani iscritti all'AIRE che vivono nei Paesi al di fuori della Comunità In totale, dunque, questi italiani sono più di 2,6 milioni e costituiscono più della metà degli italiani residenti all'estero. Ebbene, questi italiani possono votare soltanto se ritornano nel Paese d'origine a proprie spese. Una limitazione che, di fatto, impedisce di esercitare il loro diritto di voto e in ogni caso lo renderebbe molto oneroso. Molti di questi italiani hanno legami molto forti con l'Italia, molto spesso gli italiani si recano all'estero per un paio di anni e poi ritornano, molti di questi italiani vivono in Paesi come il Regno Unito (450.000 italiani) o la Svizzera (600.000 italiani) che hanno con la Comunità europea dei Trattati molto stretti, con libero scambio di merci e di persone e quindi sicuramente il destino della Comunità europea ha impatto sugli italiani che vivono in questi Paesi. Il Parlamento europeo sarà chiamato ad affrontare temi fondamentali, fra i quali il processo decisionale a maggioranza, la transizione energetica, la ricostruzione dell'Ucraina (che - ricordo a tutti quanti - è stimata in tre trilioni, quindi nessuno dei Paesi membri della Comunità europea sarà a credito); sarà chiamato a legiferare sulla difesa comune e sulla struttura del debito comune. Dopo questa legislatura, l'Europa sarà un'altra cosa e gli italiani che vivono al di fuori dei Paesi della Comunità europea ne subiranno direttamente o indirettamente le conseguenze senza aver partecipato al processo decisionale. I Paesi con cui amiamo confrontarci, tra cui la Francia, la Germania, la Spagna, consentono ai loro cittadini residenti al di fuori degli Stati dell'Unione di votare e questa è una differenza sulla quale dobbiamo riflettere. il fatto che i nostri cittadini vengano privati della possibilità di votare è inaccettabile anche per il fatto che le direttive europee offrono agli Stati membri la possibilità di legiferare e permettere agli italiani residenti in Stati non membri L'approvazione di questa proposta restituirebbe quindi la cittadinanza politica a milioni di italiani e restituirebbe milioni di italiani all'Italia.

un convegno molto interessante, al quale hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Meloni e il presidente La Russa. Cito le parole del presidente Pera, che peraltro condivido, a proposito di Patria: consapevolezza delle esperienze comuni per costituire una dimensione fisica e materiale che si è disposti a fare insieme e condividere. Mi ha inoltre colpito un'altra riflessione, sempre del presidente Pera: la Patria non è un'astrazione, ma la costruiamo e la difendiamo giorno per giorno con azioni che ci accomunano.

di votare a favore di questo emendamento; se votano contro, desidero che i sei milioni di italiani residenti all'estero ascoltino chiaro e forte il no di questo Governo di patrioti. *(Applausi)*.

motivo dobbiamo opporci a tale idea, se esiste un bravo amministratore che ha dimostrato capacità, che non necessariamente riguarda la parte politica da me sostenuta. infatti riconoscere, nel massimo della onestà intellettuale, che ci sono amministratori regionali, Presidenti di Regione che non hanno le mie idee politiche, ma che hanno fatto del bene alle loro comunità. Faccio per esempio riferimento a ciò che è avvenuto in Veneto. Ci sono Regioni che, probabilmente, dal tema della continuità amministrativa potrebbero avere dei benefici in termini, per esempio, di risoluzione dei problemi relativi al dissesto idrogeologico, alla sanità e alle politiche per lo sviluppo di quel territorio. Non si capisce quindi per quale ragione

un po' più concretezza, un po' più orgoglio, perché non si è nemmeno stati in grado di difendere i propri amministratori. Allora delle due l'una: o voi pensate che quegli amministratori e Presidenti di Regione che si battono per avere l'allungamento del mandato non siano davvero capaci, o altrimenti non si giustifica il vostro atteggiamento. Vengo poi agli amici colleghi del Partito Democratico, quali un sussulto di dignità non guasterebbe. Non devo essere io a dirvi che ci sono Presidenti di Regione, per esempio

come il presidente De Luca, che hanno gridato in tutti i modi agli esponenti del Partito Democratico che non è con la tagliola dei tre mandati che si elimina un problema politico grosso come una casa, sia a destra che a sinistra, che vi ritroverete sul campo. Allora perché non facciamo scegliere gli elettori se pensano che Bonaccini sia bravo oppure no, De Luca sia bravo oppure no, Zaia sia bravo oppure no? Perché invece decidiamo che tutto ciò debba essere risolto da una platea di colleghi compresa la sottoscritta (così evito le critiche e faccio autocritica immediata)? È vero, hanno tutta la legittimità sulla base della democrazia rappresentativa, ma in fondo stavano dentro liste bloccate, mentre in questo caso stiamo togliendo la possibilità agli elettori di giudicare, con il loro voto diretto, se i Presidenti sono all'altezza oppure no. Allora, l'ultimo appello al buon senso, alla dignità ed anche al rispetto del buon lavoro

TOSATO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare il Governo per non aver espresso un parere contrario rispetto a questo emendamento, a dimostrazione che non c'è una posizione contraria del Governo, ma lascia al Parlamento legittimamente la possibilità di avviare un dibattito su questo argomento e far esprimere liberamente ad ogni parlamentare il proprio voto senza il vincolo di votare contro l'Esecutivo. Noi difendiamo con orgoglio l'emendamento 1.0.6, a differenza di quanto è stato affermato precedentemente da un esponente dell'opposizione, perché riteniamo di interpretare non solo la posizione della Conferenza delle Regioni, che rappresenta tutti i partiti politici

i partiti politici a stabilire se un rappresentante del popolo che ha governato bene, che li ha rappresentati bene, che ha ancora l'energia e il consenso dei cittadini per poter proseguire il proprio mandato, debba essere messo fuori gioco a tavolino a causa di una decisione normativa che sicuramente non rispecchia la volontà del popolo e dei cittadini. Questa è la nostra posizione. Noi crediamo profondamente nel concetto di democrazia. Crediamo che il potere di scelta spetti al popolo e non riteniamo che siano quindi i partiti a poter stabilire se un governatore o un sindaco vada o meno ricandidato. Con queste scelte, nel limitare questa possibilità, non limitiamo esclusivamente il diritto di un rappresentante dei cittadini di ricandidarsi, noi impediamo l'esercizio libero del voto e, in democrazia, il primo potere potere che appartiene al popolo è quello di poter votare chi vuole, chi ritiene lo rappresenti meglio. *(Applausi)*. È questo il motivo per cui abbiamo presentato questo emendamento e lo difendiamo. Sappiamo di interpretare più di altri partiti la volontà di fasce fasce elettorali di tante Regioni, trasversali in alcuni casi, che vorrebbero avere la possibilità di esprimersi nuovamente sulla ricandidatura di un governatore che ha esercitato bene il proprio ruolo, che li ha rappresentati bene e che potrà farlo anche in futuro. Per questi motivi noi teniamo la posizione, l'abbiamo fatto in Commissione, lo facciamo in Aula e lo faremo anche prossimamente perché il dibattito per quanto ci riguarda non è chiuso in questa occasione *(Applausi)*, a fronte del parere che è stato appena espresso dal Governo, nella convinzione anche se andremo palesemente sotto in questa votazione, stiamo interpretando nel modo più corretto la volontà dei cittadini e degli elettori. *(Applausi)*. Signor Presidente, a beneficio di tutti e per estrema chiarezza, qui si sta votando il famoso emendamento che ha tenuto con il fiato sospeso la Commissione affari costituzionali nonché parte dell'opinione pubblica, quella che non aveva

il collega Tosato che stimo, Presidente, attraverso di lei, ha detto che la Conferenza Stato-Regioni è d'accordo, cioè che i diretti interessati sono d'accordo con l'innalzamento del limite dal secondo al terzo mandato per i Presidenti di Regione. A Roma abbiamo un bellissimo modo di dire: «Oste, il vino com'è?».

qui si usa la democrazia e la possibilità del corpo elettorale di scegliere da chi essere amministrato per violare un principio invece sacrosanto. Avete la

non dovrete convincere soltanto la maggioranza di questa Aula, ma la Corte costituzionale. Mi dispiace contraddire infatti la sottosegretaria Ferro quando dice che la sentenza n. 60 del 2023 non è pertinente rispetto al tema dei mandati dei sindaci. Io la estendo anche ai mandati dei Presidenti di Regione. Tale sentenza infatti parla di un principio, come sempre fa la Corte costituzionale che parla di principi generali di democrazia, non di casi particolari. dice che è comunemente riconosciuto che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci - e io aggiungo anche dei Presidenti di Regione - è stato pensato quale temperamento di sistema.

Corte di Cassazione del 2021, sentenze del 2012, un'altra sentenza del 2007, un'altra ancora del 2002, sempre in quella stessa direzione: in effetti, la previsione di un tale limite si presenta quale punto di equilibrio punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'Esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona. Tale sistema può produrre effetti negativi anche sulla *par condicio* delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione. È evidente che questo emendamento sia da respingere. Purtroppo, non sarà possibile respingere l'innalzamento del tetto ai mandati dei sindaci per i Comuni fino a 15.000 abitanti e l'eliminazione di qualunque tetto per i sindaci di Comuni sotto i 5.000, perché quello è direttamente nel testo di questo provvedimento che ci accingiamo a votare. Ma noi denunciamo comunque

noi riteniamo assolutamente legittima questa discussione, che non è una discussione teologica. Sul numero dei mandati e sull'elezione diretta, c'è un dibattito aperto. Ad esempio, nella discussione riguardante il premierato

questa normativa di riforma della Costituzione. Anche in tale occasione sono state fatte discussioni sulla concentrazione di potere, sul fatto che un *premier* debba avere un orizzonte temporale limitato. Il Gruppo di Forza Italia, senza farne motivo di lite o di discussione, si è attestato sulla posizione che, per le Regioni e i Comuni sopra i 15.000 abitanti, si ritiene logico mantenere il sistema del doppio mandato. Sulle Regioni c'è anche un intreccio con statuti e normative varie e quindi immagino che vi sarà una discussione che proseguirà anche in punta di diritto. Quanto a quelli che cercano di fare discussioni politiche, credo che nessuno le possa fare. C'è chi è legato a un'idea del doppio mandato in assoluto, anche in altri ambiti, per propria scelta, che a volte viene rispettata e a volte no.

del testo degli enti locali, ognuno potrà porre legittimamente la questione. Io non mi scandalizzo se i colleghi della Lega sostengono una tesi e noi abbiamo una opinione diversa, né la maggioranza di Governo è nata per fondarsi su quanti mandali debbano fare i Presidenti di Regione. Sono altri i temi che danno l'identità di un Governo: il meccanismo delle elezioni

che determinano limiti temporali. La domanda ad un concorso si presenta entro una certa data. Quindi, noi riteniamo che sul numero dei mandati sia lecito esprimere le proprie opinioni. La nostra è conforme a ciò che è vigente e a quanto il decreto introduce: liberare i mandati nei comuni sotto i 5.000 abitanti. In alcune Regioni, vi sono centinaia di Comuni di montagna, piccoli e piccolissimi, dove trovare il sindaco, praticamente gratuitamente, è impossibile. L'Italia ha 8.000 Comuni. Non dobbiamo guardare solo alla situazione della grande città. È diverso fare il sindaco di una grande metropoli, con un potere politico rilevante, e cercare una persona che, nel Comune di 500 abitanti, si occupi del bene comune, di avere l'elettricità o l'acqua. A volte, trovarne uno e poi trovarne un altro è complicato. Quindi, a nostro avviso, il decreto risponde a questi criteri. Poi questa discussione prosegue, come tante altre discussioni proseguono e non dividono assolutamente schieramenti perché - ripeto - sarà successo anche a voi, visto che ognuno ha rapporti con il territorio: qualcuno per una certa condizione vuole la legge che possa fargli proseguire i mandati, un altro invece no. Quindi non esiste una posizione ideologica su tale questione. La nostra posizione è conforme a quello che il decreto-legge dice, rispettiamo le posizioni diverse e non troviamo assolutamente assolutamente scandaloso se il Parlamento si esprime. Forse bene ha fatto il Governo a rimettere all'Assemblea la questione, perché non è un tema su cui il patto di Governo ha trovato una sua Il Governo governa indipendentemente da come discutiamo noi nel libero Parlamento su una questione come quella in esame. La nostra posizione contro questo emendamento l'ho voluta esprimere per evitare equivoci e interpretazioni. La si può esprimere tranquillamente in un Parlamento davanti alla pubblica opinione, rimanendo saldamente coesi in un'azione di Governo

Signora Presidente, non si tratta di tutelare o di violare e mortificare il diritto di elettorato attivo dei cittadini, o di limitare o violare l'altrettanto fondamentale diritto di elettorato passivo dei candidati, magari amministratori in carica. Si tratta semplicemente di tenere in equilibrio il sistema. Si tratta semplicemente di rispettare fondamentalissimi principi che la Corte costituzionale in più occasioni ha ricordato. chi prima ha paventato il rischio che respingendo questo emendamento non si garantisca ai cittadini la libertà di scegliere l'amministratore che preferiscono, mi limito a rispondere suggerendo di leggere la sentenza che è stata prima richiamata, la n. 63 del 2023, ma anche tutta la precedente giurisprudenza, che ha ricordato come un cardine del nostro ordinamento costituzionale e di tutti gli ordinamenti costituzionali pluralistici stia nel definire limiti equilibrati alla concentrazione del potere. Peraltro, onorevoli colleghi, l'emendamento che stiamo per votare rimuove qualsiasi limite, perché c'è un secondo comma che forse né l'onorevole Tosato né l'onorevole Paita hanno voluto illustrare, ma che merita di essere letto. Questo secondo comma infatti dice

provvedimento. Questo secondo emendamento affronta un tema che già è stato oggetto di controversie e di discussioni perché ha consentito in alcune Regioni, come ad esempio il Veneto, di di violare la norma oggi vigente. Infatti abbiamo nella Regione Veneto un Presidente che è al terzo mandato. I cittadini potrebbero chiedersi: ma non è in vigore una regola che stabilisce il tetto dei due mandati? No, è in vigore anche un Presidente che è al terzo mandato, perché si è avvalso di un'interpretazione, che non è stata al momento portata all'attenzione della Corte, secondo la quale l'operatività del limite dipenderebbe dal recepimento

a me questo non è chiarissimo. In ogni caso l'emendamento presentato dal senatore Tosato e l'emendamento di Italia Viva sono chiarissimi e dicono che qualsiasi limite opererà solo se e quando la Regione lo recepirà. Che questa sia una soluzione di equilibrio e che tiene insieme il fondamentale diritto dei cittadini di poter scegliere i loro amministratori e l'altrettanto fondamentale diritto degli amministratori che hanno ben amministrato di potersi ripresentare al corpo elettorale credo che sia quantomeno lecito dubitarlo. *(Applausi)*. Per questo motivo noi voteremo contro. nuova finestra"). Salutiamo in tribuna gli studenti e i docenti del Liceo scientifico «Enrico Fermi» di Catanzaro che assistono ai nostri lavori. Benvenuti.

vorrei motivare il voto contrario mio e del mio Gruppo su questo emendamento, che ha una sua finalità intelligente, che sarebbe anche condivisibile, quella cioè di far votare

dovrebbe avere la possibilità di esercitare il diritto di voto in qualunque modo possibile. Ora, la questione si pone in termini diversi a seconda delle elezioni in cui si vota. Qui, in particolare, ci occupiamo di elezioni europee

e quindi si esprimerà votando in quella circoscrizione. La cosa è differente, evidentemente, quando si tratta di Paesi extraeuropei, pensando di andare anche più lontano; pensiamo ad esempio a un argentino che voglia votare. Ovviamente per tutti coloro che sono fuori dai Paesi dell'Unione europea l'unico principio realizzabile ad oggi è quello per cui si vota soltanto tornando in Italia e questo evidentemente è sostanzialmente impossibile, salvo per qualcuno che venga a fare le vacanze La questione però si pone in altri termini, non vi è in tutta evidenza la possibilità di realizzare questo, almeno finché si vota alle elezioni europee. Alle elezioni politiche noi votiamo in un altro modo,

italiani all'estero - che eleggono i loro parlamentari votando nella cosiddetta ripartizione estero, che a sua volta poi è divisa in altre micro-circoscrizioni. Si tratta, quindi, di voto espresso all'estero e con candidati residenti all'estero. In realtà, si è variata anche questa cosa, perché possono essere eletti anche i residenti in Italia. Ora io vi pongo la questione in termini di riflessione al Parlamento. Questo era un fatto moderno e molto positivo che altri ci hanno invidiato, perché abbiamo dato la possibilità di votare a quelli che non avevano votato per decenni. Tuttavia, si è potuto verificare che il voto che noi pratichiamo (costosissimo per lo Stato) è quello per corrispondenza, che consiste nell'invio da parte delle ambasciate e dei consolati di plichi contenenti una scheda da restituire votata ai consolati stessi.

cosa è accaduto anche nelle ultime elezioni: compravendita dei voti, stampa di schede, questioni che investono la trasparenza, la segretezza e la personalità del voto. La riflessione che io vi propongo deriva da questo: se noi lo vogliamo per il prossimo turno elettorale sia delle politiche sia delle prossime elezioni europee, cominciamo a porci il problema di verificare come sia possibile realizzare un sistema elettorale che garantisca la segretezza e la personalità del voto, che ci garantisca dai brogli che - come sappiamo tutti - avvengono Personalmente, ritengo che, puntando sull'innovazione e sulla digitalizzazione, di cui tanto si parla anche nella pubblica amministrazione, la strada da seguire è quella, solo per l'estero e non per l'Italia - in Italia dove dovremmo comunque continuare a votare con le schede con la matita, anche perché di quello rimarrà sempre riscontro della identificazione digitale di ogni cittadino all'estero. Con l'identità digitale si possono fare tante cose - ognuno di noi fa operazioni bancarie, eccetera - e quindi saremmo protetti anche se volessimo lanciare questa ipotesi. Far votare tutti i 6 milioni di cittadini italiani residenti all'estero con procedura elettronica

dobbiamo riflettere anche a tutela di tutti. Io sono per il riconoscimento e da patriota vorrei trovare tanti italiani anche fuori dall'Italia. Penso che la Nazione vive anche fuori dall'Italia, ma è italiano chi si sente italiano, chi parla italiano, chi condivide i valori costituzionali, non chi ricostruisce a distanza di anni un presunto legame, con il quale vuole rivendicare una cittadinanza che però non è sentita e praticata. Ho allargato molto il campo, me ne scuso, ma ho motivato il nostro no e ho anche detto qualcosa in più.

opportunità politica ed opportunismo. In realtà, il testo afferma che è fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Tra l'altro, sessanta giorni possono essere benissimo superati. Non c'è questa urgenza. A volte la burocrazia amministrativa porta anche tempi più lunghi. Quindi, invito a votare, con il MoVimento 5 Stelle, a favore di questo emendamento. *(Applausi)*.

Signor Presidente, noi abbiamo fortemente condiviso il lavoro svolto all'interno della Commissione. Ringraziamo anche il presidente Balboni per la sensibilità dimostrata rispetto ad una battaglia che per Azione è davvero importante e rappresenta un diritto per coloro che sono fuori sede, studenti ma anche lavoratori o prestanti cura, di poter votare dove svolgono la loro attività. In Commissione è stato fatto un passo avanti per la votazione degli studenti fuori sede (poco meno di 500.000 persone), ma rimangono ancora esclusi i lavoratori fuori sede e i prestanti cura. Noi attraverso questo emendamento chiediamo che quella facoltà, che è un diritto e non una gentile concessione, venga riconosciuta riconosciuta anche ai lavoratori e a coloro che prestano cura lontano dal luogo di residenza. Auguriamo che ci possa essere su questo emendamento un voto favorevole. *(Applausi)*. Signora Presidente, nel corso dei lavori della 1a Commissione c'è stata un'importante modifica a questo testo normativo, anche grazie a un intervento da parte del presidente Balboni che ha condiviso il lavoro che abbiamo portato avanti. Quindi, si è riusciti a inserire nel testo il voto per gli studenti fuori sede. Sono rimasti fuori però i lavoratori fuori sede e le persone che sono sottoposte a cure, che purtroppo devono addirittura recarsi fuori dal loro Comune Comune di residenza. Il tema dell'elettorato attivo è serio, delicato e soprattutto deve essere affrontato concretamente. Se poi noi ci lamentiamo dell'astensionismo e del disinteresse degli elettori, ma non diamo quelle misure e quegli strumenti per consentire il voto anche a chi, per ragioni di lavoro o di cura, si trova fuori dal suo domicilio, quindi fuori dal Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, è chiaro che allora facciamo discorsi contraddittori o ci doliamo di cose alle quali non vogliamo trovare rimedio.

né mi accontento di sentirmi dire che il libretto universitario consentirebbe più agevolmente l'identificazione dell'elettore rispetto a un'attestazione che dice che un elettore si trova fuori sede perché ha un contratto di lavoro o perché ricoverato, un foglio che attesta

talvolta esitanti, al limite forse della vigliaccheria. Quello che voglio ulteriormente evidenziare è che il tema è ancora più dolente e delicato per chi risiede nelle isole nelle isole e nei territori del Sud, che sono quelli che maggiormente si devono spostare per motivi di lavoro o per motivi di cura al di fuori del loro territorio. Allora poi abbiamo la speculazione dei voli, i cui prezzi vengono innalzati in corrispondenza di determinate occasioni, ivi comprese le tornate elettorali. È una cosa che ci possiamo dire serenamente, perché lo sappiamo. allarghiamo le braccia e diciamo che purtroppo i vettori commerciali fanno quello che vogliono e non possiamo influire sulla tematica dei prezzi dei voli. Alla fine poi che cosa succede? Succede che chi si è trasferito fuori sede perché deve lavorare ...non ha le risorse per affrontare il viaggio necessario a tornare a casa per esercitare il voto e semplicemente rinuncerà all'esercizio

che è importante aver recepito una mobilitazione dei fuori sede. Questo è il dato fondamentale. Parliamoci chiaro: noi siamo qui, vogliamo rappresentare i cittadini e abbiamo presentato questi emendamenti perché c'è un movimento di fuori sede, in particolare degli studenti, che reclama un diritto

Va bene il primo passo, ma il dato fondamentale è che grazie alla lotta e alla mobilitazione fuori sede il risultato è stato ottenuto, anche se solo parzialmente, e noi non stiamo facendo invece quello che dovremmo fare, ossia rispondere anche ai lavoratori e alle lavoratrici.

per noi questo emendamento è molto importante e fissa la posizione del nostro Gruppo per quanto riguarda l'argomento del voto sui fuori sede. Sostanzialmente la valutazione che che facciamo è quella che ha appena esposto il senatore Magni. Certamente non possiamo negare che con questo intervento si compie un passo avanti. Ad oggi nessuno che sia fuori sede può votare, alle prossime elezioni europee ci saranno degli studenti che potranno farlo. Il passo in avanti allora è indubbio. Però, nel mentre riconosciamo il passo avanti, non possiamo non sottolineare che si è persa un'occasione. infatti che si era deciso di intervenire, bisognava - a nostro avviso - farlo in maniera più ampia. Non comprendiamo perché si debba dare questo diritto soltanto agli studenti fuori sede e non anche ai lavoratori fuori sede. Non comprendiamo perché non si dia questo diritto a chi si trova lontano dal suo luogo di residenza per ragioni di cura. Non comprendiamo perché questo diritto lo si riconosca soltanto per le elezioni europee e soltanto per le elezioni del 2024. *(Applausi)*. Avremmo voluto che venisse riconosciuto per tutte le elezioni e non in relazione soltanto ad un turno elettorale, quello che abbiamo davanti.

Sarebbe bene che il Governo e la maggioranza assumessero l'impegno a fare questo passo più grande in tempi molto brevi. È infatti all'esame della Commissione un disegno di legge ordinario, che sarebbe il veicolo giusto per risolvere tutti i problemi, che potrebbe essere accelerato. potrebbe essere accelerato. Se venisse assunto un impegno in questo senso, noi potremmo avere un intervento sui fuori sede molto più ampio e organico, molto più spendibile con tutti quelli che si trovano in questa situazione, di quanto non sia questo piccolo, ma insufficiente passo in avanti.

e hanno scoperto che bisogna far votare tutti. Bisogna far votare quelli in ospedale, bisogna far votare i lavoratori, bisogna far votare chiunque, compresi gli studenti fuori sede. *(Applausi)*. immagino che le opposizioni abbiano sentito i pareri dei tecnici che sono venuti a relazionare, soprattutto alla Camera, nel corso delle audizioni su questi provvedimenti. sono ben consapevoli delle difficoltà nel far votare persone fuori dal proprio collegio elettorale. Si parla di far votare i lavoratori. Mi domando: ma se un lavoratore viene trasferito tre giorni prima delle elezioni,

Sanno benissimo, le opposizioni, quali sono i problemi tecnici sottostanti a questa scelta, che è una scelta che questo Governo ha fatto con coraggio: il coraggio che non ha avuto chi ci ha preceduto. È il coraggio di avviare una sperimentazione, perché tutte le novità che comportano delle difficoltà tecniche importanti e significative vanno evidentemente sperimentate e poi messe in campo. Questo Governo e questa maggioranza si sono assunti la responsabilità, per la prima volta, dopo anni e anni di discussione, di far votare gli studenti fuori sede. Avete sicuramente ragione nel dire che ciò rappresenta soltanto un primo passo. Qualcuno ha detto che si è persa un'occasione. Ebbene, dico a quel qualcuno che quell'occasione si è persa dieci anni fa. Probabilmente, se questo dibattito si fosse svolto in passato, oggi forse avremmo la possibilità di avviare la sperimentazione anche per altre categorie. Molto banalmente, dico che siamo orgogliosi e credo che gli studenti saranno orgogliosi di poter votare nella circoscrizione nella quale studiano. E siamo orgogliosi di farlo per primi. È davvero curioso che tutte le soluzioni ai problemi dell'Italia vi siano venute in mente il giorno dopo che avete perso le elezioni.

abbiamo preso appunti e abbiamo iniziato, con il voto degli studenti fuori sede, a fare quello che voi non siete stati in grado di fare. E domani gli studenti, grazie all'emendamento di Fratelli d'Italia, grazie al Governo, potranno votare anche in altre circoscrizioni. Presidente, io sono stato studente fuori sede io sono stato studente fuori sede proprio nella città di Bologna, che conosce bene il senatore Lisei. Io penso che un passaggio come quello che stiamo facendo oggi non meriti una polemica, perché è un passaggio del quale tutti quanti ci prendiamo i meriti, sia la maggioranza che l'opposizione. Per una volta vogliamo cogliere l'occasione non di fare sterili polemiche, ma di raccogliere l'idea che abbiamo fatto una cosa buona e giusta? Forse avremmo dovuta farla prima, forse l'avremmo dovuto fare meglio? Ma prendiamoci il merito, visto che stiamo parlando davanti a degli studenti, di avere fatto una cosa utile; non è una concessione, ma è un diritto sacrosanto. Smettiamola di fare sterili polemiche. Qui non si tratta di dire quello che avrebbe potuto fare il Governo di dieci o quindici anni fa. Arriviamo in ritardo? Bene, stiamo facendo una cosa giusta. Stop alle polemiche. Forse se cogliamo questo lato, saremo riusciti a fare un passaggio pieno estendendolo dagli studenti fuori sede anche ai lavoratori e anche a chi ha compiti di cura. Non ci siamo riusciti? Peccato, ma evitiamo di sporcare con sterili polemiche una conquista che, sinceramente, oggi sarebbe merito di tutti. *(Applausi)*.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, stiamo discutendo le disposizioni urgenti che riguardano anche la revisione delle anagrafi della popolazione residente residente e la determinazione della popolazione legale. Quindi, si tratta anche di riorganizzare i nostri seggi elettorali. Il mio emendamento interviene esattamente sulla formazione degli elenchi delle elettrici e degli elettori in due modi.

Quindi, si elimina la previsione che nelle indicazioni dei nomi delle donne ci sia anche quello del cognome del marito, cosa che è davvero senza senso ormai e discriminatoria, e l'attuale criterio di formazione che è la divisione dei sessi, che risale all'inizio e che è rimasto. Superarlo significherebbe anche avere un'organizzazione del seggio più moderna, in ordine alfabetico, e penso si eviterebbero anche quelle situazioni di disagio che affrontano le persone in transizione e che attendono i documenti rettificati.

Penso che una tale divisione nelle file tra uomini e donne nei seggi sia davvero il segno di qualcosa che non c'è più e che abbiamo superato: il corpo elettorale è uno e credo che anche questa divisione vada superata. *(Applausi)*.

non viene in mente nessun'altra cosa nel nostro Paese nella quale si mettono le donne da un lato e gli uomini dall'altro. Non si capisce veramente perché. Ora, superate le prime elezioni repubblicane, quelle meravigliosamente ritratte nel film di Paola Cortellesi, direi che quando andiamo a esercitare il nostro diritto di voto siamo tutti cittadini della Repubblica italiana senza distinzioni di sesso e di genere. Questa, quindi, mi sembra una norma di civiltà e di buonsenso e voglio ringraziare i colleghi che l'hanno presentata e chiedere loro il consenso per poter aggiungere la mia firma.

Osservo che questo è un altro dei tanti emendamenti che sono stati falcidiati dal famigerato articolo 81 della Costituzione. Si dice, cioè, che questo emendamento è oneroso e quindi si dà il parere negativo e non è possibile approvarlo. però, che ci dovrebbe essere la volontà da parte di questa maggioranza di intraprendere questa strada che sembra soltanto di buonsenso, perché davvero la segregazione di genere non è certamente degna di un Paese come l'Italia, perché è un retaggio che davvero non ha più alcun motivo di sussistere per tutti i motivi che sono stati già illustrati dai colleghi che

dell'emendamento in ordine del giorno e quindi in un impegno da parte della maggioranza ad andare in questa direzione. L'emendamento non è il mio, ma mi permetto di chiedere se questa strada il Governo l'abbia valutata, perché davvero ancora oggi vedere uomini e donne divisi nei seggi elettorali ha un po' il sapore di Paesi che la maggioranza non fa altro che citare per dimostrare che lì sì che c'è discriminazione di genere, mentre qui no. Magari valutate questa strada.

all'Assemblea le ragioni e l'opportunità del testo, lo dico con grande spirito di collaborazione al ministro Ciriani e alla sottosegretaria Ferro. Colleghi, con la proposta di stralcio al nostro esame, l'articolo 101 del Regolamento non casualmente ci consente di salvare il salvabile nei casi di decreti-legge pesantemente compromessi, nonostante i tentativi di arrampicata sugli specchi che hanno fatto il presidente Balboni e il collega Lisei,

in un anno in cui si vota anche per le elezioni europee. Avreste dovuto fare solo questo per rispetto del Parlamento, per rispetto del Paese, per rispetto delle amministrazioni locali, per rispetto dei cittadini italiani, del popolo italiano. Lo dico perché prima di tutto, sottosegretaria Ferro,

non dovete vergognarvi di dire che era un emendamento costruito semplicemente per un caso politico. A voi non interessava affrontare il nodo del terzo mandato; a voi interessava affrontare da quest'Aula

prima di tutto democrazia vuol dire fiducia del popolo nelle sue leggi e il popolo queste leggi deve sentirle proprie, come scaturite, per dirla alla Calamandrei,

emendativi venuti fuori da una parte della maggioranza, che devo dire ha imbarazzato la restante parte della maggioranza, sono venuti fuori chiaramente per interessi di parte pasticciati. Presidente Balboni, le vorrei ricordare che quando eravate all'opposizione, declinavate sistematicamente i verbi al futuro: parlavate di quello che avreste fatto, di come avreste cambiato il mondo e di come avreste rafforzato la democrazia. Appena siete arrivati al Governo, il verbo e le condizioni sono cambiati. Parlate di storia, parlate di passato; non siete degli storici, perché se foste degli storici saremmo molto preoccupati, perché fareste una revisione totale della storia e non ci andrebbe molto bene, e utilizzate sempre il condizionale e tanti «forse». signora Presidente, è legata al fatto che le disposizioni in oggetto tolgono il limite dei mandati per i sindaci nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

perché vorrei davvero una risposta dal Governo: le pare questo l'obiettivo del decreto-legge elezioni? Le pare questo il modo di intervenire su una norma che noi ci saremmo aspettati fosse discussa e affrontata dentro la riforma del Testo unico degli enti locali, perché lei così ci aveva detto, così come ci aveva prospettato l'ipotesi di intervenire sul riordino delle Province, così come ci aveva prospettato l'ipotesi di intervenire anche sul personale delle amministrazioni locali, così come ci avevate prospettato l'ipotesi di riordinare un sistema che ha bisogno di più Stato, non di meno Stato. Invece, cosa accade con un decreto che doveva fissare una data? Smontate il TUEL. Ecco perché la proposta di stralcio: era un tentativo di venirvi incontro e di dire chiamiamo un *time out,* presidente Romeo, evitiamo che la destra torni alla stagione infausta delle leggi *ad personam*. Invece ci siete ricascati; è più forte di voi, non ce la fate. Però avete preso in ostaggio le amministrazioni locali. Avete preso in ostaggio le amministrazioni regionali e oggi l'aggravante di questo dibattito surreale, perché è un dibattito davvero surreale, Collega Menia, ho apprezzato anche il tentativo che ha fatto prima per giustificare il «no» al voto ai residenti all'estero. Mi creda, è un dibattito surreale. *(Commenti)*. Non vi scaldate, ogni tanto sforzatevi di ascoltare le ragioni degli altri. Poi votate,

totale della parte della maggioranza che è chiaro che non condivide né la forzatura della Lega sul terzo mandato, né la forzatura della Lega sul ballottaggio (sì, perché poi ci torneremo, presidente Balboni, glielo garantisco) non si può certo non si può certo ritenere che le prerogative del Parlamento siano compresse. Noi ci siamo, ci saremo e vigileremo fino in fondo e faremo di tutto per non farvi smontare la Repubblica. Ve lo abbiamo detto più volte e continueremo a ricordarvelo sugli enti locali, sulle Regioni e sullo Stato con la pessima riforma del premierato. Per prassi costante ed univoca presso entrambi i rami del Parlamento non è proponibile lo stralcio di disposizioni di decreti-legge in quanto trattasi di norme comunque già vigenti, anche se in corso di conversione.

sulle scelte e i risultati della politica, che avvenga sulla base del voto degli elettori e non sulla base della decisione aprioristica di un amministratore. Tra l'altro, c'è tanta penuria di amministratori, perché è sempre più difficile, ci sono sempre più responsabilità,

a tutti gli amministratori un applauso per quello che spesso devono pagare in vicende di calamità naturali e di responsabilità individuali. Capisco che c'è una certa politica che magari non ha fatto neanche un giorno di amministrazione e non si è mai presa neanche un voto di preferenza, che tenda in qualche modo a tutelarsi. Io invece vengo da quella storia e e penso che tanti amministratori abbiano il diritto di essere non soltanto ascoltati e aiutati, ma anche tutelati. Sono tra quelli che si sono spesi contro il reato dell'abuso d'ufficio, per fare in modo che questi amministratori abbiano una dignità e una tutela. La proposta in esame, nel solco del ragionamento che facevo precedentemente, prevede la possibilità

più che scomodare Calamandrei, se fossi stato in lei avrei scomodato il Cencelli. Infatti la ragione per la quale il Partito Democratico si mette contro la volontà dei Presidenti di Regione, che danno lustro all'attività del Partito Democratico, e contro la volontà dei sindaci, è un tema che riguarda le correnti interne, non riguarda la bella politica o la difesa della Costituzione. Allora le do un consiglio: anziché rileggersi Calamandrei, si vada a rileggere i principi del Cencelli che secondo me sono quelli a cui lei si ispira.

ricco di appuntamenti. Si è trasformato invece in una sorta di teatro dell'orrore. Abbiamo assistito a psicodrammi inenarrabili. Questo dei mandati dei sindaci e dei presidenti di Regione è uno degli psicodrammi più grandi. Mi dispiace, non è banalizzabile e riconducibile semplicemente a correnti interne ad alcuni partiti: la questione è molto più profonda. Ed è anche volgare accusare di

Stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2024 li ho già letti a quest'Aula ed invito tutti gli esimi colleghi e colleghe a leggerla per proprio conto, perché vi sono affermati principi che sono pilastri del funzionamento della democrazia. Viene stabilito e viene ricordato, proprio al legislatore, cioè a noi, per quale motivo eliminare questi limiti non è consigliabile consigliabile e non ha a che fare con le correnti e non ha a che fare con l'avere avuto esperienza o meno di amministrazioni locali. Ha a che fare con l'accentramento del potere nelle mani di una sola persona per un lungo periodo e con potenziali rendite di posizione. *(Applausi)*. Peccato, però, come dicevo in precedenza, che la previsione dell'innalzamento del mandato dei sindaci per i Comuni fino a 15.000 abitanti e l'eliminazione del tetto di questo mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti è compreso nel testo. È *all inclusive*, è nel testo: prendere o lasciare. Quindi, cosa sta facendo la maggioranza? Sta già agendo contro la Corte costituzionale, ma intanto agirà a beneficio di alcune situazioni o di alcune persone. Perché poi sappiamo che la democrazia, purtroppo, è lenta e prima che la Corte costituzionale emani una nuova sentenza che dirà che questa previsione è incostituzionale, voi avrete sistemato alcuni affari e alcune persone: alla faccia della democrazia e del popolo italiano. Complimenti! Signora Presidente, premesso che abbiamo già spiegato le ragioni per cui siamo contrari a questa norma e per cui ne chiediamo la soppressione,

Comuni. Questo è il dato fondamentale: non c'è un potere disgiunto tra l'eletto a sindaco e il Consiglio comunale. Questo è il problema e rappresenta un *deficit* della democrazia. Non è colpa di questa maggioranza. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che, a mio avviso, bisognerebbe discutere di questo. Invece, facciamo finta di niente e intanto la gente partecipa sempre di meno. Va a votare, ormai, il 50 per cento degli aventi diritto. Come tutti sapete, perché è così, molto spesso le leggi elettorali sono indicate decidendo prima quali sono la maggioranze, forzando, da questo punto di vista, e eliminando l'espressione libera dei cittadini e delle cittadine. Questo dovremmo discutere. Un Parlamento dovrebbe riflettere su questo dato e cercare di dare una risposta risposta razionale. Io non ho la soluzione in tasca e non voglio fare il professore di turno. Dico solo che questo problema c'è e che nessuno lo ha affrontato, mentre invece c'è tutto un dibattito sulla campagna acquisti, che invece non ci interessa.

Presidente, vorrei illustrare il contenuto dei due emendamenti a mia prima firma che riproducono il testo di emendamenti che avevamo già depositato nel corso della discussione sul cosiddetto decreto-legge Nordio, quando si discuteva dell'abuso d'ufficio. tali emendamenti vennero dichiarati inammissibili e poi vennero trasformati in ordini del giorno, peraltro bocciati dalla maggioranza. Li introducemmo nella discussione di quel decreto-legge perché li ritenevamo e li riteniamo tuttora emendamenti che propongono una soluzione efficace ai problemi che sono stati lamentati dai sindaci da tanto tempo in ordine alle loro responsabilità e ai rischi di essere indagati anche per condotte di natura spesso bagatellare e che magari portano a lunghi procedimenti penali che poi si concludono con assoluzioni. Tali emendamenti intervengono, nel modo che hanno chiesto i sindaci di affrontare, sul Testo unico degli enti locali per definire meglio il ruolo e la responsabilità dei sindaci sotto il profilo politico e amministrativo, separando meglio la responsabilità politica da quella amministrativa. Sia la parte che riguarda il Testo unico degli enti locali, sia la parte che riguarda la responsabilità erariale dei sindaci noi pensiamo siano le soluzioni che riescono ad andare incontro alle preoccupazioni legittime dei sindaci rispetto ai rischi e alle responsabilità che corrono nella loro funzione. loro funzione. Lo si fa in maniera molto più efficace di quanto ha inteso fare la maggioranza con l'abolizione dell'abuso d'ufficio, che non è né efficace, né idonea a rispondere a quelle preoccupazioni. Non è efficace perché con l'abolizione dell'abuso d'ufficio si privano di tutela i cittadini italiani nei confronti degli abusi dell'intera pubblica amministrazione, quindi è un grave errore. Tale abolizione rischia inoltre di essere addirittura controproducente perché sappiamo

questa è la vera soluzione ai problemi che sono stati enunciati ed evocati più volte anche dai nostri sindaci. Questa è la vera soluzione, non l'abolizione dell'abuso d'ufficio, e ci auguriamo che la maggioranza voglia accogliere questi emendamenti che

Signor Presidente, la riformazione riguarda l'ultimo punto della premessa: occorre altresì meglio delimitare le ipotesi in cui il sindaco può essere chiamato a rispondere del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54. 54. L'impegno al Governo invece andrebbe riformulato nella seguente maniera: impegna il Governo a valutare, in sede di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, l'opportunità di meglio valutare le ipotesi di responsabilità del sindaco.

Questo emendamento, visto che ci sono Capoluoghi di Provincia che hanno meno di 15.000 abitanti, stabilisce una regola di buonsenso che mi pareva condivisa da tutti in Commissione, secondo la quale, nel caso dei Capoluoghi di Provincia, lo *status* prevale sul criterio demografico e quindi ai Capoluoghi di Provincia, qualunque sia la loro popolazione, si applica il sistema elettorale del doppio turno e il limite dei due mandati al massimo consecutivi.

Avevamo discusso della questione in Commissione e mi era parso di capire, anzi credo sia gli atti della Commissione che il Presidente la vedeva esattamente come la vedevamo noi. Adesso, se non ho capito male, il parere è contrario su questo emendamento, sorpreso da questo cambio di orientamento. Non è possibile forse innestare adesso un dialogo. Ma, se successivamente potessimo avere ragione di come mai tra la Commissione e l'Aula l'orientamento del relatore si è modificato, rimarremmo con un dubbio in meno e - secondo me - dando parere contrario a questa nostra proposta si fa un errore serio, proprio uno sbrego istituzionale.

che in questo momento, a due mesi dal voto, modificare sostanzialmente la norma sia magari non corretto. Ci vuole un po' più di tempo e, quindi, ci può stare. Per noi, però, era importante

se nessun candidato raggiunge il 40 per cento è quindi un elemento più logico e più giusto; invece, se ci sono candidati che superano il 40 per cento, chi prende un voto in più viene eletto direttamente sindaco. Tra l'altro, ho sentito fare un appello e rivolgo un invito ai colleghi: impariamo a esprimere le nostre opinioni sulla base delle nostre considerazioni politiche. rispetto al continuo appello alla Corte costituzionale e alla magistratura, Ricordiamoci che il ruolo di fare le leggi è attribuito al Parlamento. La Corte costituzionale deve intervenire per verificare se le leggi che facciamo sono conformi alla Costituzione; la magistratura deve intervenire per applicare le leggi; i tecnici devono fare i tecnici; gli scienziati facciano gli scienziati e i politici imparino a fare i politici. Continuare a sentir dire che la politica perde potere da parte di quelle persone che poi continuano sempre a rivolgersi ad altre istituzioni è un elemento che davvero non comprendiamo. Poi ognuno si prende le proprie responsabilità.

aiuta le aggregazioni e, quindi, sostanzialmente viene un po' incontro alla formazione del campo largo. Pertanto, non dovreste essere poi così arrabbiati su questo argomento.

l'invito al ritiro dell'emendamento e alla sua trasformazione in ordine del giorno. Colleghi, la questione non è nuova: fu posta in un precedente provvedimento da un emendamento del collega Paroli, neanche quella volta si votò su questo principio e il senatore Romeo ha riproposto la questione. Dopodiché io dico che apprezzo anche il fatto di aver posto il problema e di aver accolto l'invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, perché parliamo di una questione che ci riguarda tutti. Le regole elettorali ovviamente riguardano chi vince, chi perde e le garanzie di tutti; pertanto io sono contrario a interventi improvvisi che non siano oggetto di un confronto. Questa tematica però tornerà, perché è stata discussa in occasione di un precedente provvedimento ed emerge in questo dibattito. Noi sappiamo tutti che a volte al secondo turno - è stato detto, ma lo ribadisco dei sindaci vengono eletti prendendo meno voti - per la scarsa partecipazione, spesso in estate avanzata, con un fenomeno di astensionismo che tutti deprechiamo e che tuttavia c'è,

il vincitore ha bisogno di 36.000 voti e casomai al primo turno il perdente, su 100.000 elettori, aveva preso 40.000 voti. Anche questa, quindi, è un'alterazione della democrazia.

Ogni metodo è legittimo. Quindi, anche il metodo di non svolgere il ballottaggio, se una coalizione raggiunge una percentuale congrua, tipo il 40 per cento, è legittimo. Guardate che la Corte costituzionale ha emesso sentenze sulla legge elettorale nazionale per il Parlamento dicono che il premio di maggioranza va dato se si raggiunge una cifra congrua e tutti sappiamo che si ritiene il 40 e il 45 per cento una cifra congrua per dare un premio. Non è che uno col 25 per cento può avere la maggioranza del Parlamento. I temi sono paralleli: sono una valutazione delle quantità e della rappresentatività. Quindi, l'ordine del giorno vuol dire che questa è una direzione di marcia che noi intendiamo percorrere e questo emendamento tornerà e mi auguro che la maggioranza lo approverà. Se poi il Parlamento non l'approverà, ne prenderemo atto. E non è un'alterazione della democrazia, come dice qualcuno, qualche Presidente di qualche organizzazione. È lo stesso che vuole il terzo mandato per se stesso, non vuole l'abolizione del ballottaggio. Non siamo nella Repubblica del presidente dell'ANCI: siamo nella Repubblica italiana. Quindi, non decide lui per tutti *(Applausi)*; è un punto di vista il suo, ma i toni che ha avuto oggi sono impropri ed escludo altre polemiche col Presidente dell'ANCI, perché non è questa la sede, ma ce ne saranno. Sono entrato in una Commissione in cui mi occuperò del suo Comune. Detto questo, questo, bene l'ordine del giorno, ma in Sicilia da tempo c'è una legge che prevede l'attribuzione e il successo al 40 per cento al primo turno. Il ministro Ciriani ci potrebbe raccontare del dibattito in corso nel Friuli-Venezia Giulia. Non so se è stata approvata o se è in via di approvazione anche in questa Regione una legge che prevede la possibilità di vittoria al primo turno se si raggiunge il 40 per cento dei consensi. Quindi, benissimo. Il senatore Romeo, con saggezza, ha proposto un tema che il senatore Paroli aveva proposto. Io lo condivido, credo anche la maggioranza. Non vogliamo fare cose affrettate. Si vota tra qualche settimana, alcuni hanno presentato già le liste, ma la questione tornerà e la modifica sarà approvata. Questo emendamento, che poi probabilmente verrà trasformato in ordine del giorno, non è nuovo da parte della Lega. Non è nuovo da parte della maggioranza di centrodestra, ma ciò non toglie che è un vero e proprio *blitz*, un tentativo di cambiare le regole democratiche. Lo dico per due motivi, essenzialmente. Il primo: questo è un decreto per definire l'accorpamento delle elezioni europee e delle elezioni amministrative. Se si vuole modificare una legge che ha ben funzionato, si fa la riforma del Testo unico degli enti locali. Non si tocca con un decreto-legge. *(Applausi)*. Dove di andare a piegare le regole democratiche alle vostre convenienze? Lo dico anche perché nella passata legislatura, quando l'allora ministra Lamorgese lavorò sulla riforma del Testo unico degli enti locali, chiamò tutti i partiti, tutti i rappresentanti dei Gruppi. Quando si cambiano le regole del gioco, si parla con tutti i Gruppi politici. Non ve la fate in casa solo come maggioranza. Terza questione e chiudo. Attenzione a cambiare le regole pensando di poterle piegare ai propri interessi di vincere. Non ha portato fortuna in passato. Ricordo al capogruppo Gasparri che la situazione del premierato e della sentenza della Corte costituzionale è ben diversa dalla situazione dei Comuni, perché il premio di maggioranza dei Comuni è del 60 per cento. Si avrebbe una torsione dal 40 al 60 per cento di discuteremo. Il punto è che sulle regole democratiche non si scherza e su questi temi lasciamo stare le ironie sul campo largo o non campo largo, che meriterebbero ben altra attenzione. Lo dico perché su questi temi, che riguardano appunto le regole del gioco e le regole che definiscono le elezioni dei sindaci, non c'è da scherzare. Sulle regole del gioco dovremmo riconoscerci reciprocamente. Quindi, spero che anche al Ministero dell'interno, la sottosegretaria Ferro e il ministro Piantedosi, quando parlano di questi temi e quando parleranno della riforma del Testo unico degli enti locali, abbiano la bontà di aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti di tutti i Gruppi politici.

andati davvero in scena su questo decreto-legge, ma devo dire che si assiste anche ad una sorta di campionato di giramento della frittata. Il *blitz*, infatti, senatore Romeo e colleghi della Lega, non l'avete fatto alle forze di opposizione: lo avete fatto alle forze della maggioranza di cui siete parte. Questo emendamento lo avete presentato alla chetichella qui in Aula. In Commissione non era passato. Questo è un comportamento da opposizione e anche da opposizione di quarto ordine, non di una forza di maggioranza. Punto primo quindi il *blitz* lo avete fatto ai vostri alleati. è vero che quello di far passare l'abominio qui per cui si abolisce il ballottaggio per i sindaci e chi prende il 40 per cento, qualunque sia stata l'affluenza, ha vinto e non se ne parla più, con buona pace della democrazia e della partecipazione, che avevate già provato nella riforma delle Province. Non si sente più parlare di tale riforma; evidentemente si è immersa sott'acqua e non si sa più se riemergerà. grande clamore, si era detto che non era una cosa ammissibile da infilare così in un provvedimento che si occupava di altro e cosa avete capito? Avete capito che andava infilato nel decreto elettorale per individuare le finestre per andare alle elezioni nel 2024. Davvero non ci siamo, amici della Lega. Vi state comportando come una belva agonizzante, che non sa più chi colpire e quindi colpisce alla rinfusa. Io vi invito un attimo alla calma, perché davvero avete un comportamento sconclusionato, che non credo vi gioverà.

impedire al Parlamento di prendersi le proprie responsabilità, che possono essere quelle di bocciare o di promuovere degli emendamenti. Allora che il momento non sia quello migliore è testimoniato dal fatto che siamo d'accordo nel fatto di

Sottolineo altresì il fatto che qualcuno addirittura ha detto che certi emendamenti non dovevano essere portati in votazione perché erano addirittura inammissibili. Parliamo di elezioni comunali; era certo ammissibile, così come era ammissibile

che erano legati al decreto-legge. Senatore Bazoli, l'emendamento che riguarda disposizioni in materia di responsabilità politica amministrativa dei sindaci e dei Presidenti delle Province mi sembra molto più lontano dall'argomento elettorale. Questa misura non c'entra assolutamente nulla con l'argomento elettorale. Detto questo, il presidente Balboni e il presidente La Russa lo hanno entrambi dichiarato ammissibile e, come si dice, sono insindacabili sia l'inammissibilità sia l'ammissibilità. Noto che c'è stata un'ampia apertura ad accogliere come ammissibilità - beninteso - degli emendamenti. Io credo che stiamo facendo un lavoro ben fatto, stiamo migliorando delle norme - non torno sugli argomenti che abbiamo già affrontato prima - e lo stiamo facendo nei modi dovuti. Sono poi anch'io d'accordo che, se si tratta di fare delle norme

Signor Presidente, si propone di fare un'aggiunta all'articolo 5, comma 2. Dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo e dal comma 22 dell'articolo 1-*ter*». Con il comma 22 dell'articolo 1-*ter* abbiamo infatti deciso di coprire le spese per il voto degli studenti fuori sede, che ammontano a circa 600.000 euro.

come un provvedimento molto semplice, molto lineare, legato alle disposizioni organizzative delle elezioni, oppure può anche avere

Peccato che, come abbiamo potuto osservare anche nelle ultime due competizioni regionali, ormai al voto si reca

dei giocatori che provano a piegare le regole del gioco al proprio interesse, ma come dei giocatori che vogliono semplicemente un gioco leale e soprattutto un rafforzamento della democrazia, che oggi è infragilita dalla crisi della rappresentanza. Con questo spirito abbiamo visto positivamente l'*election day*, perché legare alle elezioni europee, che purtroppo non entusiasmano (perché in questo Paese c'è un euroscetticismo che non ha prodotto partecipazione ma falsa informazione sulle ragioni dell'Unione europea), anche la europea), anche la votazione di migliaia di Comuni è un modo per concorrere a rafforzare la democrazia e la partecipazione. Poi però la maggioranza ha introdotto un tema un po' spinoso, quello dell'aumento del numero dei mandati. Anche in questo caso, noi non ne abbiamo fatto una questione di ragione di parte; abbiamo affrontato il tema dei sindaci con pragmatismo pragmatismo e chi fa politica sa che, per esempio, nei Comuni sotto i 5.000 abitanti è spesso molto difficile trovare candidati disponibili a ricoprire il ruolo di sindaco. Ci è quindi parsa improntata al buonsenso togliere il limite al numero dei mandati. Abbiamo anche condiviso l'aumento al terzo mandato per i Comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Per quanto riguarda il tema dei governatori, noi sicuramente non ci iscriviamo tra coloro che vogliono indebolire l'elettorato passivo; noi pensiamo che l'aumento del numero dei mandati dei governatori sia un tema serio, un tema serio, che non si può liquidare all'interno di un emendamento. Francamente, il dibattito in Commissione aveva portato ad una spaccatura interna alla maggioranza e alla bocciatura di quell'emendamento. Pertanto noi non abbiamo partecipato a quel voto, perché se davvero interessava a qualcuno all'interno della maggioranza portare a tre il numero dei mandati, serviva un *check and balance,* perché si tratta di una carica monocratica particolarmente incisiva, dotata di forti poteri. Se si vuole arrivare al terzo mandato, serve quindi un riequilibrio, con un protagonismo e un rafforzamento del ruolo delle assemblee elettive. Siccome, invece, ci è parso che al terzo mandato non fosse interessato nessuno all'interno della maggioranza, noi a questa contesa o a questa finta rappresentazione non abbiamo voluto partecipare, siamo disponibili, laddove la maggioranza davvero voglia riformare gli enti locali e magari il Titolo V della Costituzione, a ragionare delle 23 materie e di un rafforzamento delle assemblee elettive. Questo è un tema che abbiamo posto anche all'interno del premierato, perché rafforzare i poteri del *premier* e la stabilità del Governo ha un senso, non con il provvedimento che stiamo discutendo, ma è evidente che la centralità del Parlamento, l'abuso della decretazione d'urgenza, insomma una ridefinizione del ruolo del Parlamento, sarebbe ugualmente importante. Cosa c'è poi all'interno di questo provvedimento? Intanto si è cercato - e lo abbiamo respinto con perdite - di modificare le regole del gioco a gioco iniziato quindi non abbiamo consentito un esonero dalle liste delle firme che fosse fatto in modo da agevolare questo o quel partito. Ma il tema che a noi sta più a cuore è garantire a cittadini che sono per motivi di studio, di lavoro o di presa in carico di una persona, lontano dal luogo di residenza, di poter esercitare il diritto di voto. Alla Camera su questa battaglia le colleghe Pastorella e Grippo hanno lavorato a lungo. Purtroppo è stato approvato un provvedimento da parte della maggioranza che avrebbe avuto effetto alle calende greche. Al Senato con il collega Lombardo, la collega Versace, con Carlo Calenda abbiamo riproposto questo tema. La maggioranza si è ricreduta e mi fa piacere che all'unanimità in Commissione affari costituzionali sia passato almeno il diritto per gli studenti fuori sede di poter votare, ma la nostra battaglia andrà avanti perché noi troviamo che non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non comprendiamo perché chi lavora lontano da casa o chi si è preso in carico una persona non abbia lo stesso diritto degli studenti fuori sede di poter esercitare un diritto di voto. Poi ci lamentiamo dell'indebolimento della democrazia, dell'assenza di rappresentanza. Per queste ragioni noi ci asterremo, perché riteniamo che le regole del gioco si debbano scrivere insieme. Gli errori più gravi li abbiamo evitati, la battaglia sugli studenti fuori sede è andata in porto e ovviamente Azione continuerà per garantire il diritto di voto anche ai lavoratori. le elezioni rappresentano sicuramente la massima espressione di qualsiasi processo democratico. Negli ultimi anni però abbiamo assistito ad un vistoso calo della partecipazione da parte dei cittadini. Le ragioni sono molteplici. Probabilmente dovremmo cospargerci il capo di cenere un po' tutti quanti, perché il fatto di soffiare sul vento dell'antipolitica, la demonizzazione dell'avversario, giustamente hanno prodotto da parte dell'elettorato un allontanamento da quello che è un dovere, cioè l'espressione del voto. Naturalmente sono tutti fattori che hanno contribuito alla disaffezione e questo ha necessariamente causato nell'elettorato un distacco, un'evidente disaffezione. La storia, La storia, naturalmente, ci ha insegnato che non possiamo continuare su questo crinale. Dobbiamo invertire questa rotta, ma lo dobbiamo fare tutti quanti responsabilmente, tutte le appartenenze politiche.

come Capogruppo qui al Senato uno dei partiti storici della Repubblica italiana, uno dei partiti che dovrebbe generare un flusso di soluzioni delle problematiche

Il problema è proprio questo: tutti quanti dovremmo avere coscienza e non dovremmo meravigliarci della situazione attuale. Il nostro principale avversario è la gente che non vota. Noi dobbiamo ridare fiducia ai cittadini.

con l'obiettivo di diminuire questa disaffezione. L'esigenza di contrastare il crescente fenomeno dell'astensionismo, al quale assistiamo ormai da tempo, ci deve portare ad essere consapevoli che dobbiamo mettere in atto tutte le iniziative possibili per per facilitare l'accesso al voto di ogni cittadino, come fanno i provvedimenti che sono stati presi questa sera, come quello importantissimo e fondamentale che permette di votare

rappresentanza a livello parlamentare o a livello europeo. Sono tutte iniziative indirizzate verso un percorso fondamentale che è quello di restituire ai cittadini l'orgoglio della politica. Dobbiamo tutti quanti insieme fare in modo che questo avvenga al di là dei provvedimenti di questa sera,

Signor Presidente, colleghi, la recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 60 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna nella parte relativa al numero dei mandati per i sindaci. Nella sentenza si afferma che le autonomie speciali, pur avendo competenza primaria in materia di enti locali e delle relative circoscrizioni, sono sottoposte, in materia di mandati dei sindaci, alle disposizioni della legge statale, salvo che per particolari situazioni ambientali o condizioni peculiari locali del tutto eccezionali. Nonostante queste specificazioni, facilmente riscontrabili nel contesto della Regione Trentino-Alto Adige, la sentenza rischia di esporre i sindaci che sono in procinto di candidarsi per il terzo mandato a possibili ricorsi. In Trentino-Alto Adige infatti la legge elettorale per i Comuni fissa a tre il limite dei mandati. In particolare, se i prevedibili ricorsi dovessero essere accolti anche con ricorso indiretto alla Corte costituzionale, l'autonomia speciale della Regione Trentino-Alto Adige subirebbe un nuovo colpo a quegli *standard* di autonomia progressivamente svuotati dall'orientamento conservativo di numerose sentenze della Corte. È anche per ovviare a tutto ciò che in Commissione e in Assemblea abbiamo avanzato la proposta di elevare a tre il numero dei mandati per i Comuni con più di 15.000 abitanti. Ringrazio sul punto il Governo e la sottosegretaria Ferro per aver quantomeno accolto l'ordine del giorno con cui il Governo si impegna a tener conto delle specificità delle autonomie speciali rispetto al terzo mandato nell'imminente riforma del TUEL. del TUEL. La questione del terzo mandato non interessa tuttavia solo le autonomie speciali. Viviamo in un tempo in cui i cicli politici sono sempre più brevi e i cittadini sempre più orientati al cambiamento. Lo vediamo dai dati dei Comuni sotto i 5.000 abitanti dove, almeno sulla carta, il voto di opinione ha un peso minore. A dieci anni esatti dall'entrata in vigore della legge Delrio, appena il 14 per cento dei sindaci è al terzo mandato. Il terzo mandato insomma non è un elemento distorsivo rispetto al corretto funzionamento del processo democratico. I sindaci eletti per la terza volta sono percepiti come valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo della comunità. fatta però anche un'altra considerazione; con questa legge abbiamo giustamente esteso il terzo mandato per i Comuni fino a 15.000 abitanti. Ciò vuol dire che il 90 per cento dei Comuni italiani non avranno il vincolo dei due mandati. Il terzo mandato quindi non è più un'eccezione che riguarda pochissimi, ma un discrimine tra quel 40 per cento di cittadini che vive nei piccoli Comuni e l'altro 60 per cento che vive nei Comuni più grandi. Per tutte queste ragioni, Presidente, il nostro auspicio è che sul terzo mandato ci possa essere in futuro una riflessione libera da valutazioni e calcoli di parte. preservare un pezzo di classe dirigente che ben ha lavorato, che gode del sostegno dei cittadini, che può fare ancora tanto per la propria comunità. Inoltre, la possibilità di di una prospettiva quindicennale spingerebbe le amministrazioni a dare maggior peso ai progetti a medio e lungo termine e con un respiro strategico. Fare il sindaco non è un lavoro semplice. Comporta grandi responsabilità ed espone a tutta una serie di rischi, come in tanti hanno ricordato nel dibattito sull'abolizione dell'abuso d'ufficio. Soprattutto, non è un lavoro nel quale si può barare. I cittadini capiscono immediatamente se una Giunta sta lavorando bene o male. Per il resto, Presidente, questo è un provvedimento tecnico, su cui non c'è molto da aggiungere, se non nella norma per consentire il voto ai fuori sede, che andrebbe estesa anche agli studenti all'estero. È una norma molto importante, speriamo dia un impulso nella partecipazione al voto, nel contrasto all'astensionismo, che ormai è una malattia endemica della nostra democrazia. Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie ritiene che il provvedimento che ci accingiamo a votare sia comunque condivisibile, ma riteniamo, per le ragioni sopra esposte, che il tema dei mandati per i rappresentanti locali debba essere oggetto di un approfondimento. Per queste ragioni, il nostro voto sarà di astensione.

il decreto che abbiamo discusso fino ad ora, con un dibattito abbastanza articolato e impegnativo, avrebbe dovuto contenere esclusivamente la data per la indizione dei comizi elettorali: semplice, secco, tecnico. Invece, è diventato, nel tempo della sua permanenza in 1ª Commissione, un testo sul quale si è misurato anche un confronto fra le forze di maggioranza. Confronto, non scontro, perché ci hanno tenuto a chiarire che non hanno alcuno scontro al loro interno, ma che questa è stata l'occasione per un dibattito articolato per confrontarsi sui temi elettorali. Ammettiamo che sia effettivamente così, che questo sia stato un confronto dialettico,

così è successo. Nel momento in cui le stesse forze della maggioranza hanno deciso di introdurre nel testo determinati argomenti, va da sé, chiaramente, che la questione ha esposto i nervi, che sono più che scoperti su alcuni temi. Mi riferisco, ovviamente, alla questione del terzo mandato per i governatori regionali e alla questione del terzo mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. È davvero anomalo e, dal punto di vista normativo, contraddittorio

con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di non avere alcun limite e di poter essere rieleggibili *ad libitum*. Fintanto che agli elettori fa piacere, quel sindaco può essere rieletto.

A questo punto, non si capisce per quale motivo i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non possano godere di analoga previsione e facoltà.

a una cosa ancora più strana: il relatore ha dato parere contrario, mentre il Governo si è rimesso all'Aula: votate in scienza e coscienza e vedremo quello che succede. Chiaramente, è un modo per sfilarsi

a dire: ma noi siamo d'accordo; certamente il tema è importante e lo dobbiamo discutere, ma non è questa la sede per farlo. Peccato che la sede l'abbiate scelta voi; che lo abbiate messo voi questo testo; che l'abbiate infarcito voi di cose che non avevano motivo di starvi dentro quella norma che grida non dico vendetta, ma certamente grida aiuto di fronte alla Corte costituzionale, con la quale si è introdotta una nuova esenzione del tutto strana e molto particolaristica alle cause di ineleggibilità, ossia quelle disposizioni che prevedono che chi ricopre determinate cariche o impieghi o si trova in determinate posizioni non possa candidarsi alle elezioni se prima non si è messo in aspettativa, cioè se non ha fatto cessare quella condizione che comunque lo potrebbe astrattamente favorire in una competizione elettorale.

sempre in Commissione è stato presentato un emendamento che è stato accolto, quindi fa parte ormai del testo, con il quale si è disposto che i dipendenti regionali possono candidarsi senza doversi mettere in aspettativa e quindi non incorrono in ineleggibilità purché alla data di indizione dei comizi non svolgano funzioni amministrative. Quindi se lavorano nell'area tecnica, se sono impiegati in altre funzioni e mansioni ma non sono inquadrati nell'area amministrativa, amministrativa, allora non hanno bisogno di mettersi in aspettativa. Questo vale la possibilità di essere candidati e non incorrere nell'ineleggibilità. È evidente che questa è una norma personalistica. È evidente che abbiamo forzato un un dettato normativo e abbiamo violato il principio che vuole che la norma sia generale ed astratta *(Applausi)* e non può essere calata esattamente su un soggetto, chiunque esso sia. Non so chi sia, ma è chiaro e va da sé che è evidentemente calata su qualcuno.

ha previsto anche un'altra cosa veramente strana: in un momento in cui è sempre più difficile chiamare al voto gli elettori e avere la loro partecipazione, si dovrebbe favorire al massimo, in ogni sua forma e in qualsiasi modo la possibilità

che voleva togliere la possibilità di non dover raccogliere le firme a quei partiti che, pur avendo eletto dei rappresentanti e quindi pur avendo dei parlamentari eletti, non li avevano eletti al proporzionale, ma soltanto ai collegi uninominali. Che cosa avevano fatto di male questi partiti *(Applausi)* per meritarsi di non poter godere dell'esenzione della raccolta delle firme, che è nel testo della legge elettorale che vigeva fino a quando non è stato pubblicato questo decreto-legge? Cosa avevano fatto? Qual era il motivo? Non si sa. Fatto sta che dopo una vibrata protesta di alcuni movimenti politici, condivisibile perché questa è una norma francamente antidemocratica nel momento in cui cambi le regole del gioco a novanta giorni dalle elezioni

di piegare la normativa su qualcosa che va rimediato, sistemato, aggiustato, acconciato all'uso. L'uso è sempre prossimo: 30-60-90 giorni, come in questo caso. C'è un

le norme che consentono il voto agli studenti fuori sede. *(Applausi)*. Questo è veramente un traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme, ma non era previsto nel testo originario. Per questo dico che è un merito nostro, un merito del Parlamento, del Senato, non un merito del Governo, perché voi non lo avevate previsto. Avete fatto una legge delega che avrebbe rimandato ad altri cinque anni la soluzione di questa situazione e invece in Commissione - devo dire anche grazie a una direzione dei lavori da parte del presidente Balboni veramente oculata, intelligente e soprattutto partecipata - abbiamo finalmente introdotto le norme che consentono il voto agli studenti fuori sede. Certo, c'è il rammarico, Presidente - lo abbiamo detto prima nel corso delle votazioni degli emendamenti - che non altrettanto si è fatto per chi si trova fuori sede per motivi di lavoro. di lavoro. E non altrettanto si è fatto per chi si trova fuori sede perché magari è ricoverato in una struttura sanitaria o perché si è sottoposto a cure. *(Applausi)*. È un grande rammarico, perché questo penalizza prevalentemente gli elettori del Sud Italia,

Presidente, in realtà avendo già in sede di discussione generale spiegato le ragioni di una serie di perplessità e di contrarietà del mio Gruppo e della mia componente politica, avevo preannunciato la presentazione di una serie di emendamenti sui punti di criticità. Ovviamente, essendo stati

e partecipazione. È il frutto di un lungo e meticoloso lavoro, di un impegno che anche con la collega Ternullo come Forza Italia in 1a Commissione abbiamo portato avanti con dedizione e attenzione. Abbiamo sostenuto e promosso il diritto di voto per gli studenti universitari fuori sede, riconoscendo l'importanza di garantire a tutti i giovani italiani, ovunque si trovino, la possibilità di esercitare il loro diritto più sacro in democrazia. È un primo passo, come alcuni hanno sostenuto, ma concreto e significativo, che mai era stato compiuto. Meglio un primo passo, che in definitiva è sempre un passo in avanti, che un passo falso o un passo indietro. Il nostro lavoro non si è fermato qui. Abbiamo ascoltato le richieste e le esigenze espresse da ANCI e da UPI e in Commissione ci siamo battuti con determinazione per includere nel testo del disegno di legge modifiche fondamentali che rispondono alle richieste di enti così importanti. Questo impegno ha portato poi all'introduzione di ordini del giorno sulla tessera elettorale elettronica e quindi per ridurre l'uso della tessera cartacea e anche per impegnare il Governo a delineare chiaramente i poteri e le responsabilità dei sindaci e dei Presidenti delle Province, soprattutto in merito all'adozione delle ordinanze sindacali. Abbiamo anche portato avanti un emendamento che apre la porta a una maggiore inclusione, eliminando le barriere di ineleggibilità, incomprensibili per coloro che, svolgendo funzioni manuali o anche umili che non possono incidere sul voto, sono l'anima e il cuore pulsante della nostra società. Non è giusto che chi dedica la propria vita a servire gli altri, anche in ruoli a volte umili ma essenziali, come operai, operatori ecologici e molti altri, sia escluso dalla possibilità di rappresentare la propria comunità. Questa decisione incarna i valori di Forza Italia, un partito che crede nella dignità del lavoro, nella forza dell'inclusione, nella capacità di ogni individuo di contribuire al bene comune. In questo caso per l'emendamento c'è stata una forte opposizione, aspra e accesa, in Commissione solo perché il primo firmatario era il senatore Lotito, il quale ha il difetto - veramente ne ha tanti - di credere nelle proprie idee e di portarle avanti con molta determinazione

nel nostro percorso verso una democrazia più inclusiva, dinamica e rappresentativa. È con convinzione, quindi, che il Gruppo Forza Italia voterà a favore. Questo voto non Questo voto non è solo un segno di approvazione delle modifiche legislative proposte, ma rappresenta anche un impegno rinnovato verso i princìpi di libertà, uguaglianza e partecipazione su cui si fonda la nostra Repubblica. Il nostro voto a favore è un gesto di ottimismo verso le capacità del Paese di rinnovarsi e di affrontare le sfide che lo attendono. Per tutto questo, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il nostro voto favorevole. Signora Presidente, questo doveva essere - come ho detto in precedenza - un decreto-legge puramente tecnico per individuare le finestre elettorali dei tanti appuntamenti elettorali del 2024 e si è trasformato davvero in un vaso di Pandora in cui la maggioranza ha rischiato di rimanere risucchiata dalle proprie stesse contraddizioni. Cominciamo col dire che nello stesso testo del decreto-legge si prevede una normativa nuova per quanto riguarda il tetto ai mandati dei sindaci che molto probabilmente sarà incostituzionale. La Corte costituzionale si è già pronunciata rispetto all'innalzamento del tetto del mandato per i sindaci e lo ha fatto non settant'anni fa, ma meno di un anno fa, dicendo che quel limite ha un senso rispetto all'accentramento del potere e alle posizioni di rendita che ne che ne derivano da questo, per cui sconsigliando il legislatore di muoversi in tale direzione. Ovviamente la maggioranza ha fatto finta che la Corte costituzionale fosse quella di un altro Paese e non dell'Italia. È vero, infatti, che si riferiva alla Regione Sardegna; ma finché non avrete davvero attuato l'autonomia differenziata, la Sardegna è ancora Italia e, quindi, la Corte costituzionale vale in Sardegna e per tutto il resto del territorio italiano, finché rimane unito, come da auspicio

e quindi l'impossibilità di candidarsi per i dipendenti delle Regioni, improvvisamente meritasse un chiarimento; chiarimento che non aveva chiesto nessuno, perché non ci sono cause in corso, per cui questa oscurità l'ha vista soltanto qualcuno, probabilmente chi proponeva quell'emendamento che poi è stato approvato con grande sconcerto di tutta la Commissione, compreso il suo Presidente. Si afferma quindi che i dipendenti di Regione

anche attuali; quindi chi si è candidato in condizioni di incandidabilità, oggi, grazie alla norma che voi avete infilato nel decreto-legge in esame, si potrà trovare invece ad essere perfettamente eleggibile ed eletto risolvendo un suo problema personale, e non un problema del popolo italiano. un'altra meraviglia rispetto a questa previsione che avete infilato nel decreto-legge in esame. Istituite una disparità di trattamento tra i dipendenti dei Comuni, i dipendenti delle Province e i dipendenti delle Regioni: per i dipendenti dei Comuni e delle Province rimane vigente la legge così com'era,

comma 1, della nostra Costituzione, secondo cui tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Le condizioni di eguaglianza voi le avete abolite con questa porcheria *ad personam*. *(Applausi)*. Voi continuate a dire che non è *ad personam*, ma noi qualche nome in mente, anche non troppo lontano da Roma, ce l'abbiamo e questa è l'altra nefandezza che avete infilato. Poi avete cambiato le regole del gioco - peccato che la democrazia non è un gioco, ma è una cosa seria - a due mesi dalla scadenza elettorale delle europee. Che cosa avete fatto? Avete ristretto le condizioni per cui i partiti si possono presentare alle competizioni europee, complicando di gran lunga la situazione. Poi, evidentemente, presi da pentimento, avete allargato quelle restrizioni, per cui oggi chi deve raccogliere le firme non ne deve più raccogliere 150.000, ma 100.000. Peccato però che chi si stava preparando alle competizioni europee aveva già trovato una soluzione a norma vigente prima di questa roba che votiamo oggi. Non lo sapeva che voi avreste ristretto le firme a 100.000. Insomma, avete fatto un pasticcio inenarrabile inenarrabile e antidemocratico *(Applausi)* a due mesi dalla presentazione delle liste necessarie per competere alle elezioni europee. Per cui avete inficiato i rapporti democratici e la possibilità di partecipare democraticamente alle elezioni.

che continua a occupare i pensieri evidentemente della Lega e ne capiamo benissimo il motivo, perché hanno un problema in casa grande come una casa, anzi grande come una Regione, che si chiama Zaia. Non potete però portare i vostri problemi nell'Aula che rappresenta invece tutto il popolo italiano. *(Applausi)*. Dovreste essere in grado, da forze alleate che stanno al Governo insieme, di risolverli da soli e dietro le quinte, possibilmente. Invece, devo dire che la Commissione affari costituzionali è davvero un proscenio privilegiato, perché noi da lì vediamo davvero ogni spaccatura, che è enorme, all'interno delle forze di maggioranza. Non vanno d'accordo su nulla: sul premierato, sull'autonomia differenziata. È un disastro continuo e questo prima o poi sicuramente presenterà il conto. Non finisce qui, perché c'è stato il colpo di scena per l'Aula: la presentazione dell'emendamento che voleva addirittura abolire il ballottaggio per l'elezione dei sindaci e quindi chi arrivava al 40 per cento aveva vinto, con buona pace della democrazia e della partecipazione e chi s'è visto s'è visto, se magari alle urne ci è andata soltanto una piccola percentuale di popolazione. *(Applausi)*. Io ho sentito parlare proprio dalle file della maggioranza - sono sicura in buona fede, ma vi invito a riflettere - di antipolitica e avete detto che con questo-legge decreto voi combattete l'antipolitica e incentivate di nuovo le persone ad andare a votare. In questo decreto-legge si vede plasticamente una politica piegata su se stessa e dedicata anima e corpo a risolvere soltanto i propri problemi, i problemi che hanno anche nomi e cognomi specifici. Questo è proprio ciò che desta il sentimento dell'antipolitica, invece, negli elettori e nelle elettrici. *(Applausi)*. Voi li state allontanando, li state disgustando, perché davvero pensate soltanto ai problemi dei politici. Una cosa buona c'era in questo decreto alla fine: tramite emendamento della maggioranza siamo riusciti finalmente a consentire per queste elezioni europee agli studenti fuori sede di poter votare anche da fuori sede. Siamo molto felici e ci siamo tutti battuti per questo. Ho presentato disegni di legge già nella scorsa legislatura, ma una nota stonata la dobbiamo comunque denunciare. denunciare. In Commissione affari costituzionali solo la settimana prima ci eravamo sentiti la rampogna per cui era impossibile centrare quell'obiettivo. Non si sarebbe potuti arrivare alle elezioni europee consentendo agli studenti fuori sede di votare e, quindi, bisognava per forza accettare la delega al Governo. E voi avete trasformato il disegno di legge delle opposizioni in una delega al Governo, che ha detto che ci vorranno degli anni prima che si possa realizzare. Improvvisamente invece spunta poi l'emendamento dalla maggioranza che consente di votare in questa scadenza elettorale agli studenti fuori sede. Evviva, Evviva, però un po' di onestà intellettuale non guasterebbe davvero. conclusione, Presidente, è evidente che questo provvedimento, che doveva essere di una semplicità davvero banale, non è stato reso votabile dall'avidità

È una scelta che va fatta e va fatta anche nel prossimo futuro per due motivi: non solo per ridurre le spese, che sono comunque importanti per gestire le elezioni, ma soprattutto per cercare di non avere dei risultati in cui l'astensione è il primo partito nelle competizioni elettorali. Condividiamo poi la scelta importante di assicurare o di iniziare il percorso per concedere l'esercizio del voto per gli studenti fuori sede nelle elezioni europee. È già un buon punto di partenza; al di là di tutte le considerazioni che sono state fatte, il Governo e la maggioranza hanno trovato una strada percorribile per iniziare questa riforma. Arriviamo poi a un altro punto importante: la norma che contiene la riduzione dei limiti dei mandati dei sindaci. Anche questa è una battaglia

più importante del potere del popolo? Quello del voto. Attraverso il voto libero in democrazia si scelgono i propri rappresentanti e, quindi, noi non condividiamo la teoria secondo la quale l'esercizio del diritto di voto

Ci troviamo anche nettamente in disaccordo con il dibattito che è emerso, rispetto al quale la decisione di limitare il mandato di governatori e sindaci è legata al pericolo al pericolo che sindaci e governatori possano creare centri di potere, condizionare il voto ed esercitare una sorta di rendita di potere, d'accordo perché crediamo nella democrazia. *(Applausi)*. Crediamo che i cittadini votano i propri rappresentanti perché hanno fiducia in loro, perché hanno esercitato bene la cosa pubblica, hanno amministrato bene le risorse a loro disposizione e fornito servizi adeguati. Questo è il motivo per il quale sindaci e Governatori in una democrazia vengono votati dai cittadini, e non la visione distorta secondo la quale l'eletto è per forza una persona abietta che esercita il potere in modo distorto. Non ci troviamo assolutamente d'accordo; altrimenti passerebbe il principio secondo il quale dovremmo limitare i mandati dei sindaci e dei Governatori a un solo mandato, perché già dalla successiva competizione elettorale l'eletto dei cittadini potrebbe esercitare questa rendita di potere. Non siamo d'accordo. Questa non è una democrazia matura e noi riteniamo che in Italia esista una democrazia. i cittadini abbiano diritto di confermare i propri rappresentanti e che la politica e i partiti non possano esercitare il potere di limitare questa libertà. Ci sono sindaci e Governatori che vanno mandati a casa non dopo due o tre mandati, ma anche dopo il primo. Ma questa è una decisione che spetta al popolo. Non spetta ai partiti, non spetta alla politica e non spetta neppure alla Corte costituzionale, se mi permettete, perché le leggi le fa il Parlamento. Quindi, qual è la logica del secondo, terzo e quarto mandato? Ci sono

a geometria variabile, che noi non capiamo. Non ne capiamo le ragioni e, per tale motivo, siamo convinti che l'ultima parola debba aspettare sempre ai cittadini. Ricordiamo che il nostro concetto di democrazia è diverso dal vostro anche per passate riforme. Io non dimentico le riforme della sinistra democratica, che ha tolto il potere di voto ai cittadini per l'elezione dei propri rappresentanti nelle Province. Non dimentico le posizioni della sinistra democratica che voleva far eleggere o, meglio, nominare i senatori da parte dei consiglieri regionali. *(Applausi)*. Io queste cose non le dimentico. Per me questa non è vera democrazia. Non è il potere del popolo modo determina le elezioni dei propri rappresentanti. Quindi, noi non abbiamo alcun problema a combattere questa battaglia anche da soli, perché riteniamo che la democrazia vada difesa sempre e comunque. Il potere appartiene al popolo nell'elezione dei propri rappresentanti: che siano sindaci, Governatori, Presidenti di Provincia. Abbiamo una linea coerente. Siamo orgogliosi dei nostri amministratori sul territorio, che sono la forza della Lega anche in queste Aule parlamentari, perché, bene o male, ognuno di noi ha esercitato quell'incarico attraverso il voto dei cittadini. Riteniamo, quindi, che questo capitolo non sia chiuso. Per noi la questione è ancora aperta, soprattutto perché il Governo non ha dato parere negativo su questi emendamenti, quelli che abbiamo presentato. Quindi, c'è ancora la possibilità di arrivare ai cambiamenti che noi auspichiamo. In definitiva, noi esprimeremo un voto favorevole. Il dibattito che c'è stato ha messo in evidenza le diverse posizioni, le diverse concezioni rispetto alla democrazia. All'interno della maggioranza - ve lo dico chiaramente - non ci sono crepe. Noi non potevamo pretendere di imporre agli alleati di assumere le nostre posizioni, né loro hanno imposto a noi di fare abiura delle nostre legittime convinzioni. Vedremo se il Parlamento vorrà e potrà apportare le modifiche da noi auspicate. La strada è ancora lunga. Le decisioni sui mandati non si chiudono con questo voto. Le decisioni sui mandati non si chiudono con questo voto. In definitiva, noi siamo comunque soddisfatti di questo provvedimento e voteremo a favore.

abbiamo, sostanzialmente, solo convertito decreti-legge. Che ciò sia contrario ai limiti ai limiti che la Costituzione prevede, che ciò sia contrario alla consolidata giurisprudenza della Corte, che ciò sia contrario anche ai ripetuti moniti che diversi Presidenti della Repubblica hanno fatto, è cosa nota. Onorevoli colleghi, il fatto, però, che questa sia cosa nota e diffusa non significa che sia una pratica alla quale dobbiamo rassegnarci. rassegnarci. Il piano inclinato che in questa legislatura ha veramente toccato un fondo, che credo nessuno immaginava si potesse toccare, toccare, significa che il Governo ha esercitato il proprio indirizzo politico esclusivamente attraverso decreti-legge. È come se noi avessimo avuto, dall'inizio della legislatura ad oggi, un continuo ripetersi di casi straordinari di necessità e urgenza, perché questi sono i presupposti per l'adozione del decreto-legge. L'abuso della decretazione d'urgenza L'abuso della decretazione d'urgenza determina non soltanto una palese violazione delle prerogative del Parlamento e di quell'equilibrio tra i poteri che vede vede negli articoli 70 e seguenti della Costituzione attribuire al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa, in quanto organo direttamente espressivo della sovranità popolare. Il Governo a tutt'oggi non è direttamente eletto dai cittadini, poiché è espressione della maggioranza parlamentare, ma la maggioranza parlamentare che lo sostiene è stata espropriata delle proprie fondamentali prerogative. Sollevare questo tema non significa farlo a tutela

Corte, non violano solo e tanto le prerogative delle opposizioni, ma violano e mortificano le prerogative del Parlamento nel suo insieme, a partire da quelle della maggioranza ovviamente, che è chiamata soltanto a ratificare scelte che altrove vengono compiute. Dicevo prima che abbiamo toccato un fondo che non pensavamo di raggiungere, perché non soltanto i decreti-legge sono stati la regola, la norma, la modalità unica attraverso la quale il Governo ha legiferato, ma sono anche stati nella maggior parte dei casi decreti-legge palesemente eterogenei. Anche il limite, quello della omogeneità, è a tutela non delle opposizioni, ma delle prerogative del Parlamento e del buon funzionamento dell'attività di produzione normativa. Onorevoli colleghi, questa modalità di produzione del diritto, l'abuso di decreti-legge, alla fine produce anche cattiva legislazione: produce una legislazione frammentaria, incapace di affrontare in maniera organica e coerente i temi che pure meriterebbero di essere affrontati in questo modo. Anche nel decreto-legge in esame tocchiamo con mano cosa vuol dire dire affrontare il tema dei limiti ai mandati e il tema quindi dell'equilibrio che ci deve essere anche all'interno degli enti locali, tra funzione di rappresentanza e prerogative delle assemblee e funzione esecutiva dei sindaci. Abbiamo toccato con mano che viene inserito, all'interno di un decreto-legge che dovrebbe fissare la data delle elezioni elezioni e definire una data unica per le elezioni europee e amministrative, un articolo che rimuove ogni limite ai mandati per i sindaci nei Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Del merito abbiamo già detto. Questa disposizione - voi, onorevoli colleghi, e il Governo lo sapete bene - solleva più di un dubbio di legittimità, ma non perché l'opposizione sia per partito preso indotta ad evocare la Costituzione e la Corte costituzionale. Guardate che i limiti al potere della maggioranza sono posti a tutela di tutti i cittadini. Non so se

Colleghi, questi limiti non sono contro qualcuno, ma sono nell'interesse di tutti. Io vi chiedo di provare a liberarvi dall'insofferenza che manifestate in tutte le occasioni al rispetto di qualche limite, perché in un ordinamento costituzionale pluralista, in una democrazia liberale, la maggioranza non può tutto. Dove c'è la Costituzione, dove ci sono i diritti, dove c'è un'architettura costituzionale, la maggioranza incontra dei limiti e questi limiti vengono fatti rispettare dalla Corte costituzionale; è nella fisiologia, è nella normalità. Il continuo lamentarsi che ci sono dei giudici che fanno rispettare le norme costituzionali è incomprensibile. incomprensibile. Noi dovremmo essere tutti, invece, impegnati nel fare in modo che questi limiti siano il più possibile effettivi. È il dovere che ci accomuna.

ogni limite al mandato dei sindaci; un limite che - ripeto e lo abbiamo detto anche prima - è stato dalla Corte costituzionale, pochi mesi fa, considerato insuperabile, considerato insuperabile, e non perché la Corte costituzionale non si renda conto di quanto sia importante tutelare la libertà di voto dei cittadini, ma al contrario. Se noi leggiamo alcuni passaggi della sentenza, ci troviamo scritto che il limite in parola, cioè il limite ai mandati che una carica monocratica può ricoprire, ha lo scopo di tutelare il diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, sull'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio di potere e di gestione degli enti locali che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo. Serve a favorire il ricambio dei vertici dell'amministrazione, ad evitare la soggezione dell'uso del potere locale e, ancora, a evitare fenomeni di sclerotizzazione della situazione politico-amministrativa locale, soprattutto laddove - dice la Corte costituzionale si tratti di piccole comunità nelle quali le relazioni sono di prossimità e rispetto al voto di opinione prevale un voto di relazione. Lo dice la Corte costituzionale, e non lo dice il Partito Democratico. Onorevoli colleghi, ma è possibile

che guardi alle virtù, alle qualità dell'attuale legge e anche ai limiti che si sono palesati nel corso di questi trent'anni e farlo nell'interesse generale del Paese, nell'interesse generale del buon funzionamento degli enti locali, nell'interesse generale dei cittadini che dagli enti locali - lo sappiamo - ricevono prestazioni essenziali, e non avendo come unico obiettivo quello di determinare le sorti dell'uno o dell'altro? che noi ce l'abbiamo messa tutta per fare in modo che si aprisse un confronto di questo livello, ma avete persino respinto un ordine del giorno che si limitava a proporre di discuterne in maniera seria. Avete respinto anche questo, perché l'unica preoccupazione che anche in questo decreto, purtroppo, sembra caratterizzare l'azione politica del Governo è regolare micro-questioni, regolare i rapporti di forza all'interno della maggioranza. Ed è anche per questo motivo che noi siamo bloccati in Commissione su una proposta di riforma costituzionale insensata insensata e, a fronte di ore e ore di interventi, non c'è stato un solo esponente della maggioranza che si sia alzato a spiegare le buone ragioni della riforma,

nei confronti dei cittadini, perché il buon funzionamento delle istituzioni e la nostra capacità di operare in maniera equilibrata si ripercuotono sulla qualità della legislazione e, quindi, sulla qualità della vita delle persone che noi qui dovremmo rappresentare al meglio.

provvedimento interviene in maniera positiva su molti argomenti, istituendo delle misure che renderanno più partecipativo e più partecipato il voto delle prossime elezioni dell'8 e del 9 giugno. Il decreto-legge, ad esempio, stanzia risorse maggiori per i componenti dei seggi, ridando dignità anche al loro lavoro; sposta al 29 settembre il voto delle Province che altrimenti avrebbero votato in

però sono solo azioni a corollario di una misura più importante, quella che garantirà il voto dei nostri studenti fuori sede. Anche su questo punto siete arrivati secondi.

oggi questo piccolo passo - certamente si può fare ancora di più - diventerà realtà. Come dicevo prima, anche questo rientra nel novero del "potevamo farlo anche noi", che sentiamo spesso dire in questa legislatura. Evidentemente, mi sono convinto del fatto che noi siamo per voi quello che il genio della lampada è per Aladino: esaudiamo i vostri desideri. *(Applausi)*. Di conseguenza, vi conviene che si stia noi al Governo, in modo tale che riuscite ad approvare tutto ciò che vi piace,

di una vergogna da sanare. In questo provvedimento non c'è nulla di vergognoso: aumentare la partecipazione democratica è un fatto positivo, è un fatto costituzionale, è un fatto che aumenta la vicinanza dei cittadini alle istituzioni. in esame poniamo anche un freno alle cosiddette liste fasulle. Ho letto dei dati e alle scorse elezioni europee

libera partecipazione alle consultazioni elettorali, ma non dobbiamo neanche alterare le regole del gioco. Per questo, restringere l'ambito di chi può partecipare non avendo consenso ci sembra un fatto piuttosto naturale.

che cristallizza il *quorum* strutturale e funzionale delle elezioni dei Comuni sotto i 15.000 abitanti ed elimina le liste fittizie. Da questo punto di vista spero che la Camera faccia il prima possibile. Sul terzo mandato, per suo tramite, signora Presidente, vorrei ricordare al presidente Boccia che da questa parte dell'Emiciclo, soprattutto in quella che riguarda Fratelli d'Italia, non c'è alcun imbarazzo: noi abbiamo votato allo stesso modo in Commissione e in Aula. Chi ha avuto imbarazzo è stato il suo partito, che fino alla fine non sapeva se votare sì o votare no. Piuttosto che preoccuparvi del presidente Zaia, preoccupatevi allora delle telefonate e dei *tweet* di Emiliano, De Luca e Bonaccini che non avete saputo accontentare. Per venire al merito del terzo mandato, soprattutto con riguardo ai sindaci dei Comuni più piccoli, quelli sotto i 5.000 abitanti - ve lo dico per esperienza personale - la norma è logica, perché oggi è difficile

interessi e di rendite di posizione nei Comuni di 1.000, 2.000 o 3.000 abitanti, perché così non è; cosa che invece accade nei Comuni grandi e nelle Regioni laddove avete avuto il problema voi, perché laddove ci sono interessi il Partito Democratico ha dei problemi. Mi avvio alla conclusione, perché mi hanno anche chiesto di essere sintetico. Fratelli d'Italia voterà convintamente questo provvedimento, che dà regole migliorative per la partecipazione democratica e inserisce una misura importante come il voto degli studenti fuori sede e tante altre norme che garantiranno un corretto svolgimento per le elezioni dell'8 e del 9 giugno prossimi. È per questo, quindi, che dichiaro, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, il voto favorevole al provvedimento.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

La seduta è tolta